L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Sull'ordine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

Alberti Casellati, onorevoli colleghe e colleghi, prima di parlare oggi ho voluto ascoltare gli interventi dei colleghi dell'opposizione per comprendere il taglio che intendevano dare a questo importante dibattito politico sulla riforma costituzionale. Le confesso, Presidente, che sono rimasto piuttosto deluso. Mi è sembrato che i toni usati siano stati eccessivamente polemici e poco costruttivi. Ho sentito usare parole grosse e toni accesi, quasi apocalittici, ma nessuna autentica proposta alternativa.

anticostituzionale (è quasi un gioco di parole). Ho l'impressione, tuttavia, che si voglia contestare la riforma in modo aprioristico, non per il metodo con cui si propone di attuarla, ma addirittura per le finalità. Si dimentica però un dato di realtà. L'Italia è il Paese europeo in cui mediamente i Governi durano di meno.

Ormai, da oltre trent'anni diversi Governi e diverse maggioranze di tutti i colori politici che si sono alternati alla guida del Paese hanno intrapreso tentativi di riforma costituzionale.

Sorte analoga è toccata alla riforma voluta dal *premier* Renzi nella XVII legislatura: anche quella riforma non ha superato il vaglio del *referendum* popolare. Questi dati storici ci servono per confutare la prima delle obiezioni che ho sentito formulare in Aula in questi giorni di dibattito. Mi riferisco alla tesi secondo cui la nostra è la Costituzione più bella del mondo, nata dalla Resistenza al nazifascismo, e quindi non ci sono motivi per modificarla. In realtà, tutti i motivi di riforma che si sono succeduti nel tempo avevano la finalità di rafforzare l'Esecutivo e dimostrano che l'opzione per Governi strutturalmente deboli, nata all'indomani del secondo conflitto mondiale e dopo la fine della dittatura fascista, scelta perfettamente condivisibile quando venne promulgata nel 1947, non è più rispondente alle esigenze del tempo presente. Talune di queste proposte prevedevano addirittura un sistema presidenziale con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ricordo a tal proposito la proposta della Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole d'Alema. Tutti i Presidenti del Consiglio che si sono succeduti in questi decenni hanno ritenuto assurdo quanto previsto attualmente, cioè di non poter sostituire un Ministro del loro Esecutivo in modo autonomo, quindi, colleghi, se anche la sinistra, quando è stata al potere in questo Paese, ha avvertito l'esigenza di modificare la Costituzione, non deve considerarsi un sacrilegio o un attentato alla democrazia mettere mano da parte di un Governo di centrodestra alla seconda parte della nostra Costituzione. Una seconda questione che ho avvertito nel dibattito è relativa al modo in cui la nuova configurazione del Presidente del Consiglio, per effetto della sua elezione diretta, si riverbera sul ruolo e sui poteri del Presidente della Repubblica. Secondo gli esponenti dell'opposizione, con questa riforma il ruolo presidenziale sarebbe gravemente sminuito e ridimensionato. Mi pare anche questa una critica infondata e forzata. In realtà i poteri presidenziali restano sostanzialmente inalterati. Gli unici marginali interventi di riforma riguardano l'abolizione dei senatori a vita e la conseguente prerogativa presidenziale e il potere di sciogliere una sola Camera anziché entrambe. Si tratta in effetti di aspetti di mero dettaglio che non incidono sulla sostanza. L'elezione diretta del *Premier* vincola piuttosto il Presidente della Repubblica nell'affidamento dell'incarico al *Premier* votato e questo è certamente, se vogliamo, l'aspetto più delicato. Si tratta tuttavia di un adeguamento della Costituzione formale a quella materiale. Già oggi, quando dalla consultazione elettorale emergono una indicazione chiara del *leader* e di una maggioranza di Governo, com'è avvenuto peraltro nelle più recenti elezioni, il Presidente della Repubblica non può che prenderne atto. In questo modo però, a giudizio di chi parla, non si rafforza e non si indebolisce, ma anzi si rafforza la democrazia del nostro Paese, non nella logica del plebiscitarismo e dell'autoritarismo, come errando hanno affermato le opposizioni, ma piuttosto nella logica della democrazia dell'alternanza. Purtroppo, l'odierno disincanto e l'allontanamento dei cittadini rispetto alla politica, testimoniati in particolare dalla bassa, talvolta bassissima, affluenza ai seggi durante le consultazioni elettorali, sono in larga misura dovuti alla percezione, vera o presunta, dell'indifferenza della politica al rispetto della loro volontà. Questa riforma, invece, attribuirà certamente centralità alla volontà democratica dei cittadini e io credo rafforzerà la sensazione del cittadino elettore di contare davvero nelle decisioni che riguardano il futuro del Paese e la selezione della sua classe dirigente, riavvicinandolo alle istituzioni. La riforma che stiamo discutendo si ispira peraltro a quella che, a detta di tutti, ha funzionato meglio negli ultimi decenni: l'elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti di Regione. Il *Premier*, che questa riforma propone, è proprio una sorta di sindaco d'Italia. Ammetto, Presidente, di non poter vantare il *copyright* di questa definizione. In realtà è stato il senatore Renzi il primo a parlare, qualche stagione fa, di sindaco d'Italia, ma è una formula che giudico felice e per questo oggi mi sento di rilanciarla. Tutto questo per riaffermare il concetto che, a tempi alterni,

Tra gli argomenti critici esposti in questi giorni, c'è anche quello secondo cui questa riforma sarebbe frutto di una sorta di *pactum sceleris* tra Lega e Fratelli d'Italia, per un baratto tra autonomia e premierato. Al netto del fatto che l'autonomia differenziata altro non è che una legge ordinaria attuativa di una riforma costituzionale votata dalla sinistra nell'ormai lontanissimo 2001, mi sento oggi autorizzato a replicare, in particolare al Partito Democratico e ai suoi esponenti, che altri e più gravi baratti sono stati attuati negli anni passati ai danni della cosiddetta Costituzione più bella del mondo. Ricordo che nella scorsa legislatura il Partito Democratico non ha esitato a votare a favore dello scellerato (quello sì) taglio dei parlamentari, di cui tutti oggi in questo consesso ci lamentiamo, qualcuno pubblicamente - come il sottoscritto, che quel taglio non ha votato e che contro quel taglio ha fatto campagna elettorale referendaria - altri colleghi sottovoce e con tono confidenziale. Pur di entrare al Governo con i 5 Stelle, il PD ha cambiato, tra la prima e la seconda lettura del testo costituzionale, dalla sera alla mattina, *d'emblée*, il voto da negativo a favorevole. Dopo Dopo questo increscioso precedente, di lezioni di coerenza in materia costituzionale il Partito Democratico non è certamente in grado di impartirne. Azzardo infine una previsione. Sono convinto che, se su questa riforma costituzionale che, se su questa riforma costituzionale si dovrà alla fine celebrare un *referendum*, questo vedrà un esito positivo. Cercherò di spiegare perché. Entrambe le riforme costituzionali volute prima da Berlusconi e poi da Renzi non hanno superato il vaglio del *referendum*. Erano riforme probabilmente più ambiziose di questa, quanto a contenuti, ma avevano un difetto: apparivano agli elettori confuse e poco chiare quanto alle finalità. Troppe cose dentro, troppi cambiamenti. Questa riforma invece è - come dire - *pop*. Il suo contenuto è molto chiaro: significa attribuire al cittadino elettore la possibilità di scegliere direttamente chi sarà il *Premier* e la coalizione di Governo. Eviterà trasformismi e odiosi ed inspiegabili cambi di casacca, le furbizie italiche che tanto indignano l'opinione pubblica. Il cittadino, di fronte alla scelta semplice che gli verrà posta, a mio giudizio non avrà esitazione ad approvarla. Quanto alla legge elettorale, credo sia stato giusto escluderla dalla riforma costituzionale e rinviarla alla legge ordinaria. Le questioni sul tappeto sono numerose, segnalate anche sulla stampa da acuti studiosi della materia. Ci sarà tempo per approfondirle, evitando storture e cercando di rispettare, anzi rispettando certamente i principi sanciti già in altre occasioni dalla Corte costituzionale in materia elettorale. Ho cercato di inserire in questo dibattito, che mi è parso talvolta parossistico, qualche spunto pacato di riflessione. Spero serva ad attenuare i toni di confronto esasperato, che non giova certamente alla nostra democrazia,

inquieta constatare che, dopo quarant'anni di sforzi per dare all'Italia forme di governo più stabili, sia stata prodotta una proposta invotabile e persino inemendabile. Non c'è da considerare solo la sua inadeguatezza tecnica - lo hanno detto tanti colleghi dell'opposizione che hanno parlato prima di me - ma anche il suo palese contrasto con i principi che reggono le basi della nostra stessa democrazia rappresentativa. C'è un preciso disegno politico alla base di questa proposta: smantellare il nostro sistema istituzionale per schiacciarlo sul leaderismo che mina i capisaldi della nostra Costituzione. Al contrario di quanto affermato da qualche commentatore, infatti, il nostro non è un mero costituzionalismo ansiogeno, ma si basa su considerazioni concrete e altrettanto concrete preoccupazioni per il futuro del Paese. Facciamo un passo indietro su quello che è accaduto in queste settimane. Avete proceduto con i lavori in Commissione senza ascoltare le nostre richieste, sordi a ogni nostro tentativo di proposta e condivisione. che dice che l'opposizione non ha fatto nessuno sforzo e nessuna proposta. Basta essere andati in Commissione: il Partito Democratico, ascoltando anche il monito che è arrivato da gran parte dei costituzionalisti in audizione, attenti alla Costituzione, ha tentato di approfondire e far emergere tutte le contraddizioni contenute nel disegno di legge, spiegando gli effetti negativi della proposta di riforma. Nel corso dei lavori in Commissione, attraverso l'illustrazione degli emendamenti, non vi è stata alcuna risposta da parte della maggioranza, perché evidentemente il testo non può essere modificato, essendo parte dello scambio - sì, di questo tra autonomia differenziata e premeriato, concluso tra due delle forze politiche che sostengono questo Governo. Diciamolo con chiarezza: non si può riscrivere la Costituzione per volere di un capo politico. È inaccettabile procedere senza il pieno coinvolgimento del Parlamento e di tutte le forze politiche. Per questo, la settimana scorsa avevamo chiesto, con la nostra questione pregiudiziale, di non procedere alla discussione generale. A differenza vostra noi non abbiamo avuto alcuna paura del confronto qui in Aula. Voi avete scelto il silenzio, ma ci avrebbe fatto molto piacere ascoltare le vostre argomentazioni, quella di ognuno di voi, perché ci ascolta il Paese, perché siamo i costituenti di oggi. volete modificare la grammatica costituzionale e avete rinunciato all'ascolto e al confronto; dall'altro, ci accusate spesso di ostruzionismo, di far perdere tempo, solo perché abbiamo scelto di parlare, di argomentare e di non tacere. Eppure, siamo contenti che ieri il senatore Malan ci abbia detto che molti di voi si sono iscritti oggi per argomentare e discutere la riforma costituzionale, perché noi saremo qui ad ascoltare. Noi non abbiamo paura, appunto, del confronto e dell'ascolto, perché siamo sicuri delle nostre opinioni. Siamo ben certi del disastro istituzionale che si verrebbe a creare con l'approvazione di questa legge. Avevamo chiesto di non procedere all'esame del disegno di legge costituzionale, perché è fin troppo evidente che state utilizzando le istituzioni repubblicane per un fine politico, in piena campagna elettorale. Signora Presidente, vengo ai contenuti della proposta oggi in discussione. Com'è stato espresso molto chiaramente e a più riprese da esperti costituzionalisti, giuristi e politologi, esistono svariate argomentazioni in opposizione a questo disegno di legge costituzionale, che, partendo da un punto di vista strettamente tecnico, arrivano a minare la nostra stessa democrazia. Vorrei concentrarmi su alcuni punti, cinque in particolare, a nostro avviso esplicativi per rendere irricevibile la sostanza e il merito del testo di revisione costituzionale deliberato dalla 1a Commissione. In primo luogo, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio costituirebbe un *unicum* - l'hanno detto tanti altri miei colleghi - nella storia delle Costituzioni contemporanee, nonostante esistano svariati regimi presidenziali e semipresidenziali, però disciplinati con opportuni e robusti contrappesi. Nessuno ha pensato ad una forma di governo come quella proposta, perché è giustamente percepita la pericolosità di affidare a una persona sola per lunghi periodi di tempo un'abnorme concentrazione di poteri cruciali. Si pensi a quale accentramento si creerebbe nella guida, per esempio, delle relazioni internazionali, della sicurezza, della difesa, dell'economia, della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario; una condizione di squilibrio gravissima, acuita dalla riduzione dei poteri del Parlamento, già oggi spesso ridotto a mero redattore di decreti impacchettati e soprattutto del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Passo al secondo punto, Presidente. Con la proposta di modifica costituzionale che stiamo appunto discutendo, il Capo dello Stato non perderebbe solo il potere di nomina dei senatori a vita e la scelta di un Presidente del Consiglio, eventualmente al di fuori dei parlamentari, bensì, nell'ordine: non potrebbe più sciogliere in modo anticipato una Camera; si vedrebbe incredibilmente limitato il potere di nomina del Presidente del Consiglio e quello di scioglimento delle Camere, che sembrerebbe vincolato a situazioni specifiche prestabilite, in un certo senso vincolate e obbligate. Ancora, potrà proporre la revoca dei Ministri, ma niente è stato chiarito sul ruolo di guida e coordinamento degli Se ci fosse la necessità di sciogliere in modo anticipato le Camere per gravissimi motivi istituzionali o politici? Il Presidente della Repubblica avrebbe perso questa prerogativa importantissima per il ruolo di garante dello Stato. poi un terzo argomento di forte critica che non posso non rilevare. Con il sistema proposto dal Governo si indeboliscono gli strumenti della democrazia rappresentativa, perché, al contrario di quanto questo Governo continua a rivendicare sempre a mo' di bandiera, il corpo elettorale avrebbe possibilità di scelta solo con un'unica votazione maggioritaria ogni cinque anni e deciderebbe sulle proposte dei vertici del sistema politico senza avere successivamente modo di manifestare il suo giudizio e la sua volontà popolare. Lo traduco: rimuovendo il fumo negli occhi che si continua a gettare sui cittadini e sulle cittadine di questo Paese, l'elettorato vedrebbe ridotti i propri poteri. Inoltre, irrigidire il testo costituzionale con una scelta così specifica in termini di legge elettorale con un sistema maggioritario suscita quantomeno uno scrupolo anche derivato dal realismo e dall'esperienza: stabilire regole ferree per evitare che si verifichino manifestazioni patologiche dell'Esecutivo e del legislativo (instabilità o fluidità delle maggioranze) può essere controproducente, perché la rigidità è appropriata a situazioni precise e prestabilite, mentre la realtà (e la storia dei nostri Governi di questa Repubblica lo dimostra) è spesso mutevole e anche imprevedibile. Su questo, riferendoci all'eccessiva importanza attribuita alla figura del *leader,* quasi prescente di alcuni aspetti della proposta di modifica costituzionale che stiamo discutendo, Stefano Rodotà, audito nel 1997 dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura, offriva in prospettiva una riflessione sensata: si dice che bisogna scegliere un determinato *leader* perché altrimenti non si vincono le elezioni; quel tipo di *leadership* rispetto alla quale la coalizione sfuma e il *leader* soltanto è la condizione di successo indica però una debolezza che si trasferirà poi alla coalizione in Parlamento. In risposta a una provocazione diceva che, al contrario, la coalizione riconosciuta e la *leadership* attribuita al rappresentante del Gruppo del partito più forte è proprio la condizione perché in Parlamento vi sia maggiore stabilità. Con la vostra proposta si aggiunge un altro problema: qualsiasi uomo o donna fosse candidato alla Presidenza del Consiglio, e quindi dovesse assicurare per sé il massimo numero dei voti e anche la piena fedeltà dei parlamentari eletti a lui o a lei collegati, non spingerebbe forse per avere influenza sulla composizione delle liste elettorali, riducendo quindi così le scelte autonome dei partiti, delle sezioni territoriali, dei cittadini e delle cittadine elettori? Passerei al quarto punto, ovvero a un altro tormentone di questo Governo, probabilmente inserito per limitare i cosiddetti giochi di palazzo, con questo termine che sempre utilizzate

tra i partiti di maggioranza, come ci ha fatto notare l'onorevole Anna Finocchiaro nelle audizioni: essa non può che accendere aspirazioni competitive tra i *leader* delle forze della coalizione, promuovendo i giochi politici interni alla maggioranza e facendo decadere così l'assioma che collega la stabilità di Governo all'elezione diretta. Il soggetto forte va infatti individuato nel potenziale successore del Presidente eletto, perché è proprio il successore che detiene il potere di ricatto consistente nella reale possibilità di condurre allo scioglimento delle Camere. La stessa previsione costituzionale di questo secondo Governo è, infatti, un potenziale incentivo ad impiegare l'istituto e quindi a caratterizzare di instabilità il Governo precedente, pure eletto. Peraltro ed è bene farlo notare - bisogna tornare al periodo fascista per trovare l'unico precedente di questa bizzarra formula: era infatti previsto dall'articolo 13 della legge 2693 del ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo, che consegnò il Governo nelle mani di Badoglio dopo la rimozione di Mussolini. In secondo luogo, il Presidente è in grado di avere il voto di fiducia anche delle forze precedentemente all'opposizione, alle quali nessuna norma costituzionale può vietare di scegliere liberamente come esprimersi in sede parlamentare. Vorrei ora passare all'ultimo punto e accingermi alle conclusioni, signor Presidente. Con il presente disegno di legge costituzionale si pongono le premesse per un'ulteriore espansione dei poteri governativi a scapito della competenza Infatti, come accennavo prima, se uno dei maggiori problemi attuali consiste nella troppo accentuata influenza del potere esecutivo sulla produzione legislativa - si pensi a tutte le polemiche sugli atti con forza di legge, sull'abuso di voto di fiducia, sulle leggi e sui macroemendamenti, sui DPCM una riforma costituzionale come quella proposta si pone in piena contraddizione con le auspicabili tendenze a far recuperare al Parlamento il suo potere legislativo. Con questi argomenti, Presidente, ho cercato di spiegare le ragioni della nostra contrarietà.

Con l'autonomia differenziata volete distruggere l'unità del Paese, aumentando il divario territoriale e le diseguaglianze economiche e sociali non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centro e periferia e tra Capoluoghi all'interno di ogni Regione. Con il premierato, neutralizzate le funzioni del Presidente della Repubblica e del Parlamento per accentrare i poteri nelle mani del Presidente del Consiglio. Il mio Il mio appello è alle forze parlamentari di maggioranza: fermatevi, fermate questa riforma pericolosa per la nostra democrazia, tornate a pensare ai problemi delle persone e delle famiglie italiane, al lavoro, all'inflazione e agli aumenti del costo della vita. Vi state avvitando dentro riforme sbagliate per consegnare un po' di potere in più nelle mani di Giorgia. Non lo consentiremo, ci batteremo per fermare questa deriva e riaffermare i valori della nostra Costituzione scritta da donne e uomini che hanno avuto il sogno di consegnarci non una Carta, Presidente, ma valori, principi, buon funzionamento della democrazia e alta qualità della partecipazione.

gentile Ministra, gentili colleghe e colleghi, non volevo parlare perché in quest'Aula è stato detto tanto e bene, in maniera precisa e argomentata, in tutti i toni,

e, se c'è una cosa che nella mia vita ho saputo fare o quantomeno ho fatto per diciassette anni prima di rappresentare i cittadini in questo Parlamento, è insegnare.

Sapete quando la repubblica, ai tempi dei romani, si trasformò in impero? Intanto, dobbiamo ricordare che la repubblica romana era un sistema perfetto: c'erano due consoli che avevano il potere esecutivo; c'era il Senato, che aveva il potere elettivo, appunto di eleggere i consoli; e poi c'erano i tribuni della plebe, che avevano il compito di censurare, il compito di veto. Era un sistema equilibrato che funzionava, ma che cos'è accaduto a un certo punto? A un certo punto, la repubblica è diventata talmente vasta che andava gestita bene, la corruzione è esplosa e il popolo ha cominciato a pensare che forse era più opportuno che ci fosse solo una persona a gestire il tutto piuttosto che un sistema così complesso, completo, equilibrato e funzionante. E allora qualcuno pensò di poter ardire, con la sua presenza, di sostituirsi al potere del Senato, dei consoli e dei tribuni della plebe. Chi era questa persona? Giulio Cesare.

se li fece consegnare su un piatto d'argento. Sapete da chi? Dai senatori, dicendo loro: io non voglio i pieni poteri, voglio solo proteggervi, voglio solo fare in modo che la *res publica* possa funzionare. I senatori vollero credere a Ottaviano, a differenza dello zio, e gli consegnarono pieni poteri. Ottaviano, che poi si chiamò Ottaviano Augusto, fece un uso meraviglioso di quei poteri. Ricordiamo tutti la *pax augustea*.

Il governo di Augusto fu un ottimo governo. Egli non volle mai essere chiamato imperatore, ma solo *princeps*. Attenzione, perché in questa fase di transizione, con un Senato quasi orgoglioso di aver dato a Ottaviano ciò che aveva negato a Cesare, addirittura uccidendolo, Augusto è cominciato l'impero. È finita la *pax augustea* e abbiamo avuto Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Vespasiano, Tito, Domiziano, eccetera. Questa Questa è una fase storica e vado indietro, a Polibio e a quella che la storiografia ci insegna come l'evoluzione ciclica dei regimi politici e delle loro degenerazioni.

dare lezioni a questa maggioranza, così sicura e arrogante. Arrogante, sì, perché una riforma costituzionale, a mio avviso, avrebbe bisogno di una valutazione molto più profonda. Non invito ad ascoltare noi del MoVimento 5 Stelle, ma forse il confronto con grandi costituzionalisti, anche con grandi storici, sarebbe stato opportuno. Scusate questo retaggio della mia vita di prima, ma dopo diciannove anni tra i banchi di scuola è più forte di me. riesco a guardare tutto attraverso le materie che ho insegnato e quindi attraverso i grandi che mi hanno insegnato qualcosa. Almeno, loro ci hanno provato, io non so cosa sono riuscita a estrapolare e recuperare. Vi chiedo, però, una cosa. Facciamoci delle domande. In questo contesto,

Bisogna quindi rafforzare i poteri di un Presidente che ha già quasi i pieni poteri? No. Il Parlamento, quindi noi, abbiamo poteri sufficienti? Siamo sufficientemente forti? Noi riusciamo a legiferare? No. Quindi qual è il potere che andava rinforzato? Quello del Parlamento, se si voleva in qualche modo incidere, non certo quello del *Premier*. *(Applausi).* Il Presidente della Repubblica è stato di garanzia? È un pilastro per questo sistema delicato ed equilibrato, che i costituzionalisti, non certo Barbara Floridia, sono capaci di spiegare? Sì, lo è stato. Perché trasformarlo in passacarte? Vi un'ultima domanda. In questo momento storico, pensando al passaggio dalla Repubblica all'impero, pensando ai cicli di Polibio, alle degenerazioni dei regimi politici, secondo voi siamo in un momento in cui il tasso, il livello di corruzione, la paura delle persone e il contesto geopolitico possono condurre a quell'errore storico? Sì o no? Per me sì, ma non per me, per la storia sì. Io non dubito, o meglio, non voglio dubitare delle nobili intenzioni. Immagino che le vostre intenzioni siano nobili, ma attenzione che non accada come è accaduto con Ottaviano Augusto con la *pax au-gustea*. Le intenzioni di Augusto erano nobili e hanno anche funzionato durante il suo regime, dopo non In conclusione, Presidente, colleghi, non ascoltate me, non ascoltate il MoVimento 5 Stelle, non ascoltate l'opposizione; del resto non lo fate mai, perché lo dovreste fare proprio questa volta?

ieri - come credo molti colleghi - sono rimasto profondamente colpito dalle parole della senatrice a vita Liliana Segre. dal complesso del suo intervento, ma soprattutto da tre moniti che, con la sua saggezza, Liliana Segre ha voluto lanciare al Governo, alla maggioranza e a tutti noi. Mi riferisco alla parte del suo intervento nella quale la senatrice a vita ha invitato il Governo e la maggioranza a evitare prove di forza, sperimentazioni temerarie temerarie e scelte avventurose. Io credo che dovreste prendere molto sul serio queste parole, perché nella vostra riforma ci sono scelte avventurose e sperimentazioni temerarie. E, nel modo in cui avete portato avanti questo tentativo di riforma, c'è stata la ricerca continua delle prove di forza. forza. La ricerca continua delle prove di forza è l'altra faccia dell'ostinato rifiuto di dialogare realmente con l'opposizione, come invece bisognerebbe fare quando ci si accinge a cambiare la Costituzione, e soprattutto se si cambia la Costituzione nella sua Parte II, che riguarda il modo in cui le nostre istituzioni sono organizzate. Il rifiuto del dialogo è di per sé un grave limite dell'operazione riformatrice che avete messo in campo. Io spero che nei prossimi mesi possiate rendervene conto più di quanto non sia avvenuto nei mesi scorsi. Durante cinque mesi di dibattito in Commissione, quasi ogni giorno, vi abbiamo invitato a prendere in considerazione i campanelli di allarme che abbiamo fatto suonare con molta responsabilità, sottolineando quali erano i punti che assolutamente non andavano bene del disegno di legge che stavamo trattando. Fino a questo momento i nostri appelli alla ragionevolezza sono caduti nel vuoto. Siete andati avanti come rulli compressori e siete riusciti a confezionare una proposta che non sta in piedi da nessun punto di vista. Uno dei

negli anni Settanta dette una lezione mai più dimenticata sul fatto che le forme di governo, cioè il modo in cui in un ordinamento sono distribuiti i poteri tra gli organi di vertice, non vanno tanto distinte tra forme di governo parlamentari, presidenziali, semipresidenziali. La prima distinzione che bisogna fare è tra le forme di governo che hanno il pregio dell'equilibrio e della flessibilità, dell'elasticità e quindi della resilienza, e le forme di governo che invece hanno il difetto dello squilibrio e della eccessiva rigidità. Voi avete confezionato una proposta che ha come principale difetto quello di consegnare tra i poteri dello Stato una situazione di squilibrio assolutamente fuori dalla norma, eccessiva, estremamente rischiosa. Quel che mi sembra non riusciate a capire - lo noto da alcuni interventi che caratterizzano la vostra presenza nel dibattito pubblico

Unito e della Spagna - è in realtà il "melonato", che è un'altra cosa, e cioè è una deformazione del premierato con una versione all'italiana che non ha eguali nel mondo e non sta in piedi, non regge. In

«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Cosa ci dice l'articolo 2 della nostra Costituzione? Ci dice che l'Italia è una Repubblica che si basa sulla volontà popolare, ma prevede che la sovranità popolare tenga conto delle forme e dei limiti in cui questa può esercitarsi secondo il dettato costituzionale. Ci dice cioè - è la lezione di tutto il grande costituzionalismo liberaldemocratico - che una buona democrazia è tale se esistono al suo interno equilibrio tra i poteri, tra Governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, e una rete una rete valida di contrappesi, limiti e controlli che impedisca che ci sia un abuso e un'esondazione di uno dei poteri a danno degli altri, e particolarmente una rete di controlli e di contrappesi che impedisca le prevaricazioni del potere esecutivo. Una democrazia sana è fatta di questo. E quella che si determinerebbe se questo disegno andasse in fondo sarebbe una democrazia malata, di qualità assai inferiore a quella che abbiamo oggi, proprio per il dato abnorme degli squilibri che si creano tra Governo e Parlamento, da una parte, e tra Governo e Presidente della Repubblica, dall'altra; o per meglio dire: tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, e tra Presidente del Consiglio e Parlamento. e Parlamento. Noi non siamo conservatori ed abbiamo una nostra proposta di riforma delle istituzioni; l'abbiamo presentata più volte e guarda alle migliori forme di governo europee, che ho citate prima: la Germania e la Spagna in primo luogo. Non siamo piatti difensori dello *status quo*. Una riforma costituzionale oggi dovrebbe tener conto non degli *slogan* e della propaganda, ma della situazione reale in cui ci troviamo. Oggi noi viviamo in un Paese in cui il Parlamento è già straordinariamente debole e schiacciato dal potere esecutivo. Basta fare il conto dei decreti-legge che sono stati approvati dall'insediamento di questo Governo. Ci era stato promesso che, essendo il Governo con la più ampia maggioranza parlamentare da molti anni a questa parte, si sarebbe fatto un uso moderato di decreti-legge. Ebbene, si è fatto un uso dei decreti-legge che è il più grande da quando questo strumento esiste e non c'è alcun indizio che vogliate rallentare, anzi, probabilmente ci sarà un'accelerazione. L'abuso dei decreti-legge è conclamato

che purtroppo ha queste caratteristiche. Pertanto, insieme a quella sulla stabilità dei Governi, ci sarebbe dovuta essere una preoccupazione per un rafforzamento della dignità e dell'autorevolezza del Parlamento. Questa preoccupazione non c'è stata e, anzi, la cancellazione - direi sostanziale - dell'autonomia del Parlamento che questo disegno di legge si porta dietro è uno dei fatti più gravi su cui dobbiamo porre l'attenzione. Perché parlo di mortificazione dell'autonomia del Parlamento? Questa mortificazione deriva da una serie di disposizioni. La prima è gravissima: come in questi giorni molti hanno ricordato, diventeremo l'unica democrazia del mondo nella quale il Parlamento è eletto in maniera non indipendente e non autonoma. Non c'è al mondo una democrazia in cui il Parlamento sia eletto subordinatamente al potere esecutivo; non c'è nessuna democrazia parlamentare che sia così, non c'è nessuna democrazia presidenziale o semipresidenziale che sia così. Per questo noi accogliamo con un sorriso Per questo noi accogliamo con un sorriso le parole del Governo quando ci dice che aver abbandonato l'ipotesi presidenzialista e aver messo in campo questo disegno di legge è stato un passo verso le opposizioni. È stato un passo in direzione opposta, perché questo sistema è molto peggio del presidenzialismo o del semipresidenzialismo, che pure non ci piacciono. Infatti, lo squilibrio di poteri che genera e la mancanza di contrappesi che ha sono molto più gravi di quelli dei sistemi presidenziali e semipresidenziali. L'elezione a strascico del Parlamento, quindi, produce l'umiliazione del Parlamento. La sua elezione diventa un sottoprodotto, un cascame, un accessorio dell'elezione del Capo del Governo. Avete poi tolto al Parlamento il potere che caratterizza una forma di governo parlamentare, quello basilare che esiste in Spagna e in Germania (i modelli a cui noi ci ispiriamo): il Parlamento deve poter avere, se ha una dignità, la possibilità di sostituire il Presidente del Consiglio. Voi, invece, avete previsto che, se il Presidente del Consiglio viene sfiduciato, il Parlamento muore. Ribadite che il Parlamento può sfiduciare il *Premier*. Ma che potere è quello che, se esercitato, determina la morte di chi lo esercita? È un finto potere, è una presa in giro di potere. Ecco, questa cosa, insieme al declassamento e all'esautoramento della figura del Capo dello Stato, il cui ruolo viene compresso e schiacciato, a cui si impedisce di esercitare le proprie funzioni di garanzia istituzionale, di coordinamento, di motore di riserva nelle emergenze e nelle crisi politiche più gravi, è uno dei dati che maggiormente ci allarma e su cui io penso dovremmo discutere a lungo anche nei prossimi mesi. anche nei prossimi mesi. Infine - e questo è un punto per me fondamentale, perché ho difeso quella riforma quando ho iniziato la mia militanza politica e trovo che questa banalizzazione che se ne fa sia insopportabile continuate a sostenere, nonostante tutta la dottrina dica che è un'assurdità, la replicabilità a livello nazionale della forma di governo dei Comuni e delle Regioni. Fatela finita! Vi rivolgo un appello: fatela finita. È una cosa non seria. Dobbiamo ricordarvi ogni volta che paragonare il Parlamento a un Consiglio comunale o a un Consiglio regionale è un affronto nei confronti del Parlamento. Ma voi in Costituzione trovate scritto il modo in cui vengono eletti i Consigli comunali e i Consigli regionali? I Consigli comunali e i Consigli regionali sono un potere dello Stato? No. *(Applausi)*. Vi domando: Vi domando: l'equivalente del Presidente della Repubblica c'è nei Consigli comunali e regionali? No. Il potere di revisione costituzionale esiste a livello di Consiglio comunale? Un Consiglio comunale cambia al massimo il regolamento della TARI o un piano regolatore, non può cambiare la Costituzione.

sono cose che hanno funzionato bene nei Comuni e nelle Regioni, ma che non possono funzionare a livello nazionale per tutte le ragioni che ho enunciato. Vi mettete su una strada che può portare a degenerazioni molto gravi, a concentrazioni del potere eccessivo e a uno squilibrio che nuocerà alla qualità e alla funzionalità della nostra democrazia. arriviamo oggi a discutere una proposta di riforma costituzionale che ha visto un grande lavoro propositivo avanzato dal nostro Gruppo in Commissione. Diverse sono state le proposte emendative nel merito della riforma e diversi gli interventi che hanno provato a mettere in luce quelle che per noi risultano vere e proprie lacune del progetto presentato dal Governo. Rispetto a questo nostro lavoro, nella parte emendativa abbiamo riscontrato, purtroppo - come è già stato sottolineato da diversi colleghi che mi hanno preceduto - una resistenza da parte della maggioranza verso un confronto serio e costruttivo, unito all'assenza di volontà di discutere nel merito le proposte alternative che abbiamo avanzato. Vi sono stati una sordità e un incomprensibile immobilismo da parte dei parlamentari della stessa maggioranza, quasi a certificare sin d'ora, nei fatti, quali sarebbero gli effetti di una riforma che mira a concentrare la gran parte dei poteri nelle mani di una sola persona, a discapito del Parlamento. Parlamento. Valutando gli elementi di criticità del progetto di riforma in esame, non si può non dire che questa riforma finirà per svilire le prerogative del Capo dello Stato - come è stato detto - oltre a quelle del Parlamento. Proporre di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, quando il Presidente della Repubblica resta un organo figlio di un'elezione secondaria, non fa altro che creare i presupposti per un potenziale scontro di legittimità ogniqualvolta il Presidente della Repubblica, secondo le prerogative previste dalla stessa Costituzione, dovesse provare a far valere il proprio ruolo di garante dell'unità nazionale e la propria figura di terzietà nella rappresentanza delle istituzioni del nostro Paese rispetto a quelli invece, potrebbero essere gli intendimenti del Capo del Governo di turno eletto dal popolo, così come voi vorreste. Inoltre, un'altra stortura di cui si denuncia l'inappropriatezza e di cui la maggioranza è ben consapevole, anche se prova a negarlo in tutti i modi, è quella di proporre un disegno di legge costituzionale per eleggere direttamente il Presidente del Consiglio in contemporanea con il Parlamento, ma rimandando la definizione delle regole di elezione dello stesso Parlamento a una legge elettorale futura di cui non si conoscono assolutamente i contenuti. Addirittura, avevate provato a stabilire direttamente nel testo della Costituzione un premio di maggioranza del 55 per cento che, per fortuna, solo dietro la spinta dell'opposizione è stato poi cancellato e rimandato per la sua definizione sempre a un'inconoscibile futura legge elettorale. Su questa materia siamo a chiedere, ancora oggi, un approfondimento degli intendimenti della maggioranza e del Governo, ma suppongo - spero di sbagliarmi - che quei chiarimenti non arriveranno. non arriveranno. Tutto ciò ci porta a pensare che questo modo di procedere sia una scelta voluta per rispondere alla logica di scambio tra i maggiori partiti della maggioranza, maggioranza, che finirà per dividere l'Italia - da un lato - con l'autonomia differenziata, arrecando un *vulnus* alla democrazia parlamentare e - dall'altro - con il progetto di legge sul premierato che prevede, a cascata, un effetto diretto sul Parlamento. L'elezione diretta del *Premier* indebolisce il Parlamento e marginalizza il Presidente della Repubblica. Il collega Parrini ha detto prima che il premierato non esiste in alcun altro Paese del mondo. Perché? Non perché questo Governo si pensa più furbo degli altri, ma perché distrugge l'equilibrio tra i poteri dello Stato e rappresenta un danno per i cittadini. La logica sottesa è quella della verticalizzazione e della democrazia del capo al posto della democrazia della partecipazione e della rappresentanza; una vera regressione da contrastare, immagino, dando vita a una coalizione sociale e culturale per attuare i principi costituzionali. Un'attenzione agli equilibri tra le attuali forze politiche di maggioranza del tutto estranea alla dimensione costituzionale dovrebbe porsi a fondamento di una proposta di riforma. È questo il difetto maggiore di tutto il dibattito sul premierato. Insomma, c'è da chiedersi se le riforme costituzionali si fanno per seguire le manie di una parte politica o per risolvere i problemi di fondo della democrazia italiana. È evidente che c'è una retorica, quella che avete attuato e state attuando ormai da tempo, attraverso i *mass media*, attraverso il dibattito in Commissione e attraverso le discussioni pubbliche, che prova a tranquillizzare: quella in base alla quale, in fondo, questa riforma tocca soltanto quattro articoli della Carta. Non si modificano - provate a dire - i poteri del Capo dello Stato, né si riducono quelli del Parlamento. La verità è completamente diversa: non solo si squilibrano tutti i poteri, ma si nasconde la vera posta in gioco, che è il tentativo di passare dalla democrazia pluralista a una democrazia del capo. Questo è il discrimine che rende sostanzialmente inaccettabile il disegno di legge sul premierato, nonostante i tentativi di ridurne la portata. È l'elezione di un capo che porta a sbilanciare radicalmente il già precario equilibrio del nostro sistema democratico. Una revisione consapevole della Costituzione avrebbe dovuto innanzitutto rafforzare il Parlamento e indirettamente ristabilire i giusti rapporti con gli altri poteri dello Stato, tanto il Capo dello Stato quanto il Governo. Però, quando abbiamo discusso in Commissione di questa riforma, in molti la abbiamo legata a un'altra riforma, o un altro disegno di legge che questo ramo del Parlamento ha già approvato e che adesso è in discussione alla Camera. Mi riferisco alla riforma del premierato e alla riforma dell'autonomia differenziata. Qual è il nesso tra queste due vostre proposte? Il premierato e l'autonomia differenziata sono uno scambio politico all'interno della maggioranza. La coerenza è, ancora una volta, puramente politica, anzi partitica, priva di una dimensione propriamente costituzionale. Il programma di Governo, infatti, prevede il premierato per Fratelli d'Italia e l'autonomia differenziata per la Lega: insomma, una Costituzione fatta a fette tra le forze di maggioranza. Altro che Costituzione di tutti! A proposito di coerenza, si può però indicare un elemento che unisce tutte le forze di destra che compongono questo Governo, e cioè l'idea di verticalizzazione dei poteri. Effettivamente, pensandoci, tanto con l'autonomia differenziata quanto con il premierato si afferma la democrazia del capo, in ambito regionale a favore dei Presidenti di Regione dandogli ulteriori poteri, nel secondo caso a favore del Presidente del Consiglio. Ma d'altro canto la destra ha sempre sognato un modello di maggiore concentrazione di potere in mano al capo. Su tutto questo, noi saremo qui, pronti a fare tutto ciò che è nel nostro potere, finché ciò ci sarà concesso, per contrastare questo modo di procedere che svilisce il ruolo dell'attuale Parlamento e che disarticola quella istituzione, quegli istituti che fortunatamente la nostra Costituzione già oggi prevede a tutela e a salvaguardia della coesione territoriale, del pluralismo e della rappresentanza, riportando questi valori a un rapporto e a un livello più alto. Mi riferisco al riconoscimento vero e non solo formale del ruolo all'interno dell'ordinamento della Repubblica e che passa anche per il tramite delle azioni che siamo in grado di mettere in campo già oggi. Per tutte queste ragioni, l'opposizione del Partito Democratico al premierato è e sarà netta, forte e motivata nel Parlamento, ma soprattutto nel Paese.

come e perché questa sia non una riforma, ma un rifacimento dalle fondamenta del sistema di governo che scardina i meccanismi della divisione e del bilanciamento dei poteri dello Stato. Alcuni senatori hanno anche lanciato un appello al senso di responsabilità della maggioranza per addivenire a soluzioni meno traumatiche e divisive; un appello che è destinato a cadere nel vuoto, perché ci troviamo dinanzi non a un omicidio preterintenzionale della Costituzione antifascista del 1948, dovuto a imperizia e inadeguatezza degli ingegneri di questa riforma, riforma, ma a un omicidio premeditato e a lungo pianificato. Ci troviamo dinanzi a un disegno di liquidazione di questa Costituzione da parte di forze politiche che l'hanno sempre vissuta come fumo negli occhi, che mai si sono identificate nei suoi valori e che oggi non vogliono perdere l'occasione storica di liberarsene una volta per tutte, approfittando dei rapporti di forza contingenti. Perché questa prospettazione non sembri un indebito processo alle intenzioni, mi limito a rievocare e a lasciare a verbale del Senato alcuni dati storici inequivocabili. Fratelli d'Italia, la forza politica che di questa riforma ha fatto una bandiera, è l'erede del Movimento Sociale Italiano, che nell'immediato Dopoguerra divenne il veicolo politico del riciclaggio, nel nuovo ordine repubblicano, di quella parte del Paese che era rimasta fedele ai valori del fascismo. Il Movimento Sociale Italiano - come attestato da sentenze definitive ha giocato a lungo di sponda con varie formazioni neofasciste estremiste, come ad esempio Ordine Nuovo, protagonista della sanguinosa strategia della tensione, tramite uomini cerniera come Pino Rauti ed altri che occupavano ruoli di rilievo nel partito. L'avversione alla nuova Costituzione fu da subito apertamente dichiarata da coloro che, il 26 dicembre 1946, fondarono il Movimento Sociale Italiano. In particolare uno di essi, tra i più autorevoli, il giurista Carlo Costamagna, già docente di diritto corporativo all'Università di Pisa, nel denigrare il lavoro dei Costituenti, dichiarò che mai avrebbero accettato una Costituzione imposta dai vincitori della guerra e sin da allora impegnò il partito per l'instaurazione di una Repubblica presidenziale "intesa come alternativa allo Stato dei partiti, piegato alle istanze dei sindacati e del mondo dei lavoratori". Nel 1954 Pino Rauti, al congresso del Movimento Sociale a Viareggio, dichiarava testualmente che la democrazia è un'infezione dello spirito. Nel 1971 il Movimento Sociale Italiano raccoglieva le firme per l'elezione diretta del Capo dello Stato con una legge che concentrava il potere in un unico vertice e limitava gli spazi di mediazione. Il progetto viene sposato dai vertici della P2, cabina di regia politica di eversione della democrazia, che raccoglieva le componenti più reazionarie del Paese. Attraverso la sponsorizzazione della P2, l'aspirazione alla restaurazione, in forme moderne, del vecchio ordine piramidale e autoritario fascista viene veicolato anche in altre formazioni politiche, attraversando varie legislature. Il progetto, rilanciato da ultimo da Giorgia Meloni nella XVIII legislatura, che ne rivendica la primogenitura, oggi arriva finalmente in porto nel travestimento della forma del premierato. Bisogna dare atto di una coerenza straordinaria, che dal 1946 ha sfidato il tempo; coerenza attestata anche dalla perdurante e dichiarata fedeltà del presidente del Consiglio Meloni agli ideali di Pino Rauti e dalla celebrazione qui in Senato nel 2022, da parte di esponenti autorevoli di Fratelli d'Italia, di personaggi come il generale Maletti, già vertice dei Servizi segreti, condannato con sentenza definitiva per favoreggiamento di soggetti coinvolti nella strage neofascista alla Banca dell'agricoltura di Milano nel 1969, eseguita da esponenti di Ordine Nuovo proprio per creare uno stato di emergenza propizio all'instaurazione di una Repubblica presidenziale, come accertato con sentenza definitiva. Quanto a Forza Italia, basti ricordare che Berlusconi, fondatore del partito, era componente della P2; egli definì la Costituzione del 1948 come "vecchia e comunista" e apostrofò la Corte costituzionale come "covo di comunisti". Infine, quanto alla mancata identificazione della Lega nei valori della Costituzione, basti ricordare che il suo *leader* ha candidato alle elezioni europee, indicandolo come uomo simbolo dei valori del partito, un generale che manifesta apertamente la propria ammirazione nei confronti del fondatore del fascismo e plateale disprezzo per i più elementari valori della convivenza democratica. Detta premessa dimostra come sarebbe errato considerare questa come una partita legata solo all'attuale contingenza politica. C'è una densità del problema che può essere colta soltanto uscendo da visioni astratte e destoricizzate. In realtà, siamo dinanzi a un bivio della storia. È come se si fosse giunti, in questo tornante della storia, alla fine dei giochi di una partita che non si è mai chiusa, che è sempre rimasta aperta, tra due Italie che non riescono tutt'oggi a riconoscersi in una stessa Costituzione come casa comune, come quadro condiviso di valori fondanti del patto sociale di convivenza. Dopo che la presidente del Consiglio Meloni, in un empito entusiastico, aveva definito questa come la madre di tutte le riforme, cioè come la chiamata alle armi per una rivincita nei confronti di una Costituzione mai condivisa, si è deciso di cambiare strategia, quando si è compreso che c'è il pericolo di perdere il *referendum* se gli italiani dovessero vivere la sfida referendaria come una scelta tra la Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gode di un consenso popolare impareggiabile e il cui ruolo in in questa riforma viene svuotato. Si tenta ora di buttare acqua sul fuoco, di negare e minimizzare dirompenti e calcolati effetti a cascata di questa riforma che concentra il potere dello Stato nelle mani di un *Premier*, che sembra l'edizione italiana dei caudilli sudamericani; che annichilisce e lobotomizza il Parlamento; che svuota il ruolo del Presidente della Repubblica; che rende a portata di mano la conquista da parte di minoranze del Paese di tutte le postazioni strategiche dallo Stato, dalla Presidenza della Repubblica alla Corte costituzionale fino al Consiglio superiore della magistratura. Ho detto "la conquista da parte di minoranze" non per un *lapsus*, ma con cognizione di causa, come spiegherò tra poco. La leva strategica per raggiungere tale risultato è la costituzionalizzazione del principio maggioritario, prevista all'articolo 92 del progetto di riforma, senza indicare le condizioni di operatività dal premio di maggioranza. Viene taciuto se sarà prevista o meno una soglia minima per ottenere il premio di maggioranza, se sarà previsto o meno un ballottaggio e quale sarà la percentuale di tale premio di maggioranza. Si tratta di una manovra callida e sleale: si tiene coperta la carta strategica di una legge elettorale, da giocare in modo vincente in un secondo tempo, lasciandosi le mani libere per costruirla in modo sartoriale sulle esigenze delle attuali forze di maggioranza; mani libere per raggiungere lo scopo di illudere la pubblica opinione che sarà la maggioranza della Nazione a eleggere il *Premier* e a legittimare dunque la somma dei superpoteri che gli sono attribuiti. Ma in realtà, grazie ai maneggi del principio maggioritario e di una legge elettorale studiata a tavolino, sarà possibile l'elezione da parte di minoranze travestite da maggioranza del Paese. Mi limito a un esempio concreto ed esplicativo: nelle elezioni politiche nazionali del 2022, il corpo elettorale era costituito da 51,5 milioni di cittadini aventi diritto al voto. L'intera coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni ha raccolto 12,3 milioni di voti, pari al 26,7 per cento del corpo elettorale. Poiché la percentuale di voti si calcola non sul numero dei cittadini aventi diritto al voto, ma sui votanti effettivi, escludendo gli astenuti e quelli che hanno votato scheda bianca, la percentuale lievita dal 26,7 per cento al 43,8. Grazie al premio di maggioranza, la

Ecco come una minoranza può trasformarsi in maggioranza della Nazione che consacra e legittima i superpoteri attribuiti a un *Premier* caudillo. Concludo, Presidente. I rospi che si trasformano in principi, però, esistono solo nelle favole; nella realtà esistono invece minoranze organizzate che, grazie a questa riforma, potranno imporre la loro dittatura alle maggioranze del Paese; maggioranze private di tutti gli spazi di mediazione democratica e di tutte le garanzie contro gli abusi di un *Premier* elevato a capo assoluto e abilitato a fare strame dei diritti delle maggioranze e dei cittadini, esattamente come avvenne negli anni Venti in Italia, con l'avvento del regime fascista; un regime che non dobbiamo dimenticare, che conquistò il potere non solo con la violenza, ma anche grazie a un'abile e cinica manipolazione delle illusioni e dell'ingenuità delle masse. Oggi la democrazia è esposta agli stessi pericoli degli anni Venti: la sfida è dunque totale. Il MoVimento 5 Stelle rappresenta l'Italia che si identifica pienamente nei valori della Costituzione e si batterà con tutte le sue forze perché i nemici della Costituzione, i nemici della democrazia vengano ancora una volta sconfitti.

Signora Presidente, non intendo soffermarmi più di tanto sulle ragioni di merito per le quali noi siamo contrari a questo provvedimento, perché molti senatori di opposizione, con grande qualità degli interventi, hanno sottolineato nei lavori di Commissione e in quelli in Aula le profonde ragioni di dissenso e di contrasto. Da ultimo, la senatrice a vita Liliana Segre ieri ha svolto un intervento di grande spessore morale e intellettuale, che tutti dovrebbero ascoltare e soprattutto sul sul quale i senatori di maggioranza dovrebbero riflettere, perché non è un intervento dell'opposizione: è un intervento di una persona che ha a cuore le istituzioni democratiche del nostro Paese. È stato detto - e stamattina anche ripetuto dai pochi interventi della maggioranza - che non viene toccato il ruolo del Presidente della Repubblica. Questa è francamente un'affermazione ridicola che dovrebbe essere accantonata, perché il potere del Presidente della Repubblica viene modificato profondamente nella sua sua possibilità di sciogliere le Camere, che viene utilizzata nella prassi - come abbiamo visto anche in questi ultimi anni - come modalità per non sciogliere le Camere e, quindi, per aiutare le possibili maggioranze parlamentari nella nascita dei Governi,

con queste norme c'è uno svuotamento totale dei poteri del Parlamento e mi stupisce che i senatori votino così allegramente il loro suicidio. Nel momento in cui il Governo e il Presidente del Consiglio eletto possono portare automaticamente allo scioglimento delle Camere, è evidente che questo non è che debba avvenire, ma sarà minacciato ogni giorno. Nella concreta vita parlamentare il Presidente del Consiglio, di fronte a ogni contrasto, a ogni dissenso col Parlamento o con la propria maggioranza, minaccerà le dimissioni e quindi lo scioglimento delle Camere. Si avrà, quindi, un Parlamento tenuto sotto ricatto totale. Devo dire che dietro questa scelta, anche se negata da parole tranquillizzanti, c'è una specie di riflesso autoritario di parte della maggioranza. Vi ricordate il dottor Stranamore, a cui partiva improvvisamente il braccio e non riusciva a controllare? Mi pare che ci sia questo riflesso autoritario che scatta involontariamente, altrimenti non si può spiegare perché avete imboccato siffatta strada. Per farlo violate alcune regole di buonsenso che derivano anche dall'esperienza degli ultimi anni, che dovrebbe essere di insegnamento. La prima regola è che il cambio della Costituzione si fa solo con un'intesa tra le forze parlamentari. L'articolo 138 spinge alla modifica in questo senso: si deve cercare un'intesa tra maggioranza e opposizione; poi, naturalmente, come in tutte le norme, c'è una disposizione di chiusura,

A questo si aggiunge un'altra considerazione: si avrà il massimo dell'instabilità, e non della stabilità. Che Paese sarà quello in cui una maggioranza parlamentare, utilizzando i numeri che ha in quel momento, modifica le regole del gioco? Proviamo a immaginare se ogni maggioranza arrivata a governare il Paese modificasse le regole del gioco costituzionali e della legge elettorale approvate dalla maggioranza precedente: saremmo condannati a una perenne instabilità. Altro che stabilità! Del resto questo è successo:

che dev'essere presentata all'intesa parlamentare, non portata avanti in questo modo, con queste forzature. L'intesa non l'avete nemmeno cercata in tutto il dibattito nella Commissione e la disattenzione con cui questo dibattito avviene in Aula è la prova che comunque avete deciso di andare avanti. *(Applausi)*. State ad ascoltare le ragioni delle opposizioni solo perché dovete farlo, perché non potete farne meno.

fate questa riforma per un calcolo di presunta convenienza e state costruendo un *boomerang* che vi tornerà indietro, perché con questa riforma vi state facendo del male da soli. Questa riforma non vi conviene per alcuni motivi molto pratici.

solo. Pensiamo a quello che è successo negli ultimi anni, a cominciare dalla legge del 1953, quella che io mi rifiuto di chiamare legge truffa, che prevedeva un piccolissimo premio di maggioranza per governare meglio il Paese, che è stata fermata dal voto degli italiani.

di convincervi, perché qui la capacità di ravvedimento è molto scarsa e si va avanti distrattamente, ma vorrei delineare questo scenario:

se il sistema entrasse in vigore, con l'elezione diretta del *Premier*, l'opposizione potrà scegliere in quel momento il candidato *Premier* migliore per andare a vincere, la personalità migliore, voi dovrete candidare la presidente Meloni e non avrete alcun margine di libertà sulla scelta del momento ed è facile immaginare che a fine legislatura non ci sarà il picco di consensi che c'è oggi, dopo cinque anni, anche per le ragioni che ho detto prima. Perciò, vi state costruendo da soli una gabbia - lo dico in particolare a Forza Italia e alla Lega - e state finendo di vivere la coalizione come scelta. alla scelta di stare nella coalizione e del candidato migliore e state costruendo una gabbia che vi costringerà, qualsiasi siano le condizioni di consenso in quel momento, a candidare la Meloni.

in Parlamento e nel Paese. Stiamo cercando di farlo e cercheremo di farlo, ma le difficoltà si vedono costantemente: voi ci aprite un'autostrada, perché nel momento in cui andremo all'elezione diretta del *Premier*, non ci sarà più spazio per terze candidature e terzi poli, ma il sistema porterà a uno scontro tra due persone e tra due schieramenti, state creando il collante migliore per farci superare tutte le difficoltà di costruire un campo delle opposizioni aggregato. Dovremmo quindi, in qualche modo, ringraziarvi. State festosamente e allegramente compiendo un atto di autolesionismo politico e lo dico affettuosamente al senatore Balboni, perché siamo concittadini e siamo stati anche nelle stesse scuole negli anni della giovinezza: mi dispiace che leghi il suo nome a un atto di autolesionismo politico,

Nonostante questo, noi restiamo contrari, perché sappiamo che, al di là delle logiche di convenienza, questa riforma parlamentare reca un danno enorme al sistema democratico del Paese. Siamo quindi contrari e resteremo in ogni occasione in campo per ostacolare questa approvazione.

illustri colleghi, mi concederete un minimo di autonomia e di libertà di giudizio rispetto alle stesse parti che in quest'Aula hanno rappresentato le loro ragioni, se non altro per la lunga esperienza che ho maturato in questo Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, per oltre quarant'anni. Ho sempre cercato di servire le istituzioni senza integralismi, ma con la convinzione che qui dentro nessuno abbia il monopolio della verità. La riforma della seconda parte della Costituzione è stata più volte proposta, negli ultimi decenni, da tutte le forze politiche che si sono succedute nel Governo del Paese, allo scopo di adeguare il sistema istituzionale ai cambiamenti della società e dell'economia, nonché all'evoluzione del sistema politico. Tutti i tentativi di riforma sono falliti, non tanto per le soluzioni prospettate, quanto perché non si è cercata una forte condivisione, come diceva il collega e amico Franceschini, sia nel metodo sia nel merito delle scelte operate. Le riforme costituzionali hanno possibilità di successo quando sono frutto di scelte ponderate e condivise. Più ampia è la convergenza tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, più solida e robusta è la costruzione che ne risulta. Più coesa è la costruzione, più forte, dunque, l'impianto. Ciò dimostra la Costituzione vigente, elaborata da forze allora ideologicamente contrapposte, al culmine della guerra fredda, ma capaci di uno sforzo comune in nome dell'Italia e della sua coesione nazionale. i *referendum* confermativi di riforme approvate a maggioranza e all'esito di dinamiche politiche conflittuali hanno sempre avuto esito negativo, proprio perché quelle riforme sono state recepite dai cittadini come proposte fortemente divisive. Sul piano politico, inoltre, in quei casi si è verificato l'effetto di compattare le opposizioni contro il Governo e di spingere gli elettori a esprimere un voto più sui *leader* e sulle forze politiche in campo che non sul merito del progetto costituzionale. La politica costituzionale è, per sua natura, lo spazio della condivisione, nella misura in cui è chiamata ad assolvere a una funzione unificante e stabilizzante dell'intero sistema democratico, fissando regole in cui una comunità possa riconoscersi e attraverso le quali possa prosperare. Non a caso il costituente, nei processi di revisione, ha previsto maggioranze qualificate. Anche con riguardo alla riforma oggi all'esame del Parlamento, nonostante il dibattito in Commissione affari costituzionali sia stato lungo in termini temporali, constato che non ci sono stati una reale ricerca di condivisione né un ascolto delle soluzioni avanzate dalle opposizioni. Peraltro, è mancata finora un'attenta ponderazione delle criticità espresse anche dai costituzionalisti, i più illustri, nel dibattito pubblico. D'altro canto, in questo caso parlo all'opposizione, le opposizioni non possono utilizzare la materia costituzionale a fini ostruzionistici, né possono essere aprioristicamente oppositive rispetto alla scelta legittima della maggioranza di operare cambiamenti. Sul piano del merito, è assolutamente legittima la finalità perseguita con questo progetto di riforma, volto *in primis* a contrastare l'instabilità dei Governi e a rafforzare il ruolo e la posizione costituzionale del Presidente del Consiglio. Per certi versi, ricordo molti predecessori della Meloni, da Romano Prodi a Silvio Berlusconi, certamente di orientamenti opposti e sempre tra loro antagonisti, che si lamentarono dell'insufficienza dei poteri di indirizzo da parte di chi serve le Istituzioni a Palazzo Chigi. Questo è però un altro problema. Non condivido dunque gli orientamenti critici che intravedono sempre, in qualsiasi riforma volta al rafforzamento dell'Esecutivo, una torsione decisionista e autoritaria, lesiva dei fondamenti del nostro ordinamento democratico. Il panorama costituzionale comparato ci restituisce invece un quadro articolato di forme di governo presidenziali e semipresidenziali proprio in Paesi di lunga e riconosciuta tradizione democratica. In quei modelli però, colleghi, a fronte di un forte ruolo di vertice del potere esecutivo, che trova il suo fondamento nell'elezione a suffragio universale diretto, sono presenti adeguati contrappesi con funzioni di bilanciamento e di controllo. Facciamo l'esempio tipico: negli Stati Uniti d'America, il Congresso e il Senato hanno poteri molto intensi di iniziativa legislativa e di inchiesta e condizionano l'azione dei Governi. Non a caso si parla di anatra zoppa, quando il Presidente degli Stati Uniti d'America perde le elezioni di *midterm* e non a caso i Presidenti degli Stati Uniti d'America mantengono un dialogo permanente con il Senato e con la Camera e sono costretti a mediazioni estenuanti con l'ultimo dei parlamentari eletto nell'ultimo degli Stati americani. Al contrario, nella proposta attualmente all'esame del Parlamento il rafforzamento della posizione del *Premier* si accompagna al depotenziamento finale degli istituti di garanzia. Si è in presenza di una contraddizione di fondo: da una parte, si afferma di voler mantenere la forma di governo parlamentare scelta dai costituenti; dall'altra, se ne indeboliscono gli elementi fondamentali, quali il ruolo del Parlamento, con particolare riguardo al circuito fiduciario, e le prerogative del Capo dello Stato. L'elezione popolare diretta del *Premier* impatta infatti sull'equilibrio tra la funzione di indirizzo politico, affidata alla maggioranza ed esercitata attraverso il raccordo con corpo elettorale, Parlamento e Governo, e la funzione di controllo costituzionale, affidata ad organi neutri e imparziali, quale il Presidente della Repubblica. Soffermiamoci un attimo sul Presidente della Repubblica. Nella riforma, nonostante le affermazioni dei proponenti, i poteri del Capo dello Stato nella formazione dei Governi e nello scioglimento delle Camere si trasformano di fatto da liberi in vincolati diventano atti dovuti, non più discrezionali atti di impulso. Limitare in modo così significativo le prerogative del Presidente della Repubblica nella gestione delle crisi di Governo, sempre possibili anche in presenza di un *Premier* eletto direttamente dal popolo, per effetto della rottura dell'accordo di coalizione, significa impedire il necessario grado di flessibilità al sistema, che è, questo sì, garanzia di tenuta democratica, come dimostra la storia repubblicana. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri in carica e di sfiducia allo stesso, lo spazio di manovra del Capo dello Stato è limitatissimo; potrebbe conferire infatti l'incarico di formare il Governo solo a un altro parlamentare di maggioranza che oltretutto, rispetto alle affermazioni pubblicitarie su questa riforma costituzionale, sarebbe lì in sfregio alla sacrosanta indicazione *(Applausi)* che voi proclamate che i cittadini devono indirizzare la scelta del Presidente del Consiglio. La *moral suasion* del Presidente può essere formalmente intatta, ma viene depotenziata, circoscritta all'interno dello stesso perimetro nel quale si confinano le sue prerogative. Il Presidente della Repubblica ha un'autorevolezza menomata, a fronte di un vertice dell'Esecutivo che trova la sua legittimazione diretta nell'elezione diretta

dunque, è di perdere una risorsa straordinaria del nostro ordinamento. L'evoluzione del ruolo del Capo dello Stato ci ha consegnato una figura che non è solo quella di un notaio passivo ma, come ricorda la Corte costituzionale nella sentenza del 2013, è capace di ristabilire il funzionamento del sistema nei momenti di blocco e di crisi. Peraltro, colleghi, guardiamo un po' l'esperienza concreta: abbiamo avuto due Presidenti della Repubblica - Napolitano e Mattarella - eletti da maggioranze diverse e che, nel voto successivo di conferma, hanno allargato ai partiti che non li avevano scelti nella prima fase la condivisione, perché sono stati votati quasi unanimemente. Pertanto, l'esperienza concreta ci dice che questa flessibilità, questa possibilità di esercitare la *moral suasion* e questo ruolo del Presidente della Repubblica sono riconosciuti anche da chi in una prima fase poteva averne avversato o non scelto l'indicazione. È il meccanismo che funziona; è una delle poche cose - ve lo dico sinceramente - che in questo Paese funzionano e che noi andiamo a modificare in base a princìpi, a mio parere, sbagliati. il tema che più dovrebbe interessarci in quest'Aula è un altro e secondo me è poco evidenziato: questa riforma indebolisce il ruolo del Parlamento, soprattutto nel suo rapporto con il Governo. Il Parlamento perde infatti la funzione sostanziale di investitura del Governo e l'istituto di fiducia è un elemento cardine. In questi In questi quarant'anni - vi dico la mia esperienza - il Parlamento ha subito un processo progressivo di lateralizzazione, ma l'unica cosa che ancora resiste come potere del Parlamento è il mandato fiduciario che noi, come parlamentari, esprimiamo nei confronti del Governo. *(Applausi)*. Quando il mandato fiduciario, che è l'ultima cosa che ci rimane per esercitare una qualche influenza, viene espropriato perché trasferito direttamente agli elettori, noi che cosa facciamo? Certo, la democrazia... *(Commenti).* Vedo qualche collega che interloquisce e mi fa anche piacere. È ovvio che è sempre democratico, perché sono gli elettori che scelgono il Presidente del Consiglio, ma noi come ruolo siamo completamente depotenziati. Il ruolo del Parlamento è la vera vittima in questa riforma, prima di qualsiasi altro potere. Dunque finiremo per fare i passacarte; si continuerà ad incrementare questo processo in base al quale il Parlamento è espropriato e magari - scusatemi la battuta polemica che faccio anche verso le opposizioni - continueremo a istituire Commissioni d'inchiesta sui vari argomenti per provare per provare a fare qualcosa. Anche questa è un'altra patologia del sistema: andiamo a trovare - per così dire - spazi di azione che dovrebbero essere consegnati all'eccezionalità e che diventano quasi la normalità. Sto terminando, signor Presidente, ma vorrei anche dire che la stessa scelta che noi abbiamo fatto, a cui io mi sono opposto purtroppo solitariamente, della riduzione del numero dei parlamentari, che per molti era la panacea di una riforma del sistema, ha avuto ha avuto l'effetto di far perdere credibilità e slancio all'istituzione rappresentativa, cioè al Parlamento; ha acuito il *deficit* di rappresentanza dell'istituzione parlamentare e, al contempo, ha determinato inefficienza nel funzionamento dell'attività legislativa, soprattutto al Senato. Dunque colleghi, se questo è il contesto, vorrei dire che la scelta di inserire in Costituzione il premio di maggioranza senza prevedere contestualmente una soglia minima e ragionevole di voti ottenuti è un altro grave *vulnus*. Anche i Costituenti si erano posti il problema di disciplinare o comunque di dare indicazioni in Costituzione sul sistema elettorale, ma hanno scelto di non introdurre ulteriori elementi di rigidità, lasciando invece alla discrezionalità del legislatore ordinario la scelta del sistema più adeguato all'evoluzione delle dinamiche politiche e sociali. La Corte costituzionale, come sapete, ha affermato che l'assenza di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza rappresenta una violazione dei princìpi costituzionali. Qui però non c'è solo il principio costituzionale, ma c'è soprattutto il buonsenso. In conclusione, il nostro sistema necessita di interventi di razionalizzazione e che essi debbano essere rivolti anche a rafforzare la posizione del *Premier* all'interno del Governo nei confronti di altri organi costituzionali è una cosa su cui si può seriamente ragionare. Tuttavia, se si sceglie di rimanere nell'alveo delle forme di governo parlamentare e non virare con decisione verso forme di governo autenticamente presidenziale, corredate dagli istituti necessari di *check and balance*, non si può fare attraverso una Costituzione ibrida, che si limiti all'elezione diretta del *Premier* e alle concentrazioni di prerogative nelle sue mani; occorre contestualmente intervenire per rafforzare il ruolo del Parlamento. Non c'è traccia nella riforma di interventi volti a limitare la decretazione d'urgenza, rafforzare l'iniziativa legislativa parlamentare, restituire spazio all'istruttoria legislativa in Commissione, accrescere i poteri ispettivi e di controllo del Parlamento sull'attività di Governo. In conclusione, esprimo una speranza, una speranza, perché in tutte le cose c'è sempre una luce. La speranza è che questo dibattito, peraltro desolatamente privo della tensione ideale che ha animato le grandi scelte costituzionali del passato, sia solo un'esibizione muscolare pre-elettorale e, da qui a poco, la saggezza, pure presente anche in parti della maggioranza, sappia imporre una svolta a un dibattito su una riforma nata male e che rischia di finire peggio; una riforma non all'altezza delle risposte che l'Italia chiede e con l'umiliazione finale e definitiva del Parlamento.

Ministra, crediamo che questa riforma, voluta dal suo Governo, sia non solo profondamente sbagliata, dannosa e finanche pericolosa per il nostro Paese e per la nostra democrazia. Lo dico anche in questa sede, ma è ben noto: noi dell'Alleanza Verdi-Sinistra abbiamo presentato anche in quest'Aula oltre mille emendamenti, alcuni dei quali sono di merito e cercano di disegnare un'altra idea di assetto istituzionale, assai diversa da quella contenuta nella vostra ipotesi; molti altri, sono ostruzionistici. Lo dico e lo rivendico senza nessun imbarazzo, perché credo che, dinanzi a un tentativo così clamoroso di stravolgere la nostra Costituzione (perché di questo si tratta, non certo di un intervento chirurgico), tutti gli strumenti previsti dalle regole sono giusti: oggi l'ostruzionismo in Parlamento, domani i comitati per il no al *referendum* confermativo, che contribuiremo a costruire e ad animare. Com'è stato autorevolmente ricordato ieri dalla senatrice Segre nel suo importante intervento, di grande spessore, negli anni recenti, per ben due volte, nel 2006 e nel 2016, gli italiani hanno bocciato nelle urne due proposte di riforma che ritenevano sbagliate; io credo che anche questa volta si dimostreranno assai più saggi di chi li governa. *(Applausi)*. Perché è così sbagliata e così pericolosa questa vostra proposta di riforma? Io credo per due ragioni fondamentali. La prima è perché interviene, scardinandolo, su un punto decisivo su cui sono fondate le democrazie, cioè l'equilibrio dei poteri. un principio cardine, sancito in tutte le Costituzioni europee approvate dopo la tragedia delle guerre e delle dittature. Questa vostra riforma legittima il dominio dell'Esecutivo sul potere legislativo, con un'ulteriore espansione dei poteri del Governo: una scorciatoia demagogica che accentuerà la crisi democratica in atto, andando a minare anche l'equilibrio tra la funzione di indirizzo politico e quella del controllo costituzionale, affidata, come sappiamo, ad organi imparziali ed espressione dell'unità nazionale, come sono il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale (ma ci tornerò diffusamente). La seconda ragione, che affronto invece rapidamente, sta nel combinato disposto con l'altro provvedimento al centro dell'agenda di Governo, quello sull'autonomia differenziata, adesso in discussione alla Camera. Noi abbiamo denunciato più volte la pericolosità e la gravità di questo vero e proprio scambio. E non basta dire, signora Ministra, che questi due punti sono entrambi contenuti nel programma di Governo. Qui non si contesta il fatto che due forze politiche che compongono la stessa maggioranza possano dar vita a una sintesi programmatica. Si contesta, invece, che premierato e autonomia differenziata sembrano ispirati da due logiche diametralmente opposte, che si tengono insieme soltanto per un patto di potere (uno accentra i poteri nelle mani di una sola persona, mentre l'altro decentra tutto, spaccando drammaticamente il nostro Paese), ma che, a ben vedere, hanno un tratto in comune, cioè la marginalizzazione del Parlamento e, più in generale, della democrazia rappresentativa, la sola capace di garantire quel pluralismo su cui si fondano i sistemi istituzionali contemporanei. *(Applausi)*. Sì, perché è proprio l'estromissione del Parlamento dai poteri decisionali uno dei tratti più evidenti non solo dell'autonomia differenziata, ma anche di questa vostra riforma costituzionale. È per questo motivo che noi parliamo di una reale messa in discussione dell'equilibrio fra i poteri. Come è stato ricordato da tanti, che non ha eguali al mondo e che è stato sperimentato, con esito fallimentare, in un solo Paese soltanto per pochi anni. È un sistema nel quale, nella traduzione italiana, si concentrano nelle mani di una sola persona tutti i poteri: si elegge un Parlamento ubbidiente per trascinamento, senza più neanche la minima legittimazione popolare, e si depotenzia una figura, come quella del Capo dello Stato, che pure nella fragile democrazia italiana ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento largamente riconosciuto dai cittadini. È davvero singolare sostenere che questa riforma non toccherebbe le prerogative del Presidente della Repubblica, quando invece muterebbero in radice in senso restrittivo i suoi poteri, in particolare relativamente al procedimento di formazione di un Governo e allo scioglimento delle Camere, tanto per cominciare perché, come appare evidente, al di là di tutte le sgrammaticature che pure ci sono, il Capo dello Stato non potrà respingere la proposta di scioglimento del Parlamento fatta da un Presidente del Consiglio dimissionario, anche se, come sappiamo, a rigor di logica, a una proposta potrebbe sempre corrispondere una risposta negativa, ma evidentemente solo astrattamente. Ministra, avete presentato questa riforma come una mediazione, esattamente, tra chi? Tra di voi, forse, ma non certo con l'intero Parlamento, vista la contrarietà praticamente di tutti i Gruppi dell'opposizione, oltreché dei tanti costituzionalisti che abbiamo avuto modo di ascoltare durante le audizioni. Se possibile, signora Ministra, avete avanzato una proposta ancora peggiore del presidenzialismo da cui siete partiti. Noi - glielo dico con grande nettezza - ci saremmo opposti con forza anche a quel modello, anche al presidenzialismo, perché crediamo che oggi sia proprio l'elezione diretta del capo a essere in contrasto con un pieno sviluppo dei processi democratici, perché essa accentua, a nostro avviso, i tratti di crisi sistemica della fase storica che stiamo attraversando. Consideriamo però questa vostra proposta sul premierato ancora meno rispettosa di quel delicato meccanismo di pesi e contrappesi che è invece essenziale per garantire un sistema che funziona. Si sarebbe dovuti partire da questo, se proprio si voleva proporre una modifica della forma di governo:

che l'elezione diretta non serve certamente a mitigare. Proviamo a guardare alla situazione del nostro Paese e a farlo nella maniera meno ideologica possibile, limitandoci davvero semplicemente a fotografare la realtà. Quasi la metà della popolazione ormai non va nemmeno più a votare. È un astensionismo dilagante, che cresce sempre di più e che assume caratteristiche sempre più di classe (utilizzo non a caso questa parola). Andate a vedere dov'è concentrata la minore partecipazione al voto e scoprirete che corrisponde ai territori dov'è più acuta la sofferenza sociale e dove c'è maggiore povertà, maggiore emarginazione; è una società, la nostra, sempre più destrutturata, nella quale decine di milioni di persone non si sentono più rappresentate da nessuno, privata del tutto di quei corpi intermedi attorno ai quali si era formata la Repubblica, con i partiti spesso ridotti a formazioni personali o a comitati elettorali presenti soltanto in prossimità del voto e senza più quelle strutture - le casematte, le avremmo chiamate un tempo attraverso le quali e dentro le quali immaginare e costruire percorsi formativi e di emancipazione individuali e collettivi. Io credo e noi crediamo (e questo è il punto di maggiore dissenso con l'impianto che viene proposto) che questa crisi democratica non sia compatibile con la scorciatoia e con la soluzione che avanzate, che non risolve peraltro, come ben si vede, nemmeno il tema dell'astensionismo elettorale, che proprio nelle Regioni dove il Presidente si sceglie con l'elezione diretta raggiunge le vette più alte, come dimostrano in tutta evidenza i dati sulla partecipazione al voto in tutte le recenti elezioni regionali. Questa incompatibilità a cui ho fatto riferimento, quella tra la semplificazione dell'elezione diretta e la crisi democratica, a mio avviso oggi vale sempre, anche quando il sistema prevede un rigido schema di pesi e di robusti contrappesi, come per esempio l'autonomia del Parlamento nei Paesi dove esiste il presidenzialismo, tanto è vero che proprio in quei paesi - negli Stati Uniti e in Francia - non a caso aumentano le contrarietà all'elezione diretta, forse anche perché si assiste a lacerazioni e conflitti sempre più insanabili tra i vari schieramenti. Ebbene, figuriamoci cosa potrebbe accadere qui da noi con questo premierato di cui parlate, che forza ancora di più l'equilibrio dei poteri e che rischia davvero di aprire la strada a derive potenzialmente letali in una situazione già significativamente compromessa. Eppure quello che è accaduto in Italia negli ultimi decenni avrebbe dovuto offrire molta materia da approfondire. Abbiamo assistito a una sorta di pensiero unico trasversale: l'idea, cioè, che il problema del Paese fosse tutto nella poca stabilità, nel numero troppo ampio di Governi e nella loro durata troppo breve, problemi reali, certamente, ma sui quali si sarebbe potuto intervenire in molti modi, senza stravolgere la Costituzione. Questa tesi, ripetuta ossessivamente nel corso degli anni, ha fatto però perdere di vista l'esistenza di un'altra grande questione, a nostro avviso ancora maggiore e dannosa, cioè la crisi della rappresentanza, che non solo si è accentuata nel tempo, ma che non ha visto su di sé l'attenzione che avrebbe invece meritato. La continua ricerca della stabilità ha significato il progressivo e continuo spostamento della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, con tutto quello che questo significa: l'abuso della decretazione d'urgenza, il continuo ricorso al voto di fiducia e il cosiddetto monocameralismo alternato. I poteri del Governo non solo non si sono ridotti, ma si sono dilatati con le Camere obbligate già ora ad una funzione spesso di sola ratifica e con i parlamentari di maggioranza, com'è tristemente accaduto nell'ultima legge di bilancio, gentilmente invitati a non presentare nemmeno emendamenti. allora a me e a voi: ci sarà un nesso fra tutto questo e quanto accaduto negli ultimi tre decenni o si tratta soltanto di un destino sfavorevole? Le leggi elettorali maggioritarie, i premi di maggioranza abnormi, che in altre stagioni sono stati chiamati giustamente leggi truffe, e poi con essi la personalizzazione, il rapporto disintermediato tra il capo e l'elettore e i nomi dei *leader* nei simboli dei partiti hanno avuto un ruolo in tutto questo? Hanno inciso, cioè, questi elementi sulla crisi della rappresentanza? Hanno avuto conseguenze, per esempio, nel ridurre la partecipazione al voto? Hanno frenato - o, viceversa, come penso io - hanno accentuato la crisi dei partiti? Dopo trent'anni si può provare a fare un bilancio o si devono sempre inseguire le magnifiche sorti e progressive, facendo finta di nulla? Lei, signora Ministra, dice che quello che oggi proponete voi lo ha proposto in passato anche la sinistra. potrei avere davvero buon gioco a dirle che quella non era la sinistra nella quale ho militato io. Le rispondo invece in un altro modo, perché non è questo il punto essenziale. Le rispondo dicendole che, quando questo è stato fatto, si è sbagliato *(Applausi)*, esattamente come si è sbagliato a modificare il Titolo V della Costituzione, aprendo la strada alla sciagurata autonomia differenziata. Questi errori però non giustificano certamente le scelte di oggi; anzi, se è possibile, le rendono ancora più gravi. La vostra riforma peggiorerà lo stato di salute della rappresentanza e quindi della democrazia. Voi dite che, con l'approvazione di questa riforma, non ci saranno più Governi tecnici. Ora le voglio dire una cosa su questo, perché per me è un argomento sensibile, per così Ministra, differentemente da lei e dal suo partito, noi in questi anni i Governi tecnici non li abbiamo sostenuti, né il Governo Monti, né il Governo Draghi. *(Applausi)*. Ma è davvero, questo che proponete voi, il modo corretto per evitare i Governi tecnici? Oppure anche su questo punto servirebbe una riflessione un po' più articolata? Perché ci sono stati questi Governi tecnici? Per le scelte individuali di un Capo dello Stato oppure di un altro o anche e soprattutto perché la debolezza della politica e dei partiti ha aperto loro la strada? E ancora, se questi Governi ci sono stati e se hanno visto il supporto di larghe o larghissime intese, che dovrebbero essere una rarissima eccezione e non certo la regola, non è stato perché anche in questo caso un pensiero unico, a volte molto trasversale, ha attraversato troppo spesso la politica italiana? Se volete impedire i Governi tecnici, piuttosto che farlo per decreto, lavorate per ricostruire la democrazia e i partiti, lavorate per ricostruire i pensieri lunghi. Non fatelo per decreto, perché davvero non serve a nulla. Piuttosto che seguire la scorciatoia dell'elezione diretta, bisognerebbe oggi alimentare i canali della partecipazione popolare e ripensare le funzioni della rappresentanza nella prospettiva di una rinnovata centralità parlamentare. Servirebbe innanzitutto una legge elettorale con un impianto rigorosamente proporzionale, senza distorsioni maggioritarie, in grado di rappresentare la plurale articolazione politica del Paese. Servirebbe cioè lavorare sulla ricostruzione dei corpi intermedi, sull'articolo 49 della Costituzione, sulla trasparenza dei partiti e dei finanziamenti alla politica sugli strumenti di contrasto alla degenerazione attuale, che abbiamo visto in tutta la sua vergogna consumarsi anche nei giorni scorsi: il contrario, cioè, di una visione verticistica che propone stabilità soltanto in apparenza. Ve lo abbiamo detto con i nostri emendamenti, signora Ministra. Ci sarebbero stati molti modi per scegliere un modello capace di coniugare stabilità e rappresentanza. Vi abbiamo proposto di intervenire con la sfiducia costruttiva, per esempio, senza stravolgere gli equilibri costituzionali e tenendo ben salda l'impostazione del Governo parlamentare, che invece andate a colpire. Allo stesso modo, vi diciamo invano di lavorare sull'attuazione della nostra Costituzione. Con questa vostra riforma, invece, si mette davvero in discussione il carattere pluralista della nostra democrazia. La composizione del Parlamento e finanche la sua durata finanche, dipenderanno dall'elezione del Presidente del Consiglio. Nessun'altra democrazia contemporanea vede oggi una tale concentrazione di potere nelle mani di una sola persona. Altro che facoltà di scelta da parte degli elettori: tutta la partecipazione del corpo elettorale si tradurrà in una sola chiamata al voto per via plebiscitaria, una volta ogni cinque anni; un'investitura che determina un indirizzo politico non modificabile, se non attraverso una nuova investitura,

per noi, per l'Alleanza Verdi e Sinistra, questa riforma non presenta margini di mediazione. La riteniamo sbagliata in radice, non solo quindi inaccettabile per ragioni di inadeguatezza tecnica e di difficoltà interpretativa, che pure abbondano, ma perché in contrasto con i principi che reggono le basi della nostra democrazia parlamentare. Per questo ci opporremo con tutte le nostre forze, perché abbiamo a cuore cuore la nostra Costituzione e non consentiremo a chi ne contesta il suo carattere antifascista di stravolgerla.

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 23 maggio. La seduta di oggi prosegue con il seguito della discussione generale del disegno di legge costituzionale in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. A partire dalle ore 15 avrà inizio la discussione del decreto-legge in materia di agevolazioni fiscali. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nella giornata di oggi si terrà la discussione sulla fiducia per la durata di un'ora. Le dichiarazioni di voto avranno inizio domani mattina alle ore 8,30. Seguirà la chiama. Sempre domani, alle ore 15, si terrà il *question-time* con la presenza dei Ministri dell'interno e per la disabilità. Il calendario della prossima settimana, con inizio martedì 21 maggio, alle ore 15, prevede il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, che proseguirà anche nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 maggio.

colleghi, vorrei chiedere, per suo tramite, Presidente, ai colleghi se hanno capito che il Paese è allo stremo, che ci sono emergenze molto gravi da gestire e parto, essendo il campo di cui più mi occupo, dalla sanità. Abbiamo le liste d'attesa più lunghe di sempre; oltre 4 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure perché non possono permettersi la sanità privata. Abbiamo un aumento della povertà assoluta, se i dati Istat ci dicono che oggi i poveri assoluti sono 5,7 milioni. Abbiamo Abbiamo oltre 4 milioni di italiani che lavorano, eppure non escono dalla soglia di povertà; li chiamiamo lavoratori poveri e per loro non volete il salario minimo. Abbiamo un'altra emergenza gravissima, che è quella dei morti sul lavoro: ogni giorno tre persone vanno al lavoro e non fanno più ritorno a casa. Abbiamo quel grande piano di investimenti che è il PNRR, che dovremmo gestire e di cui dovremmo utilizzare le risorse, e invece abbiamo speso meno del 4 per cento dei fondi dedicati alla sanità e meno dell'1 per cento di quelli dedicati alla formazione.

da settimane a parlare di una riforma costituzionale, quella del premierato, dopo aver lavorato per più di un anno a un'altra riforma, quella dell'autonomia differenziata, e io sono certa che, se chiediamo ai cittadini se queste sono emergenze per il Paese, non lo sono. *(Applausi)*. E non dite che era il mandato elettorale che avevate avuto, perché nel vostro programma elettorale, come hanno detto tanti colleghi che mi hanno preceduto, c'era l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, non del Presidente del Consiglio. Del resto, è stato depositato un disegno di legge, a prima firma Meloni, nella scorsa legislatura, che prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, e questo è il disegno di legge che è entrato anche nel vostro programma elettorale. Quindi non si tratta di un mandato elettorale che avete avuto. Inoltre, avevate fatto tante altre promesse che poi avete tradito: l'eliminazione delle accise sulla benzina, invece avete tolto gli sconti; il blocco navale per arginare il fenomeno migratorio, invece il numero degli sbarchi è il più alto di sempre; portare la sovranità italiana in Europa, mentre avete accettato un Patto di stabilità che ci costerà 13 miliardi all'anno di nuovi tagli e nuove tasse.

al Governo, a occuparvi di poltrone di terzi mandati dei governatori, a introdurre di nuovo i vitalizi alla Camera. Non volete vedere che c'è una questione morale urgente da affrontare e infatti state provando perfino a ridimensionare, mettendo in dubbio il lavoro della magistratura, ciò che sta avvenendo in Liguria. Entro ora nel merito di questa riforma costituzionale, partendo però da una cosa secondo me molto importante che ha detto un grande costituzionalista: le riforme non si possono fare nei momenti in cui non c'è pace sociale.

Quando si deve fare un intervento chirurgico a un organo vitale - penso al cuore, al fegato o al pancreas - si aspetta che il paziente sia in una condizione stabile, in una condizione stabile, in cui può sopportare quell'intervento. È la stessa cosa di quando un Parlamento decide di intervenire con una riforma costituzionale in un momento in cui non c'è pace sociale e non c'è giustizia sociale. *(Applausi)*. È esattamente la stessa cosa. cosa. Entriamo nel merito di questa forzatura che avete deciso di fare. Avete creato un pastrocchio; noi lo definiamo pastrocchio perché nelle settimane di discussione in Commissione sembrava che stessimo lavorando a un decreto milleproroghe: abbiamo visto inserire commi, virgole, taglia e cuci. Sembrava veramente un milleproroghe e alla fine è venuto fuori un pastrocchio pericolosissimo in cui si alterano tutti gli equilibri tra i poteri dello Stato. La nostra Costituzione prevede un contrappeso perfino per il Presidente della Repubblica, invece in questa vostra riforma non ci sarà nessun contrappeso. Il Presidente del Consiglio avrà poteri sproporzionati, eleggerà a traino il Parlamento, ancora non sappiamo con che percentuale di premio di maggioranza, perché questo l'avete rimandato a una futura ipotetica riforma della legge elettorale. Questo Presidente del Consiglio con a traino il Parlamento chiaramente influenzerà le elezioni del Presidente della Repubblica e quindi la nomina dei giudici della Corte costituzionale, quindi la nomina di tutti gli organi costituzionali. Non è più un premierato: rischiamo di arrivare a una vera e propria dittatura. dittatura. Non ci lamentiamo poi se a tutte le tornate elettorali l'astensionismo ormai è altissimo: un cittadino su due degli aventi diritto al voto decide di non andare a votare perché non si sente più rappresentato da questa politica autoreferenziale che, anziché occuparsi dei problemi del Paese, si occupa di tutt'altro. Non dite che darete più potere ai cittadini che potranno eleggere il Presidente del Consiglio, perché a questi stessi cittadini invece state chiedendo una delega in bianco, che bianco, che è anche quella che poi, dall'altro lato, state dando ai venti piccoli *Premier* che create con la riforma dell'autonomia differenziata.

finalmente viva? Perché non ci occupiamo di tutelare il diritto alla salute se ogni anno dobbiamo spendere oltre 4 miliardi di euro in migrazione sanitaria, visto che tanti cittadini sono costretti a lasciare i luoghi in cui vivono per andarsi a curare?

se nel ciclo scolastico di scuola primaria un bambino del Sud perde un anno di scuola? Perché non ci occupiamo di garantire veramente quella rimozione degli ostacoli per avere una vita dignitosa, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione? Questa riforma non servirà ad aumentare la stabilità del Governo. Vi avevamo dato le soluzioni e non potete dire che il MoVimento 5 Stelle ha fatto ostruzionismo, perché i nostri emendamenti si contavano sulle punta delle dita, erano pochissimi e tutti mirati. Vi abbiamo proposto di introdurre la sfiducia costruttiva, la fiducia a Camere riunite, il potere di revoca di un solo Ministro, la riduzione del *quorum* per i *referendum* abrogativi e un perimetro più ristretto per i decreti che oggi limitano invece l'attività del del Parlamento. Vi avevamo anche detto di rendere omogenei i Regolamenti di Camera e Senato sui disegni di legge di iniziativa popolare. Tutto è stato chiaramente bocciato, perché questo è il modo in cui vi comportate: dite di confrontarvi con le opposizioni, ma poi non lo fate. fate. Vi do una notizia perché evidentemente non ve ne siete resi conto: voi siete al Governo da quasi due anni e, anziché raccontare come volete risolvere i problemi delle persone, continuate ancora a dare la colpa a chi vi ha preceduto. Dite di essere patrioti, ma poi vendete gli *asset* strategici e presentate un DEF che è solo tendenziale.

profitti bancari. Ad esempio, volete dare la colpa al superbonus senza dire che il ministro Giorgetti è lo stesso che lo segue da almeno tre anni. E non basterà far finta di essere un'altra persona. Se anche chiamiamo Giorgia la Presidente del Consiglio, così come lei stessa chiede, questa Giorgia è la stessa che ha voltato le spalle ai poveri e ai malati che non si possono curare e al Sud, che ha svenduto alla Lega. È la stessa che ha accettato il Patto di stabilità e sta aumentando le spese in armamenti e difesa. Quindi, basta: basta dire bugie alle persone; basta cercare di nascondere le vostre bugie mettendo anche i bavagli alla stampa indipendente e censurando l'informazione; basta repressione violenta delle delle proteste dei nostri giovani che invece vanno sempre ascoltati. *(Applausi)*. Dovreste veramente cominciare a pensare come applicare la Costituzione. Non abbiate paura di identificarvi nei valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione. Voglio riprendere le parole di qualche giorno fa del Presidente della Repubblica, che ha richiamato proprio questo impegno dicendo che la nostra Costituzione è una conquista e va conosciuta, amata, difesa e vissuta ogni giorno per accogliere i nuovi bisogni, tutelare chi si trova ai margini, per avere cura soprattutto dei più fragili e affrontare le nuove sfide di convivenza e pace. questo impegno e questo obiettivo e continuerà a lavorare per tutelare soprattutto i più fragili e costruire una pace e una giustizia sociale. Tutto questo lo abbiamo inserito anche nel nostro programma elettorale per le prossime elezioni europee, perché noi rispondiamo davvero alle esigenze dei cittadini e al mandato elettorale dei nostri elettori. Voi state invece tradendo tutte le promesse che avete fatto.

Signora Presidente, signora Ministra, onorevoli senatrici e senatori, nell'intervenire oggi non vi nascondo che avverto appieno la discrasia tra la solennità della materia oggetto della nostra discussione, vale a dire le modifiche della Costituzione sul tema cardine del funzionamento della democrazia repubblicana, e l'inadeguatezza del testo su cui siamo chiamati a legiferare. Le molteplici ragioni di questa inadeguatezza sono state illustrate con argomenti convincenti da molti colleghi, oltre che dai più autorevoli costituzionalisti intervenuti negli ultimi mesi, sia nelle audizioni in Commissione che nel dibattito pubblico. Quindi, io mi soffermo solo su alcuni aspetti che ritengo descrivano l'irragionevolezza della proposta dell'Esecutivo. In primo luogo, mi soffermo sul metodo: si è lungamente e opportunamente denunciata una deriva mercantile nella condotta del Governo. Il testo che oggi prendiamo in esame in questa versione aggiornata, che in realtà è ancora più confusa e improvvisata delle precedenti, altro non è che il frutto di un mercanteggiamento tra le priorità del principale partito della maggioranza e la bandiera della Lega, quell'autonomia differenziata che porta con sé semplicemente la disgregazione dell'unità nazionale: da una parte, l'accentramento dei poteri, proprio di una cultura politica impregnata del decisionismo dell'uomo solo al comando e intrinsecamente allergica al parlamentarismo e, dall'altra parte, la scomposizione preordinata della pur perfettibile *governance* multilivello su cui è imperniata la nostra architettura istituzionale. Il tutto a meno di un mese da uno degli appuntamenti democratici più delicati dell'ultimo decennio. Così la Costituzione viene portata strumentalmente in campagna elettorale, arena di competizione interna tra i partiti del centrodestra. Opporsi a questo disegno è un tributo ai valori su cui è nata la nostra Repubblica, di cui fra pochi giorni, il 2 giugno, celebreremo il settantottesimo anniversario. Nel merito la proposta è un inganno nei confronti dei cittadini. Il messaggio che viene trasmesso al Paese è infatti generico e fuorviante. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio non determina necessariamente un rafforzamento del principio democratico, né tantomeno costituisce di per sé un elemento di stabilizzazione del sistema. Al contrario, in contesti politici frammentati e polarizzati come quello italiano, il premierato congegnato dal Governo finisce paradossalmente per configurarsi come un motore di destabilizzazione e di impoverimento delle istituzioni. Dunque, oltre alla più classica delle eterogenesi dei fini, ciò che ne deriva è una profonda contraddittorietà rispetto agli obiettivi dichiarati. L'elezione diretta del Capo del Governo, infatti, favorisce stabilità e dunque governabilità solo nelle società politicamente pacificate, con sistemi solidamente bipolari o addirittura bipartitici, come accade per esempio nel Regno Unito, dove l'elemento di equilibrio e razionalizzazione è rappresentato dalla presenza di partiti forti che conservano nella sostanza l'affidamento dell'elettorato. Al contrario, in scenari politici conflittuali qual è quello italiano, dove anche all'interno delle coalizioni di maggioranza e opposizione non c'è pieno allineamento politico e ideologico, l'elezione diretta non può che rivelarsi divisiva, tutt'altro che pacificatrice. la previsione della possibilità della sostituzione del Presidente del Consiglio eletto determina una potenziale conflittualità permanente nell'ambito della maggioranza. Altro che stabilità! Voi, Governo e maggioranza, fate confusione tra concetti: democrazia ed elezione diretta, infatti, non sono la stessa cosa. L'elezione dei soggetti titolari del potere pubblico è solo uno degli elementi caratterizzanti la democrazia e non esaurisce certo la categoria complessa di un sistema democratico che si fonda sull'equilibrio, su pesi e contrappesi, tutto ciò che questa riforma azzera. È infatti evidente che l'effetto trascinamento per cui dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio, senza neppure la previsione di una soglia che assicuri che la scelta sia affidata alla maggioranza degli elettori, si determina l'elezione di una maggioranza parlamentare, produce l'esito di scardinare l'equilibrio dei poteri, di alterare la funzione delle istituzioni di garanzia. In altri termini, da una elezione del *Premier*, che potrebbe essere determinata anche da una minoranza degli elettori, il trascinamento produrrebbe potenzialmente le elezioni della maggioranza parlamentare, del Presidente della Repubblica, della maggioranza dei componenti della Corte costituzionale e della rappresentanza parlamentare negli organi di autogoverno della magistratura. Vi rendete conto, Governo e colleghi della maggioranza, che si tratta di un effetto drammatico? Se pensate davvero di essere destinatari degli effetti di questa riforma, vi ricordo che mai negli ultimi trent'anni chi ha realizzato riforme o tentativi di riforme costituzionali ne ha potuto trarre beneficio, perché ha perso le successive elezioni o i *referendum* costituzionali. Invece voi state riproducendo l'errore per cui pensate che questo obbrobrio, che chiamate premierato, si applicherebbe solo alla vostra maggioranza e alla vostra Presidente del Consiglio. Questa è la verità. La seconda grande incoerenza, rispetto sia agli iniziali propositi del Governo, sia alle rassicurazioni fornite successivamente, anche in quest'Aula, dalla Presidente del Consiglio, investe la figura del Presidente della Repubblica. Formalmente, il disegno di legge non interviene a disciplinare le prerogative del Capo dello Stato. Nella sostanza, tuttavia, il premierato così disegnato finirebbe per depauperarne le funzioni e svilire quel ruolo di mediazione e garanzia esercitato in particolare in frangenti di *impasse* politica e istituzionale e ormai consolidato nella prassi e nelle convenzioni costituzionali. Riassumo: impoverimento delle prerogative e della centralità del Parlamento e contestuale esautoramento della figura del Presidente della Repubblica; il tutto ufficialmente nel nome di un modello di democrazia decidente, che, se passasse questa riforma, porterebbe un esito esattamente inverso: meno democrazia, con rappresentanza parlamentare fortemente decurtata, e minore carica decidente, con un sistema fisiologicamente incline al conflitto e alla parcellizzazione delle influenze, lasciato in balia del solo potere esecutivo e della sua per natura necessariamente oscillante forza nel Paese e presso la pubblica opinione. Sullo sfondo si ha una tendenza alla frammentazione che ormai investe la gran parte dei Paesi dell'Occidente. Non è un caso che, alla moltiplicazione delle sollecitazioni dal basso e all'incremento dell'indice di conflittualità sociale e politica, anche le democrazie di tipo presidenziale di più antica tradizione, come gli Stati Uniti e la Francia, faticano ad adattarsi, tanto da avallare, se non ricercare, una per molti versi inaspettata riconquista della scena da parte delle assemblee parlamentari. Dinanzi a tutto questo, chi ha a cuore l'interesse della Nazione, anziché inseguire la sirena autocratica, se proprio non vogliamo definirla autoritaria, del capo che comanda, con tutti gli altri a fare da contorno, dovrebbe lavorare in direzione di una riforma seria del potere esecutivo, che miri a legittimare una maggioranza capace di esprimere una guida affidabile e funzionale al conseguimento degli obiettivi di stabilità dei Governi e di efficacia dei processi decisionali. Vedete, noi vorremmo semplicemente questo: maggiore forza e stabilità degli Esecutivi e maggiore forza del Parlamento, ovvero della rappresentanza popolare che il Parlamento esprime, ovvero dei cittadini. Sono obiettivi possibili, se si dismette il populismo costituzionale e si assume un atteggiamento più concreto e pragmatico. *(Applausi)*. Cosa si può fare? Cosa proponiamo noi del Partito Democratico? Anzitutto, confermando l'assetto parlamentare della forma di governo, si deve rivitalizzare il legame tra rappresentati e rappresentanti, tra rappresentanti in Parlamento e cittadini, attraverso una legge elettorale che, abolendo definitivamente le liste bloccate, razionalizzi senza distorcere la volontà dell'elettorato, con attenzione alla parità di genere. Al tempo stesso, si può prevedere l'indicazione del nome del o della Presidente del Consiglio nella scheda elettorale, così da ottenere un'indicazione vincolante a garanzia tanto della coesione delle coalizioni, quanto del rispetto della volontà popolare. Si deve rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio, destinatario unico del voto di fiducia e dotato del potere di proporre la sostituzione dei Ministri. Si deve legare la possibilità di cambi di Governo alla sfiducia costruttiva, in modo da dare elasticità e adattabilità al sistema, senza minare la stabilità dei Governi. Infine, si dovrebbero modificare i Regolamenti parlamentari, per garantire l'attuazione del programma di Governo e il rispetto di tempi certi per l'approvazione delle leggi, senza dover alterare l'equilibrio dei poteri attraverso

Possiamo o potete ancora fare la cosa fondamentale quando si affronta una riforma delle regole della democrazia, delle regole in cui tutti i cittadini si devono poter riconoscere. Queste regole non possono essere espressione di una sola parte politica, ma devono rappresentare il risultato di un percorso che, anche partendo da elaborazioni distinte, porti alla più ampia condivisione parlamentare. Questa è l'unica via per evitare che le regole che reggono il funzionamento delle istituzioni democratiche, anziché essere il terreno all'interno del quale si dispiegano il confronto e anche il legittimo contrasto tra le parti politiche, divengano esse stesse l'oggetto di tale dialettica. Per un Paese come il nostro, dalle strutture democratiche e sociali particolarmente fragili, sarebbe davvero una sciagura. Come sarebbe una sciagura, simile a quella della legislatura 2013-2018 - stavolta sul versante della destra - la perdita di un enorme capitale politico investito su una riforma delle istituzioni. Io, in quella legislatura, anche dissentendo dal mio partito, non ho mai votato le leggi elettorali proposte a maggioranza ed ero consapevole del rischio di una riforma costituzionale destinata al *referendum* senza la ricerca della necessaria condivisione parlamentare. parlamentare. Fu un grave errore. Perché ripeterlo? Perché volete ripeterlo? Abbiamo già perso dieci anni dal 2013 e voi correte il rischio di perderne altri dieci, cosa che dobbiamo purtroppo augurarci se la riforma rimarrà questa. Dunque, il mio auspicio è che il Governo e la maggioranza, anziché ostinarsi nell'intento di stravolgere la Costituzione a colpi di maggioranza, tornino sui loro passi e cerchino la condivisione della larga maggioranza di questo Parlamento. Se non lo faranno, la nostra opposizione in Parlamento e nel Paese sarà tenace e durissima, così come esigono la storia della Repubblica e il sacrificio dei tanti che hanno combattuto per costruirla.

Ma non è la madre delle riforme in funzione dell'eletto: è la madre delle riforme in funzione dei cittadini elettori, che finalmente saranno chiamati a scegliere direttamente chi li potrà governare nei prossimi cinque anni. È quindi la più alta forma di democrazia che possiamo donare ai cittadini italiani nel momento in cui saranno loro a scegliere a chi affidare il destino di questa Nazione. Non è - come più volte è stato detto in quest'Aula - un baratto, perché la riforma costituzionale, l'autonomia differenziata e la riforma della giustizia erano iscritte nel programma di Governo del centrodestra. Si chiama coerenza, che in politica ha un solo significato *(Applausi)*, quello di rispettare il programma presentato agli elettori. È un sinallagma che prevede un programma concreto e poi il rispetto di ciò che si è detto agli elettori.

inneggiavano alla fine degli sbarchi, perché l'Italia non doveva essere il campo profughi d'Italia, salvo poi votare contro tutte le norme di questo Governo che invece vanno in quella direzione. Coerenza - lo dico agli amici del PD non è dichiararsi paladini della lotta all'evasione fiscale e poi strizzare l'occhio agli amici delle *lobby* delle *slot* *machine*. Coerenza è un'altra cosa: è il rispetto delle regole, è il rispetto di quello che si dice e di quello che si fa. Peraltro, noi doniamo al popolo il potere di scelta. Potere al popolo è una dizione che vi dovrebbe piacere; addirittura nel vostro campo largo sterminato c'è un partito che si chiama così. Pertanto, non dovreste neanche osteggiarle questa riforma e invece parlate di attentato alla Costituzione, di prevaricazione, di atto di forza, e poc'anzi ho addirittura sentito parlare di dittatura. E lo dite correndo

non c'è riforma elettorale che preveda l'elezione diretta che non sia un *unicum* in Europa e nel mondo: penso alla Francia, penso agli Stati Uniti d'America. In entrambi i casi, ma ne potremmo citare altri, ogni sistema elettorale, nel suo modo di essere, è un *unicum* e a noi questo non spaventa. Voi pensate che non si possa transigere dalla forma di governo parlamentare. Per noi questo non è un dogma; preferiamo l'elezione diretta, preferiamo dare voce ai cittadini. Ecco perché non ci spaventa l'elezione diretta del Capo del Governo, perché riteniamo che siano i cittadini sovrani a dover scegliere chi li deve governare e non gli inciuci di palazzo. Così vale anche per le prerogative del Capo dello Stato: quelle precipue, quelle effettive, quelle reali sono contenute nel Titolo II, Parte II, della Costituzione. Leggete l'articolo 87, che è rimasto intoccato da questa riforma:

Le altre, quelle previste dalla Parte III, attengono invece ai poteri del Governo e in quella parte il Capo dello Stato ha una funzione di coordinamento, non di preminenza.

voleva cambiare la forma di governo in senso semipresidenziale in maniera molto più invasiva di quello che stiamo facendo noi oggi, ma allora non gridaste allo scandalo. Per questo oggi non comprendo le

abbiamo ascoltato molti auditi, abbiamo acquisito molti documenti e alla fine il testo è stato modificato. In questa sede non entro nel merito di tutti gli emendamenti che hanno modificato il testo originario, ma intanto ricordo che è stata eliminata

Abbiamo misurato e calibrato anche dei contrappesi: penso al limite dei due mandati che dovrà avere il *Premier,* alla norma antiribaltone che consentirà di non cambiare in corsa le maggioranze. quindi, di riforme sostanziali con pesi e contrappesi. Quanto al potere di scioglimento, al potere di scioglimento, è ovvio che esso ricada nelle mani di chi è eletto dal popolo. Quando si prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, è lui ad avere la fiducia degli elettori. E, quando quella fiducia manca sia perché non c'è più fiducia nell'Assemblea del Parlamento, sia perché manca proprio l'afflato con i cittadini - è giusto che sia lui a decidere di andare a casa e di ridare la parola al popolo, perché questa si chiama democrazia. Comprendo che per voi questo non vada bene, anni siete abituati a governare senza essere eletti grazie agli inciuci di palazzo, che con questa riforma non saranno più possibili. La riforma mira a rendere stabile e governabile il nostro Paese che, a causa delle crisi di Governo che ci hanno visti visti coinvolti negli ultimi anni, ha speso oltre 200 miliardi solo negli ultimi dieci anni; abbiamo perso 200 miliardi nel bilancio dello Stato a causa delle crisi di Governo e questo non ce lo possiamo più permettere. Garantire stabilità e governabilità significa anche essere attrattivi per gli investitori esteri, ma anche per i nostri investitori interni; significa dare una speranza a questo Paese. Siamo convinti che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio garantirà agli italiani una maggiore vicinanza con le istituzioni; consentirà loro di essere più vicini a chi eleggono ed eliminerà quelle storture che abbiamo visto negli ultimi anni e che hanno visto purtroppo il Parlamento oggetto di mercanzia e scambi, anche poco eticamente validi, nella scelta di chi doveva poi salire sullo scranno di Palazzo Chigi. Noi voteremo quindi convintamente a favore di questa riforma. Chi mi succederà mi succederà della mia parte politica saprà ancor di più portare alla vostra attenzione le motivazioni valide per cui anche voi dovreste guardare in maniera diversa questo provvedimento, che noi invece appoggiamo e che per noi è e anzi resta la stella polare del nostro mandato elettorale. *(Applausi)*.

quelli come me, entrati in Parlamento nella XVII legislatura, quella data non dimenticheranno - quando l'allora rieletto Presidente della Repubblica, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica italiana, Giorgio Napolitano giurava davanti alle Camere riunite pavesate a festa come quando il Presidente della Repubblica giura. Quel discorso di Giorgio Napolitano fu uno schiaffo a mani aperte sul volto di quel Parlamento che lo aveva appena rieletto. Il presidente Napolitano era molto anziano, aveva già preparato gli scatoloni, era pronto a passare la mano, ma quel Parlamento eletto da così poco non era riuscito ad adempiere al suo dovere di trovare un nuovo Capo dello Stato. E il Presidente della Repubblica non mancò di farcelo notare e ci chiese a viva voce, tra gli applausi scroscianti del Parlamento, di arrivare a una riforma costituzionale. Io credo che quel monito del Presidente della Repubblica, che ormai risale a più di undici anni fa, sia ancora valido e noi dobbiamo prendere atto, come Parlamento, che la riforma costituzionale è ormai non più procrastinabile. Questo perché l'assenza di un meccanismo istituzionale che funzioni non è neutra. Voglio dire che il passaggio del tempo rende la situazione sempre più grave: non fare la riforma in una situazione conclamata di malfunzionamento istituzionale produce danni che si radicano, che si approfondiscono, che peggiorano. Il mio grande timore è che anche in questa occasione, signora Ministra, noi perdiamo la *chance* di dare a questo Paese delle istituzioni funzionanti, perché - diciamocelo - allo stato

il fatto che le Camere siano umiliate quotidianamente - noi, cari colleghi e colleghe, in questa Camera e nell'altra Camera spesso, ci limitiamo a ratificare atti approvati dall'altro ramo del Parlamento - dimostra come siamo arrivati a una forma di monocameralismo alternato che, signora Ministra, in Costituzione non c'è, la Costituzione materiale vivente non assomiglia più a quella che è stata scritta. Anche l'unica riforma fatta negli ultimi anni, quella della riduzione del numero dei parlamentari, ha ancor più umiliato il Parlamento. Queste Camere funzionano molto peggio oggi di quanto non funzionassero quando erano a pieni ranghi, non foss'altro per il fatto che i Regolamenti sono rimasti gli stessi e noi, con un terzo di forza lavoro in meno, dobbiamo fare lo stesso lavoro di prima e oggettivamente chiunque si occupi di processi organizzativi deve riconoscere che questo è materialmente impossibile. La prima cosa che vorrei dire è che non è lecito per nessuno buttare la palla in tribuna e perdere questa occasione. Non possiamo fare come Bertoldo che, condannato a morte, disse "Sì, basta che mi fate scegliere l'albero a cui impiccarmi" e rimandò la cosa *sine die*. La riforma costituzionale va ed è per questo, signora Ministra, che noi abbiamo dato, sin dall'inizio, un segno di apertura nei suoi confronti. Pensiamo che, chiunque sia a governare, la riforma non possa essere più procrastinata, proprio perché - come dicevo - il passaggio del tempo lascia dei problemi aperti che peggiorano la situazione. secondo punto, il collega Della Porta prima diceva che non dobbiamo avere paura di forme presidenzialistiche e personalmente lo condivido. Esistono fior di Paesi democratici che hanno forme di governo presidenziali e non dobbiamo averne paura perché, se decidiamo di avere una forma di governo di questo genere va bene, si può fare. L'importante è che sia fatta bene. Non ci nascondiamo - come ha fatto prima il collega Scarpinato - dietro il totem della Costituzione immutabile. Francamente fa anche un po' sorridere il MoVimento 5 Stelle che si fa paladino della Costituzione, essendo nato su un meccanismo eversivo della Costituzione: il superamento della democrazia rappresentativa e l'adozione della democrazia diretta, per cui il parlamentare non è altro che un portavoce, sono evidentemente eversivi del contenuto, contenuto, del nucleo della Costituzione. Quindi, diciamo che certe posizioni fanno un po' sorridere. Ciò che però è importante, signora Ministra, è che le cose siano fatte bene e purtroppo questo disegno di legge costituzionale non ci restituisce una forma istituzionale che sia più efficiente. Io glielo chiedo direttamente: in scienza e coscienza - come si dice - lei si sente di dire che ci consegna un meccanismo istituzionale meglio funzionante oppure no? In questo In questo disegno di legge di riforma c'è davvero una serie di problemi molto grossi. Noi abbiamo da sempre sostenuto il modello del sindaco d'Italia proprio consapevoli del fatto che il meccanismo di elezione dei sindaci nei Comuni superiori a 15.000 abitanti oggi è il miglior sistema sistema elettorale e istituzionale che abbiamo nella Repubblica; è quello più riconosciuto dai cittadini e, anzi, la invito, signora Ministra, a vigilare che la sua maggioranza non modifichi la legge sui sindaci dei Comuni fino a 15.000 abitanti, come vuol fare. Quella legge,

proprio perché esiste il ballottaggio. Non esiste mai un sindaco di minoranza. Non esiste un sindaco, come quello che la sua maggioranza vorrebbe introdurre, eletto con il 40 per cento dei voti e, quindi, rappresentativo di una minoranza dei cittadini. Il sindaco è eletto sempre dalla maggioranza ed è per questo che noi le chiediamo quale diavolo sarà la legge elettorale. Il collega Della Porta diceva che la legge elettorale deve essere una conseguenza della riforma costituzionale.

legge elettorale deve essere fatta in un certo modo, cioè che deve assicurare un premio di maggioranza, allora ci dovete dire anche come sarà fatta questa legge elettorale. Altrimenti noi votiamo sulla fiducia una legge elettorale che verrà, della quale non conosciamo, per esempio, se avrà una soglia minima. Il premio di maggioranza lo prenderà qualcuno che ha preso il 26-27 per cento Ci sarà il ballottaggio? Ci garantite che il Primo Ministro eletto sarà rappresentativo della maggioranza assoluta dei votanti, sebbene al secondo turno, come per esempio accade in Francia?

- diventando irriconoscibile rispetto alla volontà degli elettori. Già i cinque anni di oggi sono più veloci e dilatati dei cinque anni del 1948 o degli anni successivi, perché il tempo, in questa fase storica, corre molto più veloce.

Se gli elettori hanno scelto un Presidente del Consiglio, non può succedere improvvisamente che ve ne sia un secondo. Questo è un elemento chiaramente poco coerente. Tra le altre cose, quello che secondo me è importante sottolineare è che questa riforma non tocca poi tutta una serie di altre questioni. Oggi il collega Parrini parlava dell'eccesso di decretazione d'urgenza, all'esempio che facevo all'inizio parlando del bicameralismo paritario. Come si fa ad affrontare una riforma costituzionale senza toccare l'elefante nella stanza soprattutto in questa stanza - che è la diminuzione di poteri e la mortificazione del Parlamento? Signora Ministra, io ho guardato con simpatia e con apertura al suo tentativo e tuttora lo faccio. Le chiedo però di consegnarci una Costituzione che funzioni e delle istituzioni che funzionino meglio. Il rischio che stiamo correndo è di rispondere all'appello del 2013 del presidente Napolitano e dare a questo Paese delle riforme, ma consegnare al Paese delle istituzioni che funzionano peggio di quanto non funzionassero nel 2013.

non è nient'altro che l'ultimo capitolo, quello più recente, di una favoletta, una storiella, chiamiamola nenia, che ci raccontate ormai negli ultimi mesi. Questa riforma, il premierato, è da intendersi come parte di un progetto molto più grande, anche più dannoso, che ben rappresenta il vostro modo di intendere il funzionamento delle istituzioni e la gestione del potere. Da mesi ascoltiamo quindi quella lieta novella della giovane donna che fa politica da quasi trent'anni e che è giunta al successo contro ogni pronostico e con il fato avverso. Secondo questa fiaba, colleghi, quella giovane e sempre sottovalutata ragazza di periferia, dopo tante peripezie, finalmente arriva alla guida del nostro Paese. Ci arriva, si siede sul suo scranno e ci dice: bene la donna, benissimo la mamma, ma da questo momento in poi chiamatemi "il Presidente". Insieme a lei vediamo Ministri che nella stessa giornata, paradossalmente, riescono a incassare il diniego di firma sul loro ultimo decreto, mentre contemporaneamente parlano di un fortunato e siccitoso Sud; altri Ministri indagati per truffa aggravata; Sottosegretari costretti alle dimissioni perché eccessivamente appassionati d'arte e che, al pari di qualche dipinto, troveranno certamente riparo all'estero, visto che si candidano all'estero; qualcun altro, che ormai è all'ultima spiaggia, non fa altro che parlarci di un fantomatico ponte. Incompetenti, inadatti e pure indagati, perché c'è gente tra di voi che, pur avendo patteggiato per corruzione, continua a candidarsi e viene chiaramente, fieramente

che non trova lavoro, che di lavoro muore o che spesso, sì, lo trova, ma è sottopagato, quindi abbiamo cittadini sfruttati (ma a voi la legge sul salario minimo non piace); famiglie che non riescono a pagare i mutui alle banche, quelle banche che anche grazie a voi diventano sempre più ricche. Mentre c'è il rischio di una guerra mondiale, voi continuate voi continuate ad inviare armi e a farvi prendere per mano dall'America. Su migranti e benzina in questo contesto preferisco non infierire. Torniamo ai vostri temi: parlate di merito, parlate di merito, ma la gente non riesce a mandare a scuola e all'università i propri figli. Basta con la storia "diteci voi che cosa avete fatto: i banchi a rotelle?". Siete voi invece che dovete dirci che cosa state facendo, facendo, perché noi qualcosa l'abbiamo fatta. Lo dico per suo tramite, Presidente, anche per lasciare agli atti una correzione a quanto detto dal senatore Scalfarotto: noi la Costituzione l'abbiamo difesa; in tempi non molto lontani da questo, siamo saliti sui tetti di Montecitorio per difendere la Costituzione *(Applausi)*, che stava per essere svergognata dal suo attuale capo politico. Altra cosa, giusto per parlarci e farci intendere: noi in Costituzione abbiamo inserito la tutela dell'ambiente. Ecco che cos'è per noi la Costituzione: una bellissima Costituzione da tutelare e, semmai, migliorare e aggiornare con i nuovi temi attuali. Insomma, voi di fronte alla drammaticità della situazione che viviamo che cosa proponete? Quali sono le vostre soluzioni? Riattaccate con il solito ritornello della madre, ma stavolta è la madre di tutte le riforme: il premierato. È bene ricordarlo: nel vostro programma elettorale non c'era, perché c'era il presidenzialismo. Premierato, sì, perché la Presidente di cui ho parlato poco fa finora ha avuto troppi ostacoli e quindi è meglio assicurarsi mano libera in futuro. Cosa vorrà fare ancora? Nominare ministro un cavallo? l'altro giorno, in un convegno intitolato, immagino con la vostra consueta ironia, «la Costituzione di tutti», il presidente Meloni ha detto che questa riforma a lei non serve e che la fa per tutti noi, la fa per il Paese. Un premierato inteso in questi termini, come voi l'avete strutturato in questo disegno di legge, certo che non serve, perché non raggiunge minimamente l'obiettivo in termini di maggiore governabilità. E allora, vedete, la democrazia è una cosa assai complessa: è fatta di equilibri davvero molto delicati. Voi invece andate a creare un *unicum* dagli effetti nefasti, minando alla base il principio della separazione dei poteri. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che prevedete all'articolo 5, svilisce tra le altre cose il ruolo del Parlamento. I parlamentari, stando infatti all'attuale legge e probabilmente anche quella che sarà, quella che avete in mente di fare, saranno eletti a totale strascico del Presidente, dando vita ad un sistema di rapporti tra potere esecutivo e legislativo che non esiste in nessun Paese del mondo. In altre parole, le due Camere saranno sottomesse rispetto al vertice di Governo, creando in tal modo una evidente, direi pericolosa, concentrazione di potere nelle mani dell'Esecutivo. ulteriore mortificazione del Parlamento arriva con l'articolo 7 del vostro disegno di legge che modifica l'articolo 94 della Costituzione. Se la fiducia iniziale al Governo viene negata, il Parlamento verrà automaticamente sciolto. Allo stesso modo, il Presidente del Consiglio potrà imporre lo scioglimento delle Camere, qualora gli venga negata la fiducia durante il corso di una legislatura. Ma davvero avete il coraggio di affermare che il potere del Parlamento resterà intatto? Ne siete certi? Riuscite a leggere quello che scrivete? La stessa cosa dite, mentendo spudoratamente all'Assemblea e al Paese, ai cittadini che sono fuori da quest'Aula, dei poteri e delle prerogative del Presidente della Repubblica. Noi sappiamo benissimo che non è come dite voi, perché la Presidenza non avrà più prerogative, ma solo vincoli. E questo a serio danno delle proprie alte funzioni di arbitraggio e garanzia, e con una posizione che risulterà in ombra e marginale rispetto a quella del Presidente del Consiglio, anche per sbilanciamento di investitura. Colleghi della maggioranza, voi difettate di forma e sostanza, a mio avviso. Avete la malcelata ambizione di riscrivere la storia del Paese, ma siete stati votati ed eletti per immaginarne il futuro, per scriverne il futuro, il domani, secondo le vostre intenzioni. In entrambi i casi, però, alla vostra penna manca il necessario inchiostro e a voi l'essenziale grammatica istituzionale e per tale motivo sul foglio dell'Italia - un po' più Ungheria che avete in mente, ad oggi c'è solo uno scarabocchio informe. Siete annebbiati dal potere e dalla vostra innata voglia di rivalsa. Nell'antichità, Presidente, voglio ricordare questo, dinanzi al Sommo Pontefice appena eletto, il cerimoniere bruciava un batuffolo di cotone ripetendo per tre volte la frase: *sic transit gloria mundi*, proprio a sottolineare la caducità delle cose umane e quindi del potere. Ora, voi siete stati anche bravi ad accendere un bel fuoco, una bella fiamma, ma quando questo fuoco si spegnerà, all'auspicabile sussulto della vostra coscienza politica e istituzionale dovrete farvi una domanda. Sarà la stessa domanda che si faranno i cittadini là fuori. Quando vi chiederete faranno i cittadini là fuori. Quando vi chiederete che fine hanno fatto la libertà di stampa e d'opinione; quando vi chiederete ancora che fine ha fatto la lotta alla corruzione; quando vedrete gli evasori godere dei vantaggi loro assicurati; quando non troverete più i mezzi fondamentali di contrasto alla criminalità, come le intercettazioni; quando vedrete i colletti bianchi approfittare dell'abolizione del reato d'abuso d'ufficio; allora, quando toccherete con mano la distruzione del sistema sanitario nazionale a favore dei privati; quando vedrete un Paese dilaniato e una persona sola al comando, che vi racconta cosa più vi piace e che tiene il Parlamento in pugno; insomma, solo allora vi chiederete: ma come siamo finiti così in basso? E quando lo farete, perché lo farete, in quanto sarete chiamati a farlo, come risposta scrivete solo «Giorgia». siamo ormai quasi al termine di questa discussione generale su un provvedimento tanto importante decisivo per il nostro assetto costituzionale e di Repubblica parlamentare. Aggiungo solo qualche considerazione a quelle già fatte dai colleghi del Gruppo Partito Democratico e da tanti colleghi dell'opposizione. Non mi voglio soffermare per l'ennesima volta sullo scambio fatto nella maggioranza, tra ragioni politiche e fini elettorali, così come non mi soffermerò - lo abbiamo già sentito tanto - sull'assenza totale di confronto di merito, a partire dal lavoro che è stato fatto in Commissione, fino ad arrivare a quello di quest'Aula, che è sotto gli occhi di tutti. Proverò Proverò a fare uno sforzo e parlerò a partire non dal mio o dal nostro punto di vista, ma da quello della maggioranza, provando ad assumere cioè il suo punto di vista. Lo voglio fare per affermare una pratica diversa, denunciare la mancanza di rispetto e di dialogo, vorrei che provassimo a praticare un modo diverso. Parto ovviamente da me e provo ad assumere il punto di vista della maggioranza. La maggioranza sostiene di aver varato un disegno di legge che, sostanzialmente, ha due grandi, importanti e preziosi obiettivi, primo tra tutti la governabilità e la stabilità dei Governi, lamentando e ricordando a tutti noi che cosa è successo in questi anni,

questo assunto; certo che stabilità e governabilità possono essere beni preziosi. Starei sempre attenta però a fare una distinzione, come pure ci hanno ricordato importanti e autorevoli esperti di diritto costituzionale e costituzionalisti del nostro Paese: non è questo

voi pensate davvero che con questo disegno di legge perseguirete di più e meglio questi due principi? Mi permetto di esprimermi molto sommessamente, con pacatezza e con rispetto delle posizioni degli altri, senza gridare in qualche modo a un atteggiamento sovversivo. Voglio stare al merito e vi dico che, secondo me, non solo questo provvedimento è totalmente inefficace rispetto all'obiettivo che si propone, ma è anche purtroppo un grande *bluff* e rischia di essere una presa in giro nei confronti dei cittadini. Perché? stabilità e governabilità, intanto dovremmo sempre guardarci attorno e pensare che la scelta fatta nel merito e nel contenuto da questo provvedimento è assolutamente solitaria nel contesto mondiale. Chi l'ha perseguita, che pure poteva avere le nostre stesse ragioni, evidentemente ha fatto un passo indietro, fatto un passo indietro, rispetto anche a un tema di sistema che era abbastanza simile a quello che abbiamo adesso di fronte dal punto di vista della legge elettorale. Su questo però tornerò dopo. Alla fine voi provate a perseguire la stabilità e la governabilità solo irrigidendo il sistema,

sostanzialmente dicendo al Parlamento: non sarai più tu a decidere.

questo principio non sarà perseguito. Voglio fare un ulteriore sforzo. Ci dite che noi critichiamo. Noi non abbiamo soltanto criticato, perché in Commissione abbiamo anche provato a fare tante proposte di merito.

non solo elegge direttamente il Presidente del Consiglio, ma mette in discussione un sistema parlamentare senza poi riconfigurare - come diceva stamattina il presidente Casini - pesi e contrappesi, avremmo potuto pensare che ci fosse qualche altro istituto a garantirlo. Abbiamo detto che la sfiducia costruttiva era sicuramente uno strumento

dicendogli: bene, tu vuoi cambiare Governo perché non pensi più che questo Presidente del Consiglio ti rappresenti? Trova un'altra soluzione: assumiti le sue responsabilità, cerca al tuo interno, nelle forze che sono espresse dentro l'Assemblea parlamentare, un'altra sintesi e offri al Paese un'altra soluzione, perché il Paese non può pagare le tue incapacità o le tue sofferenze. Allora, noi vi abbiamo data un'altra strada, ve l'abbiamo indicata. Non ci siamo limitati solo a dire che non va bene quello che ci indicate ed è totalmente inefficace rispetto alla volontà o all'obiettivo che dichiarate di voler perseguire.

i cittadini scelgono una volta, presumibilmente ogni cinque anni, a questo punto, se dovesse essere perseguito il tema della stabilità e della governabilità, quindi anche della lunghezza e della durata dei Governi e delle legislature (ma io ho A quei cittadini viene chiesta sostanzialmente una delega in bianco: votate, esercitate il vostro sacrosanto diritto di voto (per fortuna, è sancito dalla Carta costituzionale il diritto al suffragio universale: votavano prima, i cittadini, e voteranno oggi, non è che voteranno soltanto con la vostra riforma) e poi a tutto pensiamo noi;

come impatta sul resto del sistema, quindi servono garanzie, pesi, contrappesi e bilanciamenti per evitare la concentrazione. Non è questo però il centro del ragionamento che voglio fare: quello che voglio dire, invece, è come questi cittadini da due punti di vista partecipano effettivamente. Innanzitutto, quali cittadini riescono poi effettivamente a contare, perché certo il voto lo esprimono tutti, ma poi il voto di chi conterà? Quale voto sarà rappresentato in queste Aule parlamentari? Quale voto peserà? Allora, innanzitutto va fatto un ragionamento: i cittadini qua cosa scelgono? Non ci avete fatto capire con quale legge elettorale; ve lo abbiamo chiesto in tutti i modi: non mettete solo un riferimento, la legge elettorale deve camminare di pari passo con la riforma.

Con il sistema di premio che avete configurato all'interno del disegno di legge in esame, ovvero un premio che può arrivare al 51 per cento senza prevedere nessuna soglia, così come prescrive la Carta costituzionale, noi potremmo trovarci che quella

avrà espresso non solo la maggioranza, ma tutto: avrà eletto il Presidente della Repubblica, gli organi di garanzia, i giudici della Corte costituzionale, ossia tutto.

nel Parlamento, nel confronto parlamentare, nella dialettica e nel riconoscimento del pluralismo c'è il sale della democrazia nel senso più profondo del termine, per come l'hanno pensata e voluta i nostri Padri e Madri costituenti.

limiti; invece la nostra Carta costituzionale, votata da tutte le forze antifasciste nel dopoguerra, dimostra la sua solidità, probabilmente anche per questo.

e, insieme ad essa, forse mettere al centro la partecipazione dei cittadini significava finalmente dare seguito a una parte della Costituzione ancora inattuata, cioè l'articolo 49, perché attraverso la riforma dei partiti si dei partiti si interviene su come essi scelgono e indicano quei nomi tra i quali i cittadini dovranno scegliere anche il candidato P*remier.* Come arrivano a scegliere le *leadership*? I partiti al loro interno che vita democratica hanno oggi? Come compongono le liste di candidati in un sistema elettorale che noi ci auguriamo possa essere, per esempio, più sui collegi e che abbandoni il sistema delle liste bloccate? Abbiamo proposto una nuova legge elettorale; tuttavia, a fianco a essa, che doveva essere definita prima e contemporaneamente, vi abbiamo detto di mettere mano all'articolo 49. *(Applausi)*. Questo significava per noi perseguire con coerenza gli obiettivi che dichiaravate di voler perseguire e, soprattutto, rispondere alla crisi di democrazia e di partecipazione che oggi esiste e che è un grave, gravissimo, problema. Si pensava di affrontare così il buon funzionamento del Parlamento,

legge elettorale e la riforma dell'articolo 49 erano per noi dei capisaldi. Concludo con un riferimento all'articolo 1 della Carta costituzionale, al secondo comma: «La sovranità appartiene al popolo che la esercita». Esercitare è un verbo sul quale dovremmo riflettere tutti, non è un termine scelto a caso dai nostri Padri e Madri costituenti, per cui ogni parola ha avuto un senso: non è che i cittadini affidano o delegano a qualcuno, ma esercitano la sovranità. Questo significa che la esercitano tutti i cittadini, quindi dobbiamo rappresentare tutti dentro queste Aule parlamentari e l'unico che lo può fare è il Parlamento. Significa riconsegnare un protagonismo, quindi perseguire l'obiettivo di una sana, vera e autentica partecipazione con scelte più coerenti e coraggiose rispetto agli obiettivi che vi eravate prefissati. Non cogliete nessuno di quegli obiettivi, soprattutto indicate strade che, oltre a essere totalmente inefficaci per noi, rischiano di essere pericolose per il nostro sistema democratico.

per il nostro popolo di esercitare la sovranità che gli appartiene, se non quello di scegliere da chi essere governato e quindi a chi affidare un indirizzo programmatico coerente con quello che il cittadino e l'elettore ne

uno degli elementi importanti e fondamentali del nostro programma e delle nostre stesse idee ed è stato frutto di un lunghissimo, partecipato

nonostante quello che alcune volte ascoltiamo in quest'Aula, della compattezza e della determinazione della maggioranza, ma anche della grande capacità di ascolto, innanzitutto da parte del Governo, del ministro Casellati e di tutta la maggioranza. Ricordiamo infatti che, all'esito

in questo dibattito, più o meno gli stessi temi che sono stati riproposti costantemente, ovvero l'accentramento dei poteri nelle mani del Presidente del Consiglio,

Ovviamente sono accuse che abbiamo potuto e possiamo confutare una per una, perché, come altri hanno ricordato, i poteri del Presidente della Repubblica delineati nell'articolo 87 sono assolutamente invariati, anzi; un emendamento del presidente Pera all'articolo 89 della Costituzione non prevede la controfirma dei Ministri per alcuni atti del Presidente della Repubblica. Quali sono allora - perché questo poi è l'elemento cruciale in qualche modo, attraverso un premierato all'italiana quale quello che stiamo proponendo, vengono meno? Sono funzioni di fatto esercitate negli anni durante alcune crisi parlamentari, che sono esattamente una delle motivazioni per cui da tanti anni tante forze politiche, sicuramente anche quella della quale rappresentiamo una tradizione, quella della destra politica italiana, ma non solo, hanno proposto hanno proposto una modifica dell'assetto istituzionale per evitare che i Governi vengano scelti in Parlamento anche contro le indicazioni e gli indirizzi espressi chiaramente dal popolo italiano, E allora se viene meno quel ruolo che, per supplenza e per volontà di risolvere delle crisi, alcuni Presidenti della Repubblica hanno svolto, il nostro obiettivo è di far venir meno quel *vulnus* che aveva reso necessario quell'intervento. Quale sarebbe allora la proposta delle opposizioni? Teniamo in vita quei poteri perché dobbiamo tenere in vita quelle difficoltà e quelle problematiche che spesso hanno portato il Parlamento ad essere assolutamente più lontano dagli elettori e dai cittadini.

Ecco, questo significa accettare implicitamente che noi siamo qui per difendere non gli interessi, gli indirizzi e le necessità del popolo italiano, ma la nostra poltrona. Dovremmo aver paura infatti di mandare a casa un Governo che non esprime gli indirizzi

che possano essere percepite e comprese dagli italiani e che possano avvicinare il Parlamento agli italiani e non allontanarlo come negli anni è successo. Questo è un po' il cuore della nostra riforma. Noi vogliamo che l'attività del Parlamento possa essere verificata, come quella del Governo. Noi vogliamo in questo senso un avvicinamento. Certo, ci sono poi altri interventi

e con questo sistema. Sul tema dell'accentramento dei poteri abbiamo sentito un po' di tutto, anche la lezione di storia della senatrice professoressa Floridia, che ci ha parlato dell'evoluzione dalla repubblica verso il cesarismo, poi verso l'impero. Diciamo però che, pur senza essere professori di storia, non ci risulta che né Giulio Cesare né Ottaviano Augusto siano stati eletti dai cittadini e noi qui stiamo portando avanti una riforma il potere lo dà ai cittadini, che saranno liberi di scegliere da chi essere governati. Questo tema, che sembra molto distante da molte delle forze di opposizione - non tutte fortunatamente, ma la maggior parte - è per noi importante, importante, perché non diamo più poteri al Presidente del Consiglio, se non quello di prendere atto di non avere più la sua maggioranza, o quello - che, incredibilmente, fino ad oggi non c'è stato - di revocare un suo Ministro (un membro della sua squadra che magari non lavora bene, lavora male o addirittura lavora contro gli indirizzi del Governo è doveroso che finalmente con questa riforma possa essere indirettamente evocato). però qualcuno qui - in questo caso, mi riferisco soprattutto al Partito Democratico - si è talmente abituato negli anni a governare anche senza aver ricevuto il mandato dai cittadini che ha preoccupazione verso una riforma che non fa altro che dire che i cittadini sceglieranno da chi essere governati. Questo è un punto che per noi è molto importante. *(Applausi)*. Non ci sono contrappesi che vengono meno. I contrappesi sono ben presenti nella Costituzione, la innervano, la costituiscono, la rappresentano in tutte le sue parti e non vengono intaccati. Comunque a tale riguardo abbiamo anche approvato un ordine del giorno che parla di statuto dell'opposizione, e i Regolamenti potranno e dovranno

rivendicando anche il legittimo ostruzionismo, che la sua forza politica e l'opposizione si opporranno con tutte le forze a questo provvedimento. Noi invece di questo provvedimento siamo orgogliosi ci impegneremo a sostenerlo con tutte le nostre forze, a difenderlo e a consegnarlo, probabilmente attraverso un *referendum* che è evidente che ci potrà essere, alla scelta del popolo italiano, che potrà giudicare su questo. Non dovrà giudicare

il nuovo assetto costituzionale che noi proponiamo li possa rappresentare, possa dare loro un maggiore protagonismo, possa dare maggiore stabilità, maggiore governabilità e anche un risvolto economico importante, perché se l'Italia ha il debito pubblico che ha è anche perché l'instabilità politica si paga. paga. Stiamo vedendo, al contrario, quanto invece i mercati e il mondo economico stanno apprezzando la stabilità che in questo momento c'è perché si sono determinate delle particolari condizioni elettorali che hanno consentito a Giorgia Meloni di vincere in modo netto e quindi di governare con stabilità.

è quello che uno non si aspetta: è la Costituzione stessa, con l'articolo 138 che i Padri costituenti, certamente saldi nei princìpi costituzionali e repubblicani, per noi sacri, avevano delineato. Avevano infatti immaginato che la Costituzione e l'assetto istituzionale, che allora doveva essere quello per la situazione dell'Italia, si sarebbe potuto mutare. Noi vogliamo fare esattamente questo, perché se la nostra Costituzione è ispirata ed innervata dal principio della libertà, è vero pure, come diceva Gaber, che la libertà è partecipazione, e non c'è migliore partecipazione per i cittadini di far scegliere loro da chi essere governati. *(Applausi)*.

*dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro delle imprese e del made in Italy* «Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,

onorevoli colleghe e colleghi, ringrazio il signor Ministro, che è presente in Aula, ci segue in questo dibattito e ci ha seguito in tutti i lavori della Commissione. È stato un piacere, insieme al relatore, senatore Balboni, poterci confrontare su questa riforma, perché, come ho detto in più di un'occasione, sicuramente stiamo compiendo un percorso che segnerà la storia della nostra Repubblica, la storia dei nostri giorni, la nostra storia, quindi è un piacere avere anche la consapevolezza di esserne interpreti e attori

del nostro sistema parlamentare e le sue particolarità, compresi gli elementi che lo hanno messo in crisi, che evidentemente non lo fanno funzionare più come era previsto che funzionasse nella nostra Carta costituzionale. Carta costituzionale che è di mirabile bellezza, invidiata da tutti i Paesi e da tutte le democrazie occidentali, per una sua caratteristica fondamentale fra le altre, espressione di equilibrio, di un sistema di contrappesi che le ha garantito la sua permanenza e la sua messa in opera. Soprattutto la nostra Carta costituzionale si caratterizza per la sua elasticità, cioè per la sua capacità

dice chiaramente che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questa è la grandezza della Costituzione italiana. I Costituenti hanno voluto consegnare un testo che non soltanto dicesse come si doveva gestire la democrazia nel momento in cui la Costituzione sarebbe entrata in vigore, ma hanno voluto anche fissare dei capisaldi immanenti, dicendo che anche se domani gli elettori impazzissero, anche se domani qualcuno pensasse di potere sovvertire l'ordine delle cose, i limiti della Costituzione sono immanenti e nessuno li potrà sovvertire, perché se si tentasse una riforma costituzionale che ne alterasse la natura natura la Corte costituzionale avrebbe in sé i modi per combattere questo germe, potrebbe da sola già contrastare il germe antidemocratico, il germe del totalitarismo. In questo risiede la grandezza della nostra Carta costituzionale, che però non è una Carta alla quale noi dobbiamo guardare con il timore di apportarvi una riforma, di migliorarla, di prendere atto di quelli che sono diventati nel tempo i suoi limiti e di intervenire per farla diventare sempre più aderente al suo scopo, sempre più uno strumento efficace. La nostra forma parlamentare si fonda sul bicameralismo perfetto. All'epoca, quando è stata promulgata la nostra Costituzione, era la soluzione perfetta, ideale perfetta, ideale per i fatti storici dai quali si usciva. Due Camere dovevano pronunciarsi sui testi di legge e solo all'esito di una pronuncia uguale sullo stesso testo, senza modifiche, quel testo sarebbe potuto diventare legge. Essa prevedeva però anche una forma semplificata di legislazione, nel senso che prevedeva il decreto legislativo e il decreto-legge, che sono strumenti tuttora vigenti. Nulla è cambiato dall'epoca. Il decreto-legge era una forma di decretazione d'urgenza che i Padri costituenti immaginavano

sempre fatta salva poi l'approvazione da parte delle Camere. Nel tempo, però, che cosa è successo? Il bicameralismo perfetto si è in qualche modo arenato, ha cominciato a mostrare la fatica di questo doppio passaggio che talvolta diventa triplo e talvolta anche quadruplo, perché i tempi della discussione, i tempi degli uffici, i tempi del passaggio hanno cominciato a ingolfare la macchina, il procedimento. E allora, come sempre succede, la soluzione è stata quella di forzare il dettato normativo e fare sempre più spesso ricorso alla decretazione d'urgenza per arrivare all'obiettivo, che è quello di promulgare le leggi, di adottare i provvedimenti necessari per dare le risposte ai cittadini. I parlamentari, infatti, svolgono la funzione legislativa per dare le leggi ai cittadini che forniscono gli strumenti del vivere civile, perché il vivere civile è fatto dalle leggi, non c'è dubbio. Questi sono gli strumenti,

nei fatti era diventata una difficoltà del bicameralismo perfetto a dare risposte tempestivamente. Allora, se questa è la genesi del problema, non si può non dire che il bicameralismo perfetto non debba andare incontro a una modifica, un ripensamento, un miglioramento, certo non a uno snaturamento, certo non all'abolizione della forma repubblicana. Questo non lo pensa nessuno e non è neanche in questo disegno di legge.

a giurare nuovamente per assumere il secondo mandato, con veemenza ha richiamato il Parlamento alle sue responsabilità e l'ha invitato a procedere in tempi rapidi a una riforma costituzionale attesa attesa e necessaria. Eppure sono passati undici anni e di questa riforma non c'è traccia, se non nei tentativi che vengono portati avanti, fra i quali c'è anche questo disegno di legge di riforma costituzionale.

di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, perché la riteniamo la migliore espressione per dare attuazione all'articolo 1 della Costituzione, secondo cui la sovranità appartiene al popolo. E come meglio di così, di un'elezione diretta, il popolo potrebbe esprimere ed esercitare questa sovranità? Credo che sia proprio la sublimazione della *ratio* di questo articolo: un'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, al quale gli italiani, eleggendolo, danno il potere, ma anche la responsabilità, di attuare quel programma di Governo in forza del quale lo hanno votato.

Abbiamo tentato di dirlo in Commissione, dove più volte ho fatto degli interventi, e lo abbiamo ribadito anche nella discussione sulla questione pregiudiziale. Il primo è un richiamo formale, all'interno dello stesso disegno di riforma costituzionale, a una legge elettorale di cui non conosciamo il contenuto. Possiamo dire mai che vogliamo eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri senza sapere come lo eleggeremo? Se c'è un premio di maggioranza? Se è previsto un ballottaggio? Come e se si verificherà un effetto di trascinamento tra le liste dei partiti che eleggono il Presidente del Consiglio dei ministri e in che misura sarà garantita la rappresentatività dentro il Parlamento delle liste che formeranno l'opposizione? Sono troppe le domande e i quesiti che restano senza risposta e che ci costringono a continuare a dirle, signora Ministro, che votare questo disegno di legge sarebbe un atto fideistico alla cieca. Non ci sentiamo di continuare questo percorso, perché sono troppi i quesiti irrisolti e perché è necessario che sulla legge elettorale sia fatta un'opportuna fatta un'opportuna e approfondita riflessione, proprio perché la legge elettorale è quella che poi determina la composizione del Parlamento e dalla legge elettorale passa la stabilità di un Parlamento. Eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri è senza dubbio una forma di esercizio altissima della democrazia diretta, ma la stabilità di un Parlamento e di un Governo passa certamente dalla formazione di questo Parlamento e dalla sua legge elettorale. Non sono d'accordo - mi avvio alla conclusione, signora Presidente - con chi dice che la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio dei ministri, determinando lo scioglimento delle Camere e quindi la fine di quel Governo, metterebbe i parlamentari sotto il ricatto del Presidente del Consiglio dei ministri. Semmai io la vedo esattamente al contrario: è il Presidente del Consiglio dei ministri che a quel punto sa di dover stare attento ai rapporti con i parlamentari, sa di essere chiamato alle sue responsabilità, sa che, se non sarà data attuazione al suo programma di Governo, i parlamentari avranno l'arma migliore e sicuramente più convincente per tenerlo in coerenza al suo programma di Governo. Ma certamente, affinché quest'arma sia efficace, ci vuole un senso di responsabilità da parte dei parlamentari, che a quel punto non potranno neanche più pensare di fare ricorso alle strategie parlamentari o alla formazione di nuovi Governi tecnici per perpetuare la loro esistenza in vita. Sia chiaro: se c'è una cosa che demotiva totalmente l'elettore, che lo spinge a non presentarsi alle urne e che lo fa guardare con crescente distacco alle dinamiche della politica, è la formazione dei Governi tecnici, il ricorrere ai Governi tecnici, cioè lo snaturare dei Governi che si susseguono dopo quello che viene eletto e che talvolta arrivano a composizioni di maggioranza che sono completamente distanti da quelle iniziali e talvolta, ancor di più e peggio, arrivano ad adottare provvedimenti che non c'entravano assolutamente nulla con il programma elettorale originario. il cittadino viene responsabilizzato e gli viene data la possibilità di scegliere e di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri e i parlamentari allo stesso modo. In maniera quasi corrispondente, i cittadini vengono responsabilizzati a dire che il Governo dipende dalle loro scelte e nel momento in cui queste scelte sono compiute con responsabilità, se quel Presidente del Consiglio dei ministri non aderisce più al disegno, viene proposta una mozione di sfiducia. Questa ritengo che sia la forma più democratica di esercizio del potere. iscritta a parlare la senatrice Floridia oggi più che mai in quest'Aula sento forte sulle mie spalle la responsabilità del compito che sono stata chiamata a svolgere, anche per salvaguardare la tenuta democratica e pluralistica del nostro Paese, sancita dalla nostra meravigliosa Costituzione, tenuta che è messa a dura prova dai tentativi costituzionalmente distruttivi del Governo Meloni, per di più in un periodo storico di globale fragilità che di tutto ha bisogno, ma non certamente di divisione e dello smantellamento di principi cardine che hanno guidato la nostra democrazia fino ai giorni giorni nostri. Al termine dell'asfissiante propaganda politica con cui voi della maggioranza avete monopolizzato il dibattito pubblico in questo primo anno e mezzo di legislatura, con un atteggiamento - lasciatemelo dire - di enorme superficialità e faciloneria rispetto alle vere priorità del Paese, siamo giunti a dover discutere in prima lettura di un progetto di riforma costituzionale pericoloso e pasticciato. È già stato detto, è già stato ripetuto e oggi sento anch'io il dovere di dirlo: è una riforma altamente lesiva dell'equilibrio democratico che le Madri e i Padri Costituenti di tutti i partiti avevano invece mirabilmente delineato nel 1948, con innegabile

non fanno altro che esautorare il Parlamento da qualsivoglia potere legislativo e decisorio, imbrigliandolo alle volontà e alla volubilità del Presidente del Consiglio di turno e della sua stretta cerchia di eletti, togliendo a cittadine e cittadini fondamentali diritti di partecipazione democratica e non sicuramente ampliandoli, come erroneamente volete far credere al Paese. Dietro questa riforma, confezionata con il pretesto di restituire centralità e potere ai cittadini, si persegue esattamente il contrario; si strozza, infatti la rappresentanza e il libero dibattito, si azzera la possibilità di un sano confronto politico. Parallelamente, questa riforma concede un enorme potere decisionale ad un'unica figura istituzionale, oscurando notevoli profili costituzionali garanti della nostra democrazia e del suo funzionamento. Anch'io qui mi riferisco alla vostra triste e irrispettosa decisione di ridurre il Presidente della Repubblica a mero notaio e ratificatore di scelte imposte da altri, togliendogli irresponsabilmente quella funzione cruciale di garante dell'ordine e dell'equilibrio costituzionale, vera e propria valvola di sicurezza nei momenti storicamente e istituzionalmente più delicati della vita repubblicana, chiamato all'importante funzione di vigilare sul rispetto dei principi democratici nel nostro Paese, per evitare derive antidemocratiche e autoritarie. Ammettiamolo che oggi ci troviamo a votare un progetto di riforma costituzionale acerbo. Nessuno dei presenti in quest'Aula ha perfettamente chiaro quali saranno i meccanismi per poterlo far funzionare funzionare e quale nuova forma avrà la legge elettorale. Com'è possibile un caos e una pressapochezza del genere? Portate pazienza, ma veramente non siamo qui a votare un regolamento condominiale. Inoltre, la vostra idea di governabilità, figurativamente attribuita al *leader* forte, a una specie di supereroe che nel vostro immaginario collettivo risolve da solo tutti i problemi, cozza non solo con la storia, ma anche con i principi democratici su cui si fonda la nostra Repubblica. La vostra idea di accentrare tutti i poteri in un'unica figura si scontra inoltre, in maniera evidente, anche con il funzionamento dell'autonomia differenziata, la quale, al contrario, intende accentrare in capo alle Regioni la competenza di diverse materie, come l'istruzione, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la sanità. Solo per fare un banale esempio, la sanità è già in capo alle Regioni e si trova già in profonda crisi guarda caso anche al Nord, considerato fiore all'occhiello del sistema sanitario. una contraddizione così evidente e così assurda che la dice lunga sulla mancanza di una visione condivisa all'interno del Governo Meloni e che di fatto apre le porte al caos: chi deciderà e farà cosa con l'autonomia e con il premierato? Con questo *modus operandi* in perfetto stile azzeccagarbugli da un anno e mezzo il Governo Meloni e voi della maggioranza state poi spostando l'attenzione dei cittadini dalla vostra palese difficoltà nell'affrontare seriamente e con metodo le vere questioni urgenti che stanno affliggendo il nostro Paese. Sicuramente non è prioritario approvare qui in Aula provvedimenti quali l'istituzione dei premi del maestro del *made in Italy* o del maestro dell'arte della cucina italiana. Ne cito solo due che nel loro piccolo avranno anche il loro senso e utilità, ma che ingolfano i nostri lavori in Commissione e in Aula, evidenziando la totale o a questo punto direi la voluta mancanza di priorità, di visione, di organicità e di prospettiva rispetto ai gravi problemi dell'Italia cui siamo chiamati a rispondere urgentemente. Così, in mancanza di una seria scala delle priorità da affrontare, vengono tagliate fuori dall'agenda di Governo questioni cruciali che continuiamo a ripetere da un anno e mezzo a questa parte, come la crisi climatica, che sta cambiando le nostre vite e sta mettendo in ginocchio l'economia, costringendoci a vivere in ambienti sempre più inquinati e nocivi per la nostra l'urgenza di mettere in sicurezza il nostro Paese dal dissesto idrogeologico; l'urgenza di garantire la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture portanti del nostro Paese (ponti, strade, ferrovie, fognature, rete idrica); vi è l'esigenza di traghettare il nostro sistema economico verso la decarbonizzazione e verso la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, per assicurare uno sviluppo ambientalmente, economicamente e socialmente sostenibile per le presenti e le future generazioni. all'essenziale rafforzamento del nostro sistema sanitario, in grave crisi in numerose Regioni della Penisola; alla necessità di introdurre misure per combattere il precariato e garantire la sicurezza dei lavoratori, restituendo loro valore e dignità; al bisogno di incrementare i fondi per la scuola, per l'università, per l'edilizia scolastica, per permettere ai cittadini e al Paese di avere gli strumenti necessari per cogliere le sfide del presente e del futuro. Potrei andare avanti, ma queste sono tutte questioni chiuse a chiave nel cassetto del Governo, nella consapevolezza che l'inazione politica sta già producendo danni incalcolabili a tutto il Paese. Voi della maggioranza, stranamente, state accelerando solo sulla riforma del premierato e dell'autonomia differenziata, senza peraltro avere una concreta consapevolezza di quali saranno gli effetti che queste riforme produrranno nel nostro ordinamento costituzionale. un vero salto nel buio che state chiedendo al Paese di fare proprio in questo momento storico flagellato anche dalle guerre; chiedete di fare un viaggio improvvisato verso un futuro senza coordinate ben chiare e definite. Purtroppo, neanche di fronte alle perplessità espresse dai più illustri costituzionalisti, che hanno affermato che si sarebbe potuto fare meglio, avete avuto ripensamenti. Lasciatemi dire allora che invece si può fare di meglio, che l'Italia si merita il meglio e che il meglio va pensato e attuato oggi. e attuato oggi. La leggerezza con la quale volete mettere mano alla struttura pressoché perfetta e bilanciata di una tra le Carte costituzionali più belle al mondo e il pressapochismo con cui la state bistrattando Auguro veramente, francamente, sinceramente al Governo Meloni, a lei, signora Ministra, e voi della maggioranza, di recuperare al più presto un po' di quella lucidità e lungimiranza che ha guidato così coraggiosamente le nostre Madri e i nostri Padri costituenti nella redazione della nostra Carta, che oggi costituisce la spina dorsale di tutto il nostro ordinamento costituzionale. Serve più umiltà, serve una visione d'insieme, un serio dialogo con le opposizioni; vanno messe in campo tutte le nostre risorse ed energie per evitare che la nostra Costituzione, il gioiello più prezioso che abbiamo ereditato dal nostro passato, venga irrecuperabilmente sfregiata. La Costituzione va rispettata e attuata, come ha sottolineato ieri anche la senatrice Liliana Segre, che qui ringrazio. Tornate sui vostri passi, fatelo per il nostro Paese, c'è ancora tempo, c'è ancora domani.

con questo provvedimento penso che siamo arrivati al terzo capitolo della nuova saga, il grande inganno o l'arte dell'inganno.

che venivano utilizzate e vengono ancora oggi utilizzate dagli *hacker* per poter penetrare le reti, tecniche di manipolazione e di inganno, espedienti che servono per usare e carpire la buona fede delle persone e, con la loro ingenuità, poter recare danni. Ebbene, Presidente, come non definire inganno l'atto di questo Governo, di questa maggioranza, che inganna e lusinga i cittadini dicendo loro di votare

Tra l'altro, Presidente, è un sistema facilmente replicabile in altre competizioni elettorali e quindi rende ancora più oscuro e meno trasparente il processo. Mi permetto di rivolgermi tramite lei, Presidente, al collega Della Porta, ricordando che

regaleremo per i prossimi cinque anni 650 milioni al presidente Rama in Albania per gestire 2.000 immigrati l'anno. Per me è ingannevole anche dire agli italiani che li aiuteremo, quando poi magari non si tassano gli extraprofitti delle banche e gli italiani continuano a pagare il doppio del mutuo e aumenta l'IVA sui pannolini. Esistono elementi per dire questa maggioranza prova sempre di più a ingannare i cittadini e non certo a rendere più trasparente il sistema. La fredda cronaca racconta che a colpi di piccone la maggioranza prova continuamente a smantellare l'apparato istituzionale che regge la nostra Repubblica con un misero testo, con pochi articoli, oltretutto semplicemente abbozzati e incompleti. Per l'ennesima volta, la stessa destra tenta di modificare e riscrivere la nostra Carta costituzionale. Signor Presidente, prima di ogni altra considerazione in merito, devo dire che il MoVimento 5 Stelle difenderà ancora, convintamente e sempre di più la legge delle leggi, che la maggioranza continua a utilizzare sempre più come carta straccia e se non dovesse riuscirci per i numeri, la forza politica a cui appartengo lo farà con tutti gli strumenti democratici, insieme ai cittadini, per i cittadini e con i cittadini. È ormai palese a tutti che questa forma di premierato è semplicemente un baratto disonorevole tra Lega e Fratelli d'Italia, tra l'autonomia differenziata e il premierato. La spaccatura dell'Italia a danno non solo del Sud e delle aree interne, in cambio della concentrazione del potere nelle mani del Presidente del Consiglio, ritengo che sia una becera propaganda. Due riforme che viaggiano sullo stesso binario, quello dell'antidemocrazia, una vera e propria umiliazione del Parlamento, depauperandolo dall'alto con il premierato e dal basso con l'autonomia. Con questa riforma viene del tutto inficiata la separazione dei poteri: il Parlamento, quale organo sovrano della Repubblica, diventerebbe organo in pugno a una sola persona, la Giorgia di turno. Ingannevole è affermare che trattasi di una legge che conferirebbe ai cittadini maggiori poteri. La verità è che il diritto dei cittadini si ridurrebbe all'esercizio del mero voto una sola volta ogni cinque anni, senza avere alcuna rappresentanza nelle istituzioni tramite i parlamentari. Altrettanto ingannevole è dire che i poteri del Quirinale non verranno colpiti. State organizzando in essere una vera e propria delegittimazione dello stesso, una riforma che prevede la modifica di diversi articoli della nostra Costituzione. L'attuale contenuto dell'articolo 92, in cui è stabilito che il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri e che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri, verrebbe per opera della riforma costituzionale in esame riformulato, prevedendo l'elezione del Presidente del Consiglio a suffragio universale e diretto per cinque anni e per non più di due legislature consecutive che diventerebbero tre in caso di una contingenza esclusiva ovvero nel caso in cui il Presidente del Consiglio avesse ricoperto l'incarico di Primo Ministro per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Sempre per opera della riforma, le elezioni della Camera e del Presidente del Consiglio avrebbero luogo contestualmente e il Presidente del Consiglio verrebbe eletto nella Camera in cui ha presentato la candidatura. Una legge elettorale ancora da approvare - e questo non dice poco sulla trasparenza, ma molto sulla grossolanità di questa riforma - regolerebbe il sistema per le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste dei candidati collegati al Presidente del Consiglio. Questa destra, però, Presidente, non solo pensa male, ma pensa anche poco non considerando i vari scenari possibili. Il sistema delineato, infatti, presenta un grosso *vulnus* al suo interno. Vi spiego: scrivendo la legge elettorale dovrà essere designata una soglia minima di voti affinché scatti il premio dei seggi, soglia indispensabile per la maggioranza parlamentare. Se però il vincitore delle elezioni non dovesse superare la soglia indicata, cosa accadrebbe? Potrebbe verificarsi il ballottaggio tra i due vincitori, potrebbe non scattare il premio di maggioranza per far valere ancora la legge elettorale precedente, quindi il *Premier* non sarebbe eletto direttamente ma scelto e votato in Parlamento e, infine, si potrebbe votare all'infinito perché non si raggiungerebbe e supererebbe quella soglia elettorale, situazione che costituirebbe certamente per l'instabilità politica esattamente il male che la maggioranza avrebbe voluto curare con la riforma, ovviamente senza riuscirci. Una riforma, quella studiata - per modo di dire - lontano dalla stabilità e dal rapporto fiduciario tra elettori e Istituzioni. Ancora: con tale riforma, dove finirebbe la sovranità popolare sancita dalla nostra Costituzione? Rimettere con queste modalità superficiali e zotiche all'elezione popolare diretta la scelta del Primo Ministro è pericoloso ed è una faccenda insidiosa per le aspettative di partecipazione democratica; una soluzione inedita e ingannevole. Ricordiamo che esiste solo uno Stato nel panorama internazionale dove il premierato, inteso come elezione diretta del *Premier*, è diventato realtà Israele. L'esperienza è iniziata nel 1992, ma è finita male nel 2002. Persino nel modello Westminster, che pure costituisce il riferimento ideale del cosiddetto premierato, la continuità in coerenza tra voto popolare, maggioranza parlamentare e *premiership*, non è il risvolto di un vincolo normativo che guida il registro e il voto e vi conforma l'ordine di governo, ma è un esito di prassi costituzionali e soprattutto del piazzamento della competizione politica in uno spirito popolare, nei collegi uninominali tra i due partiti maggiori. Il Capo del Governo verrebbe eletto privando il Parlamento della sua funzione sostanziale, quella di rappresentare in modo compiuto il popolo sovrano, esprimere l'indirizzo politico scaturito dalle urne e determinato dei fatti, dare voce e peso anche alle minoranze. Prevede inoltre un Primo Ministro elettivo, un Parlamento gregario e un Presidente della Repubblica dimezzato. La riforma contempla inoltre una drastica riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica, rendendo fortissimo il Capo del Governo, con una concreta ed effettiva impossibilità del Presidente della Repubblica di opporsi a sua volta in sede di scelta. Il Presidente della Repubblica conferirebbe al Presidente del Consiglio l'incarico di formare il Governo e nominerebbe e revocherebbe, su proposta di questo, i Ministri. Utilizzando le parole di un costituzionalista, la nomina dei Ministri scelti dal Presidente del Consiglio diventerebbe per il Capo dello Stato un atto praticamente dovuto. Il Presidente della Repubblica si troverebbe di fronte a un Presidente del Consiglio con una legittimazione popolare e, quindi, molto più forte della sua e difficilmente potrebbe rifiutarsi di nominare un Ministro proposto dal Capo del Governo. Leggendo il testo della riforma, che prevede anche ulteriori modifiche della Carta costituzionale, è evidente l'accanimento nel voler superare in un modo o nell'altro e definitivamente la Costituzione uscita dalla Resistenza. Questa volta il bersaglio scelto è la democrazia. Deve Deve esservi chiaro che la sovranità appartiene al popolo, non allo Stato e non alla Nazione; l'apparato né è solo lo strumento. Lo Stato repubblicano è fondato unicamente sul consenso popolare. Farò mie le parole del presidente Conte: non potrà mai definirsi sovranità la possibilità di andare in cabina a limitarsi a votare ogni cinque anni un *Premier* dotato di pieni poteri, per di più in un Paese come il nostro, dove spesso l'astensionismo è protagonista; un *Premier* che quindi rappresenterebbe solo una minoranza dei cittadini e che inoltre imporrebbe di tutto e senza limiti anche al Quirinale, al Parlamento e a tutta la filiera delle autorità di garanzia che verrebbe eletta da un Parlamento sotto ricatto. La sovranità che appartiene solo al popolo è un'altra cosa: è partecipazione democratica in tutte le sue forme. *(Applausi)*.

n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

ai risultati che un provvedimento di tal genere ha portato. Freddi numeri ci mettono di fronte a una realtà incontrovertibile e ci danno la possibilità in questo momento di poter prendere una decisione che reputiamo giusta,

i conti in salvo, in modo da poter liberamente investire sul futuro della nostra Italia, prendendo delle decisioni libere e non condizionate da un peso enorme che un provvedimento di tal genere, nel caso in cui avessimo lasciato correre, avrebbe portato in seguito. Si tratta di un provvedimento

all'evoluzione del nostro patrimonio edilizio italiano, ma è altrettanto vero che lo si farà con coscienza e tenendo ben presente i conti e le possibilità che abbiamo di poter portare avanti provvedimenti di siffatto genere. di siffatto genere. Devo dire effettivamente che il lavoro di Commissione è stato ottimo, portato avanti dal presidente Garavaglia

per portare risultati molto più concreti e nelle possibilità di questo Stato. E dico ciò anche perché quanto generato dai crediti in genere

poneva naturalmente e inevitabilmente davanti a un bivio che abbiamo superato nella nuova formulazione, migliorata attraverso il lavoro di Commissione svolto - come dicevo precedentemente - in modo tale da poter continuare su questo percorso, ma mantenendo i

sarà possibile, attraverso un emendamento presentato dal Governo stesso, intervenire anche su aree diverse rispetto a quelle precedentemente identificate. identificate. Si parla di sismi, ma anche di alluvioni; si fa riferimento all'Emilia Romagna, si fa riferimento al Molise, si fa riferimento a Ischia, si fa riferimento a Catania, si fa riferimento al cosiddetto Calabria-Basilicata e, quindi, alla possibilità di continuare

Signor Presidente, ieri si è concluso il teatrino che avete creato in Commissione. Come sempre Forza Italia ha fatto il passo del gambero: prima ha fatto vedere che era dalla parte delle imprese e poi ha accettato la decisione del Ministro, che si è svegliato tutto a un tratto e ha capito che questo provvedimento per lui diventava insostenibile, dopo averlo gestito per tre anni e mezzo. L'ha capito negli ultimi giorni. negli ultimi giorni. Sono tre anni e mezzo che Giorgetti gestisce il superbonus e adesso ci dice che è troppo costoso. In Commissione anche Italia Viva ha dimostrato di essere contro le imprese dell'edilizia, sostenendo dell'ENEA e vedere i dati di quanto la misura è costata mese per mese.

al panico causato dal Ministro e all'incapacità di gestire questa misura, che - lo ricordo - era emergenziale. Il 110 era una misura che andava gestita in maniera corretta; serviva l'impulso e il 110, questa percentuale così alta, ha fatto il suo lavoro: ha fatto crescere l'economia,

nei primi anni della sua vita e che poi è stata distrutta da questo Governo, che non è stato in grado di trasformare una misura emergenziale, pensata per risolvere la crisi economica causata dalla pandemia, in una misura strutturale, con un *décalage* e con delle percentuali più basse. Non è stato capace di fare quello che avete fatto per il reddito di cittadinanza: ne avete parlato per mesi e, in pochissimi mesi, avete tolto il reddito di cittadinanza, risparmiando 900 milioni. Adesso l'assegno di inclusione, più i costi, costa 7 miliardi e 100 milioni allo Stato, 900 milioni in meno del reddito di cittadinanza come era stato pensato dai Governi precedenti. Avete fatto un'operazione mediatica per risparmiare 900 milioni e non vi siete accorti, in un anno e mezzo, che il superbonus con il vostro Governo cresceva di 70 miliardi. Avete dimostrato una completa incapacità di fare un'analisi costi-benefici, di fare della pianificazione e degli scenari su questa misura, che era

è avanti rispetto alla nuova normativa europea sulle Case *green*. Però questo non glielo andate a dire; anzi, con il disegno di legge

viste? State mettendo i cittadini italiani davanti al fatto che dovranno autofinanziarsi tutti gli interventi di efficientamento energetico, perché state addirittura abbassando l'ecobonus dal 50 al 30 per cento, oppure vedranno la loro casa svalutata. Perché non andate a dire questo in campagna elettorale, il grandioso risultato che state ottenendo sulla pelle degli italiani? Quando c'era da tagliare ai poveri siete stati velocissimi, per risparmiare 900 milioni di euro. Il superbonus invece andava pensato

una volta insediati al Governo, trasformare questa misura con una percentuale dell'80-90 per cento, per le famiglie in difficoltà,

e non ci saranno nuove costruzioni. Dopo tutto questo, andate pure a fermare ogni possibilità di intervento di efficientamento energetico, nella direzione di quella che ormai, colleghi, non è più un'alternativa. I cambiamenti climatici sono reali e l'efficientamento energetico delle nostre case è necessario. È un qualcosa che dobbiamo affrontare e voi state facendo finta che i *target* che l'Unione europea ci chiede non esistano. Andate in Europa e non portate nulla. Invece di distruggere l'edilizia, le imprese e le famiglie italiane, andate a fare la voce grossa in Europa, chiedendo degli chiedendo degli incentivi e dei finanziamenti, un nuovo PNRR proprio sulle Case *green*. Andate lì a fare quello che il presidente Conte ha fatto, portando 209 miliardi *(Applausi)*. Voi ve ne siete venuti con 16 miliardi all'anno di

così diabolico il vostro progetto: volete depotenziare la magistratura per evitare i nuovi casi Liguria, che vi mettono in forte imparare imbarazzo. Volete pieni poteri e un controllo assoluto da parte del *Premier* con il premierato. Volete distruggere la sanità pubblica. Volete impoverire le Regioni del Sud con l'autonomia differenziata. Volete svalutare il patrimonio immobiliare, facendo passare addirittura la percentuale degli interventi di risanamento energetico dal 50 al 30 per cento. State distruggendo il Paese: è un combinato di leggi che metterà in ginocchio il Paese. Non pensavo che sareste potuti arrivare fino a questo livello. Oltre a non lanciare nulla come idea, tutti i vostri provvedimenti sono assolutamente pericolosi per questa Nazione. Non avete un progetto. Avete combattuto il reddito di cittadinanza per risparmiare delle delle briciole. Avete distrutto il superbonus che aveva creato + 12 per cento di PIL. Allora perché non parlate su TeleMeloni di quanto ha fatto entrare il superbonus? Però siete stati grandiosi a manipolare l'informazione pubblica. Non si è mai vista una protesta dei giornalisti come quella che c'è stata negli ultimi giorni sulla Rai. Rai. Il vostro obiettivo è quello di ingannare i cittadini, di dire che non riuscirà a fare le cose per colpa del superbonus e non dite la verità. *(Applausi)*. Non riuscite a fare le cose per la vostra incapacità, perché non siete stati in grado di pianificare

Purtroppo, l'unico difetto del superbonus è che da tre anni e mezzo lo gestite voi. *(Applausi)*. Per colpa vostra abbiamo perso un'opportunità grandiosa: quella di un grandissimo volano per l'economia, per far ripartire le imprese e gli investimenti in un progetto di medio-lungo periodo. Bravissimi! *(Applausi)*. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Signor Presidente, con questo provvedimento una promessa l'abbiamo mantenuta, che è quella della *sugar tax*. La tassa sulle bevande zuccherate è stata rinviata e, salvi ulteriori rinvii, che siamo fiduciosi di verificare nel prosieguo di questa annata, entrerà in vigore a partire dal luglio 2025 e non dal 1° luglio 2024, com'era previsto; insieme alla *plastic tax*, che è stata rinviata al 2026, rappresenta un balzello vessatorio e pericoloso per il mantenimento e lo sviluppo di molte imprese e di molti lavoratori italiani. Ieri la 6a Commissione del Senato, presieduta dal senatore Garavaglia, che ringrazio perché ho avuto modo di constatare la serietà e anche l'attenzione con cui ha condotto i lavori, è andata incontro alle richieste di molti parlamentari di categoria e ha approvato il nostro emendamento che prevede il rinvio di un anno, con una modifica introdotta nel decreto-legge oggi all'esame Abbiamo così confermato l'orientamento, più volte manifestato anche da questo Governo, di voler intervenire a sostegno delle aziende, del lavoro e delle fasce più deboli della popolazione. Tutto questo avviene a fronte di una situazione economica estremamente complessa, ulteriormente aggravata dalla difficilissima congiuntura internazionale. Ciononostante, in questi mesi abbiamo sempre cercato, per quanto possibile, di ascoltare le parti sociali, le categorie produttive e anche le associazioni sindacali e di recepirne le istanze. Due sono gli aspetti che più degli altri pesano oggi sull'economia del nostro Paese: gli effetti dell'inflazione e del carovita in generale che, sebbene in timida discesa, continuano a incidere negativamente sul potere d'acquisto delle famiglie, e le ulteriori incertezze generate dallo scoppio del nuovo conflitto in Medio Oriente. evidente che questa imposta avrebbe avuto un impatto forte sul settore delle bibite e sui consumatori e, di conseguenza, sull'economia del nostro Paese. Le ricadute della tassa, seppur ridotta, sul settore delle bevande analcoliche sarebbero infatti state molto gravi. A farne le spese in primo luogo sono il comparto, che conta circa 100 stabilimenti in Italia, tra multinazionali radicate sul territorio e piccole e medie imprese, per un totale di oltre 84.000 occupati e un valore di mercato di oltre 5 miliardi di euro, con un valore complessivo di esportazioni superiore ai 420 milioni di euro nello scorso anno. Quali potrebbero essere le conseguenze dell'entrata in vigore di questa tassa? Intanto, secondo le stime di Nomisma, la nuova imposta sulla produzione genererebbe un aumento del 28 per cento della pressione fiscale su un litro di bevanda alcolica, con una conseguente riduzione del 12 per cento degli investimenti in Italia e l'indebolimento della filiera del *made in Italy*. Le conseguenze sarebbero quindi una contrazione del mercato nel primo biennio in Italia del 16 per cento e, quindi, l'incertezza da parte delle aziende e l'impossibilità di fare una programmazione economica seria in ambito aziendale. I posti di lavoro a rischio sarebbero oltre 5.000 e ci sarebbe comunque un freno agli investimenti. Dal punto di vista della burocrazia, si avrebbero ulteriori 70 procedure da adempiere. Ieri si è quindi scelto di votare convintamente lo slittamento al 1° luglio 2025, al fine di non introdurre questa nuova forma di prelievo fiscale in un momento economico - come ho già detto - così complesso. Questo perché noi vogliamo - come sappiamo bene - una politica che ascolta le ragioni del tessuto imprenditoriale e produttivo e non vuole decimare il sistema che già fatica a reggersi in piedi. Ricordo che i consumi nazionali di bevande zuccherate son già in calo costante da dieci anni. La *sugar tax* colpirebbe inoltre anche tante piccole e medie imprese italiane, rischiando di affossare per sempre alcuni marchi storici della nostra tradizione; senza contare che l'applicazione di una tassa sulle bevande zuccherate in Italia, che graverebbe sulle bibite gassate e non, potrebbe attivare un nuovo pericoloso processo inflattivo sui beni di consumo e, di conseguenza, danneggiare le nostre esportazioni in tutto il mondo. Questo - lo dico soprattutto a quest'Assemblea - alla vigilia di scadenze importantissime come il rinnovo del Parlamento europeo, dove è già forte la pressione a favore dell'applicazione di tasse non solo sulle bevande zuccherate, ma anche sulle bevande alcoliche e su tutti i prodotti ricchi di sale, grassi o zuccheri, cioè i nostri vini, i nostri formaggi, i nostri salumi e tutti i principali prodotti del *made in Italy*. È in atto una vera e propria battaglia contro di noi alla quale noi diciamo no, perché questo per noi non va assolutamente bene. Vogliamo difendere la nostra economia, il nostro cibo, la nostra enogastronomia. Dobbiamo quindi immaginare che l'applicazione di una tassa sui generi alimentari in Italia potrebbe anche dare nuova linfa ai fautori del Nutri-score e di altre misure discriminatorie verso il *made in Italy*. Ricordo poi che l'attuale Governo è sempre stato contrario, anche in ambito internazionale, a misure che attribuissero a un singolo alimento e a un singolo ingrediente la responsabilità dell'aumento dell'obesità. le aziende italiane hanno già raggiunto risultati significativi in termini di riduzione di calorie e di zucchero, superiori al 41 questo senza tasse ma investendo soprattutto in innovazione, nella capacità di produrre un cibo sano e salubre. È cruciale riconoscere che il problema non è nello zucchero, di per sé. Addirittura negli otto Paesi europei in cui la tassa è stata introdotta l'obesità - secondo dati certi - è aumentata, ma il contesto del consumo all'interno di uno stile di vita complessivo è fondamentale. L'obesità è una patologia multifattoriale che può essere combattuta efficacemente non con l'introduzione di tasse punitive sui singoli ingredienti, ma solo attraverso l'educazione alimentare, un'informazione efficace e la promozione di stili di vita sani. E allora cosa c'è di meglio della dieta mediterranea? Valorizziamo la nostra dieta mediterranea, questo è fondamentale. Se l'obiettivo della misura è migliorare la salute pubblica, allora lo scopo da ricercare è quello di incentivare il diffondersi, a partire dalla cultura tra i giovani, della dieta mediterranea, che è provato che favorisce benessere fisico e longevità. benessere fisico e longevità. Serve cioè, al nostro parere, un approccio più complesso che non si limiti a misure punitive, ma che fornisca ai cittadini gli strumenti necessari per compiere scelte informate sui cibi. Con una tassa sulle bevande zuccherate, si rischia solo di aumentare i costi, spingendo le persone verso mercati alternativi con prodotti anche più costosi, finendo per danneggiare un settore economicamente fondamentale, ma dal punto di vista della salute non giova a nessuno. Per tali motivi, su questo abbiamo investito con un nostro emendamento, in cui abbiamo creduto, e ringrazio la Commissione per averlo accolto. Al di là delle polemiche che ci sono state da parte di alcuni Gruppi di maggioranza che si fanno fautori, ma poi non l'hanno votato, per noi è fondamentale il risultato ottenuto. *(Applausi)*.

il *premier* slovacco Robert Fico è stato oggetto di un attentato con arma da fuoco. Purtroppo, la campagna elettorale nell'Unione europea si sta dimostrando particolarmente complicata dopo gli attentati che nelle scorse settimane hanno coinvolto anche esponenti della mia famiglia politica, dell'SPD. quindi massima solidarietà oggi al *premier* slovacco Robert Fico, immaginando di interpretare anche il sentimento dell'Assemblea.

le regole parlamentari calpestate e piegate agli interessi di parte della maggioranza; un *blitz*, per fortuna, che il presidente La Russa ha voluto stoppare. Resta un precedente gravissimo il tentativo di modifica delle regole per imporre con la forza dei numeri una norma retroattiva che colpisce le aziende e rompe unilateralmente il patto con quei cittadini che si erano fidati dello Stato. Questa maggioranza si sta caratterizzando per una protervia e un mancato rispetto delle regole che inquietano e dovrebbero far riflettere. Non è la prima volta che accade sul salario minimo. Ad esempio, nell'altro ramo del Parlamento avete provveduto a far ripetere un voto quando il Governo era andato sotto. I limiti e le divisioni politiche della maggioranza vengono superati con un aggiramento delle regole del Parlamento, come se il lavoro della Commissione andasse bene solo quando certifica la volontà del principale partito. Quando così non è, si procede per strappi e forzature, mettendo in campo un vero e proprio attacco all'autonomia e alle prerogative del Parlamento. Ieri è andata in scena una maggioranza provvisoria e rabberciata, più simile a quella di un Governo in crisi che a quella di un Governo che dice di voler durare per cinque anni. Ma la forzatura delle regole non cancella il nodo politico. Nella maggioranza si è consumato uno scontro all'arma bianca tra le forze politiche; uno scontro che si è concluso non con la mediazione politica, ma con l'umiliazione di una delle forze della maggioranza. Dopo quello che è accaduto ieri, in che modo i colleghi di Forza Italia, che non vedo in Aula e forse ne hanno qualche ragione, possono votare questo provvedimento? Davvero, è un fatto non di merito, ma di metodo e di rispetto politico. Se una cosa del genere fosse successa nel centrosinistra, cari colleghi, non oso immaginare cosa avreste detto e avreste avuto ragione. Il punto - spero ve ne rendiate conto tutti è che questo è quello che succede in un Parlamento sottomesso al Governo ed è quella che diventerà la regola con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Se poi andiamo nel merito, non basta dire oggi che i *bonus* edilizi vanno fermati per scongiurare una voragine nei conti pubblici. Non basta, perché questa sensibilità non l'avete avuta durante il Governo Draghi, quando chiedevate addirittura di rendere strutturali le misure. Poi, voglio ricordare che siete al Governo da un anno e mezzo: perché non siete intervenuti prima? Perché avete sprecato tutto questo tempo per prorogare, da un lato, e per introdurre inutili complicazioni, dall'altro? Introdurre norme retroattive significa fare carta straccia di uno dei principali principi costitutivi del patto tra Stato e cittadini. È un danno enorme per i cittadini e le imprese, un colpo inferto alla credibilità dello Stato e delle istituzioni che dà fiato all'antipolitica. Soprattutto, è l'esatto contrario di uno Stato chiaro con i propri cittadini e con quelle imprese che, da tempo, non fanno altro che chiedere regole certe e stabili per gestire al meglio l'uscita dal *bonus* 110 e per la programmazione delle proprie attività negli anni a venire. venire. Il tema vero che questo Governo ancora non affronta è di offrire un orizzonte normativo e temporale certo per le imprese e le famiglie; disciplinare, cioè, l'intera materia dei *bonus* edilizi, che - va sottolineato - sono stati un importante stimolo per l'emersione fiscale, per la fuoriuscita dal lavoro nero di migliaia di lavoratori. lavoratori. Non dobbiamo dimenticare che le detrazioni fiscali edilizie sono nate in passato con l'obiettivo primario di fare emergere il lavoro nero. Poi, nel corso degli anni, hanno avuto anche un ruolo anticongiunturale, successivamente finalizzato al risparmio energetico e all'adeguamento sismico. In questo contesto, la volontà del Governo Meloni di ridurre tutti gli incentivi al 30 per cento dal prossimo anno non causerà soltanto problemi economici ai cittadini e alle imprese del settore, ma potrebbe anche incentivare, dopo decenni, l'evasione fiscale e soprattutto la manodopera illegale. Senza controlli adeguati nei cantieri, che vanno promossi con risorse ad assunzioni, si rischiano nuove stragi, questa volta ampiamente annunciate. Da quando si è insediato questo Governo non vi è stata pace per il settore. Si è preferito intervenire in maniera estemporanea, volta per volta, puntando alla strozzatura della misura nel suo complesso e non alla revisione, che pure sarebbe stata opportuna per evitare le storture che oggettivamente ci sono state. Oggi persino l'ABI vi certifica, dati alla mano, che la retroattività della norma porterà effetti negativi per tutto il sistema delle imprese e del credito. La verità è che ci si muove in chiave ideologica, con un approccio maccartista e privo di visione. Chiunque sa che intervenire sul settore edile ha effetti anticiclici in economia e consente di affrontare periodi di crisi. Ricalibrare la misura sarebbe stata la cosa più ovvia, senza destabilizzarla e criminalizzarla. Mettere ordine era necessario, anche per evitare speculazioni sui costi dei materiali e anche sulla manodopera. Troppe imprese si sono improvvisate in ambiti delicatissimi per la sicurezza e così avete finito per buttare il bambino con l'acqua sporca, senza mettere in sicurezza la validità di uno strumento di grande rilevanza economica e sociale. Il superbonus ha generato più di 40 miliardi di entrate dirette e più di 30 di entrate indirette, creando quasi 300.000 nuovi posti di lavoro soltanto nel settore edile, che sono stati molti di più se si considera anche l'indotto; 3 miliardi di euro l'anno risparmiati in bolletta per chi vive in abitazioni riqualificate e di benefici ambientali, che si traducono in una notevole riduzione di CO2. Appare quindi evidente che questo *bonus* è stato demonizzato e manipolato dal Governo Meloni, senza prendere in considerazione gli effetti diversificati, spesso incrementali e interconnessi, che avranno benefici per anni. Noi in questi mesi abbiamo chiesto al Governo di attivarsi con urgenza, coinvolgendo tutti i soggetti interessati per individuare modalità e soluzioni definitive di acquisto sia dei crediti pregressi già nei cassetti fiscali, sia dei crediti che verranno maturati relativamente ai cantieri già in corso, di adoperarsi per dare attuazione alla piattaforma finanziaria per l'assorbimento dei crediti incagliati. Vi abbiamo chiesto, con emendamenti e atti di indirizzo nel corso del tempo, di adottare iniziative volte a superare definitivamente gli ostacoli che attualmente bloccano la circolazione dei crediti fiscali, anche mediante la possibilità per gli istituti bancari di usare le quote annuali dei crediti attraverso i modelli F24, con il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti o altre soluzioni per evitare il fallimento delle imprese. Non da ultimo vi avevamo chiesto l'impegno affinché fosse riconosciuta a Regioni ed enti locali la possibilità di assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali. tutte soluzioni alla portata che potevano essere benissimo condivise. Il vostro però è un approccio sempre alla ricerca di un nemico. Vi opponete al superbonus e, al tempo stesso, agitate la direttiva comunitaria come uno spauracchio, come se non sapeste che riqualificare il nostro patrimonio edilizio dovrebbe essere una priorità non perché lo chiede l'Europa, ma perché è interesse dei cittadini. Siete arrivati persino a mettere in dubbio questi strumenti nelle aree terremotate. L'efficientamento energetico dei nostri edifici è un tema che va affrontato e non solo perché adesso c'è una direttiva europea. Va affrontato perché c'è un tema complessivo di costi delle bollette e di qualità della vita che interessa soprattutto le fasce più deboli della nostra popolazione. Va affrontato perché, soprattutto nelle Regioni del Sud, l'edilizia rappresenta la prima voce economica. Un danno a questo settore significherebbe condannare il Mezzogiorno a una recessione economica. Voi però ancora non riuscite a fare tutto questo. Scrivete oggi un provvedimento tossico nelle modalità, nei contenuti e soprattutto negli effetti. La questione, oggettivamente, non poteva essere gestita in modo peggiore e a pagarne il prezzo, come sempre, saranno le famiglie e le imprese.

per un un'opera importante per salvare le vite delle persone. Mi riferisco in particolare ai residenti della Pianura Padana. Come sapete, le Regioni che si affacciano sulla Pianura Padana sono sotto procedura di infrazione UE di inquinamento delle polveri sottili e del biossido di azoto. Il problema però è che questo inquinamento causa ogni anno decine di migliaia di morti. Parlo dei dati della Lombardia: 15.000 persone muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento. Diversamente da quanto accade per un terremoto o per un'alluvione, sono morti invisibili. L'inquinamento è un *killer* invisibile, non si vede come agisce, ma purtroppo

In Lombardia le cause dell'inquinamento sono molteplici, ma in questo caso quello che ci interessa è il riscaldamento degli edifici, che è una delle cause principali, efficientamento, al di là del cambiamento climatico e delle case *green* che tanto non vi piacciono. Stiamo parlando di dati concreti. Le persone muoiono a causa dell'inquinamento. Una delle cause fondamentali dell'inquinamento è il riscaldamento degli edifici. L'intervento di efficientamento degli edifici riduce il fabbisogno energetico e dimezza le emissioni nocive, quindi salva vite umane. Ho chiesto che questo Governo investisse dei soldi per salvare la vita a coloro i quali lavorano per produrre il 50 per cento del PIL e che invece muoiono. In queste Regioni non sono tutti i nababbi; c'è gente che vive del proprio lavoro, che non riesce neanche a curarsi, perché ci sono le file per il servizio sanitario e non ha i soldi per pagarsi le cure mediche. La Lombardia, per esempio, è una delle Regioni più densamente abitate: ha 10 milioni di abitanti. Le edificazioni in Lombardia sono principalmente nelle zone periferiche delle grandi città e sono costruzioni che risalgono al *boom* economico Settanta), quindi sono tutte case a bassissime prestazioni energetiche. L'intervento che veniva chiesto al Governo era di investire qualche spicciolo per agevolare fiscalmente gli interventi di efficientamento energetico degli edifici al fine di salvare vite umane, perché queste sono morti evitabili. Se il Governo si impegnasse, non morirebbero così tante persone. Mi è stato però risposto di no

Qual è l'ordine delle priorità di questo Governo? Possiamo dire ai cittadini padani che possono morire, perché dobbiamo sovvenzionare una guerra? L'ordine di priorità mi sembra assurdo. Se si vuole, i soldi si trovano, si sa. Abbiamo gli extraprofitti delle banche e delle stesse imprese militari, ma non si sono voluti trovare i soldi per finanziare queste che non sono altro che opere meritevoli. Lo ribadisco: c'è una grossa responsabilità di questo Governo perché queste sono morti evitabili. Possiamo dire ai cittadini della Pianura padana che il Governo ha deciso di mandarli indirettamente al fronte.

con tanti provvedimenti. Soprattutto anche l'altra manovra del PNRR siete riusciti a trasformarla nel piano dei ritardi e dei rinvii. Queste erano le due note positive che vi abbiamo lasciato come Governo

Avete fermato la produzione economica di questo Paese: la produzione dello sviluppo industriale è praticamente stagnante da un anno a questa parte. Avete tolto tutte le protezioni

Tutto questo tradendo promesse elettorali, dalle accise all'immigrazione, ma sempre con un pallino fisso che dirigeva i lavori, quello di distruggere ciò che era stato fatto dal Governo Conte, senza considerare nessuno dei danni collaterali che potevate causare a questo Paese. Il Paese è molto in difficoltà, come dicevo, ma adesso questi danni collaterali sono diventati propaganda. State continuamente attaccando i provvedimenti senza capire cosa succede intorno ad essi. Dovevate uscire con noi, ieri, in piazza, dove c'erano gli esodati del superbonus che protestavano e chiedevano di essere ascoltati. Nessuno li ha ascoltati. Il provvedimento è andato avanti per la sua strada. Non avete ascoltato gli esodati, non avete ascoltato le persone

nella passata legislatura, almeno alcuni di noi, e abbiamo visto tantissimi emendamenti di questa maggioranza sul provvedimento del superbonus. Tantissimi di questa maggioranza hanno sistemato case con il superbonus, senza guardare quello che, tra l'altro, è successo in Commissione.

che doveva affrontare questo tema, invece di prenderlo in maniera seria, è andato avanti per mesi e mesi a parlare di un buco di bilancio. Io lo vorrei vedere questo buco di bilancio. Continuiamo ad andare avanti avendo detto certe cose in passato per poi negarle in futuro. Continuare a ripetere menzogne non le fa diventare

ha ridotto i costi in bolletta; ha dato la possibilità alle famiglie di ristrutturare la propria casa, soprattutto alle persone che non potevano farlo. È stata una manovra che ha rialzato il PIL del nostro Paese, ha inserito liquidità all'interno delle tasche degli italiani ha spinto i consumatori, le categorie e gli imprenditori ad assumere e i commercianti a lavorare. Tale manovra ha dato la possibilità al nostro Paese di fare un passaggio dalle energie fossili a quelle rinnovabili. È ora di assumersi la responsabilità di facendo su questo tema e su questo argomento. Ammettetelo, secondo me veramente non avete capito nulla su questo tema, senza contare i paragoni, i temi e le discussioni che sono stati fatti su questo argomento, soprattutto in Commissione, dove solamente una persona ha capito come si doveva operare, cioè il Presidente, che ringrazio per come ci ha fatto lavorare perché ha cercato di tenere la barra dritta davanti a un provvedimento sul quale la maggior parte delle forze politiche della maggioranza non aveva la minima idea di come comportarsi. In Commissione il Ministro - lo dobbiamo dire - non è mai venuto in audizione realmente e quindi non ha mai parlato direttamente con i commissari. È stato trovato un *escamotage* dal Presidente per farci confrontare più e più volte. C'è stato un tira e molla sugli emendamenti. Non vedo gli amici di Forza Italia in Aula, quindi mi viene da pensare che qualcosa fino all'ultimo secondo sia successo,

E soprattutto la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e delle persone che ascoltano la politica è stata dimostrata tramite le dichiarazioni che continuamente sono state fatte intorno a questo provvedimento. Si è parlato di un provvedimento drogato e di

temi sensibilissimi, come le zone alluvionate e i territori che hanno subìto drammatici eventi climatici. Fare questo tipo di paragone su un tema e su una discussione così importanti è assolutamente fuori luogo e ci tengo a rimarcarlo,

che non sapranno come fare. Concludo, Presidente. Mi dispiace questo continuo racconto di Giorgia nel paese delle meraviglie, ma presto, secondo me, vi dovrete svegliare. State facendo dei gravi danni a questo Paese.

a discutere oggi è l'ennesimo provvedimento *omnibus*. Se n'è parlato in particolare per il superbonus, ma vi è contenuto di tutto. Quando sento i colleghi parlare dell'importanza di difendere le imprese, vorrei dire che sono importanti anche quelle che nel nostro Paese producono bevande

tutto ha bisogno questo Paese tranne che di nuove tasse. Ovviamente non voglio eludere l'argomento principale, quello che tutti hanno trattato, ossia il superbonus,

pensando in questo modo che, soltanto con il raddoppio della spesa, si sarebbe partiti e si sarebbe fatto un passo avanti per il recupero delle case. L'elemento che è sempre che è sempre stato in contraddizione rispetto a questa indicazione originaria è che la cessione del credito, cioè il fatto che il proprietario di casa, non pagando niente, otteneva subito una riqualificazione del 110 per cento, ha fatto moltiplicare la domanda (non è stato soltanto un semplice raddoppio), in modo tale che la spesa risultata immediatamente impazzita. Chi lo dice e chi lo scrive, in questi giorni, penso che non sia ascrivibile né alle file di Italia Viva, né alle file di altri partiti. È un economista di fama mondiale come Tito Boeri, che, nella sua rivista «Eco», fa la fotografia di un fallimento annunciato, dicendo che né il Governo Draghi, né la prima parte del Governo Meloni sono riusciti a dare una soluzione e che sicuramente questa ultima soluzione è altrettanto drastica e altrettanto ingiusta per le imprese che hanno rispettato la legge e si vedono oggi cambiare per l'ennesima volta le regole del gioco: tali imprese hanno rispettato leggi dello Stato evidentemente scritte male. scritte male. Quando sento i colleghi che dicono «dovevate ascoltare gli esodati fuori», rispondo che anche quando è stata scritta quella regola bisognava ascoltare per esempio l'ANCE, che aveva detto che non sarebbe andata a buon fine, scritta

Ora a me verrebbe da dire: durante gli anni di opposizione mi sono sentita le lezioni degli amici di Fratelli d'Italia, che dicevano che quando sarebbero andati al Governo avrebbero trovato la soluzione. Questa è la dimostrazione che non era così facile, come il vostro racconto ha detto per interi anni. Io ringrazio la collega Musolino per aver portato avanti i nostri due emendamenti, che cercavano di mettere una pezza su questa rivisitazione che riguardava la parte delle aree terremotate e le parti del terzo settore; sicuramente non come avrebbero voluto né le aree terremotate, né il terzo settore, ma rispetto a una troncatura tal quale, anche per loro si è avuta almeno una speranza e una prospettiva.

si vedranno completamente distrutti i loro *project financing*, l'impatto economico di quello che avevano previsto in buona fede, credendo nelle regole dello Stato. tutta la nostra solidarietà, mentre non va a chi ha scritto male le regole, a cui non succederà niente, perché purtroppo il merito in questo Paese non verrà mai premiato. Lo dico perché ormai sfornate decreti ogni settimana e quindi sicuramente dopo le elezioni bisognerà mettere mano a un provvedimento che salvaguardi le aziende che rischiano il il fallimento. Mi permetto anch'io, nella chiusura di questo breve intervento in discussione generale (poi ci saranno quelli del presidente Borghi durante la discussione sulla fiducia e della collega Musolino, che ha seguito il provvedimento nella dichiarazione di voto finale), di esprimere la solidarietà e l'augurio che che il *premier* slovacco Fico non sia in fin di vita e che l'attentato non porti all'ennesima vittima del fanatismo politico sulla strada dell'Unione europea. Mi collego quindi a quanto detto dal collega del Partito Democratico e mi auguro che ci sia un approfondimento, tra la fine della discussione generale e l'inizio delle dichiarazioni di voto,

ricordare a tutti noi che cosa è successo ieri. Credo che sia successo un fatto grave, che non si è consumato,

fatta presente al presidente La Russa, che ha impedito questo fatto, ma la cosa che davvero mi ha sconcertato è che a domanda - ed è testimone, perché l'ha detto in Aula

ma arrivare a depositare la proposta lo è ancora di più. Per fortuna ci siamo fermati, però questo è un *vulnus* dal punto di vista democratico. Seconda cosa: per dimostrare quante sono state le difficoltà (poi la maggioranza, ovviamente può dirla come vuole), noi oggi avremmo potuto essere qua a fare una discussione diversa, sempre

votato con la maggioranza, e grazie al voto su quell'emendamento di Italia Viva. Quindi il dato fondamentale è una crisi evidente della maggioranza, perché se non fossero successi questi fatti, oggi staremmo discutendo di un'altra cosa,

della norma mette a dura prova il rapporto tra lo Stato e il cittadino. La detraibilità

vorrei ricordare che già nel mio primo intervento dissi che la toppa era peggio del buco, perché non affrontava il tema che ci eravamo posti, però, c'è un dato

Quanto vale dal punto di vista del pagamento delle tasse, visto e considerato che non io, ma tutti i dati dicono che, tra diretti e indiretti, ha creato oltre

casa propria, calcola quanto spende e quanto ricava, quindi ognuno di noi se gestisce bene la propria famiglia fa queste operazioni. Ora, non si può dire che siamo sempre di fronte a un buco, guarda caso, quel buco non si va a chiuderlo magari chiedendo gli extraprofitti a chi aumenta il patrimonio e così via, ma si fa pagare ai cittadini e alle imprese, come in questo caso.

Se gli altri procedono su questa strada e noi continuiamo a pensare che bisogna frenare e ritardare, arriveremo sempre secondi; arriveremo sempre dopo e ne pagheremo le conseguenze. Ergo, forse il modo migliore di affrontare

ci racconta di un Governo allo sbaraglio e di una maggioranza litigiosa, perché i fatti dicono questo, con il Ministro e la sua forza politica che fanno proposte e un altro Ministro, nonché vice Presidente del Consiglio, che fa proposte diametralmente opposte e cerca di cancellare quello che ha appena chiesto il Ministro dell'economia. I fatti sono questi, poi le chiacchiere stanno a zero, direi. Vediamo una forza di maggioranza che si astiene in Commissione e che probabilmente era pronta a fare altrettanto in Aula e quindi per rimediare alle baruffe di maggioranza viene posta la fiducia anche laddove non se ne sentiva alcuna necessità, giusto per alzare ancora di più la media, ma vorrei far presente che eravate già il Governo dei *record* sulle fiducie, battendo persino Draghi in pandemia. Parliamo del merito, poi, del famigerato superbonus devastatore del Paese, sconquassatore di conti, creatore di voragini nel bilancio dello Stato, Stato, che non esistono in nessun documento pubblico, ma che voi sbandierate comunque indisturbati a reti unificate. Più che Più che di sconquasso dei conti pubblici o di superbonus, parliamo del superalibi al 110 per cento di questa maggioranza, che non fa che inanellare fallimenti uno dopo l'altro e che viene usato come arma di distrazione di massa per coprire una crescita che sta allo zero virgola nel 2023, *idem* nel 2024 e supera appena l'uno per cento nell'anno successivo. L'aumento del debito pubblico non è da ascriversi al super bonus, che avete contabilizzato nell'anno di generazione dei crediti, ma quanto più alla mancata crescita. Negli anni in cui il superbonus spingeva l'economia e la faceva crescere del 13 per cento, al di sopra di qualsiasi altro Paese dell'Unione europea (per la prima volta negli ultimi quarant'anni eravamo i primi nell'Unione europea e non di nuovo gli ultimi e fanalino di coda, come saremo in questi anni),

considerato anche che la propensione al risparmio degli italiani è al livello più basso dal 1995 e che gli stratosferici finanziamenti alla sanità pubblica - udite, udite - ammontano al 6,3 per cento del PIL, il livello più basso dal 2007. Un altro *record* del Governo Meloni è quello delle persone in povertà: mai così tante negli ultimi dieci anni. Meno male che ci avete detto che era colpa nostra, invece è l'Unione europea che addita la vostra misura di assegno di inclusione, che sostituisce il reddito di cittadinanza, come discriminatoria e causa della maggiore maggiore povertà nel nostro Paese. Un altro *record*: quattordici mesi consecutivi di calo della produzione industriale, e ci piacerebbe tanto sapere che fine ha fatto il decreto attuativo di Transizione 5.0. Un altro fallimento del Governo è quello del carrello tricolore, che fa crescere il carrello della spesa del 9,5 per cento nel 2023, addirittura più di quanto era salito nel 2024, anno di picco dell'inflazione. Ripeto: il dubbio che stiate sbagliando qualcosa non vi viene? Fatevelo venire qualche dubbio.

rispetto al 2022, però tassare gli extraprofitti era una vergogna. Poverini, magari dobbiamo dare loro qualcos'altro per dargli una mano, perché dieci miliardi di dividendi agli azionisti mi sembrano veramente una miseria che grida vendetta, in questo Paese dove abbiamo solo dieci milioni di poveri. Suvvia, che volete che siano soli dieci miliardi di utili? Davvero, non avete neanche un briciolo di vergogna, per quello che state facendo e per le bugie che raccontate sul superbonus. Ha detto bene, infatti, il senatore Magni prima. Parlate solo dei costi, che ogni giorno crescono vertiginosamente (Enea certifica 160 miliardi, voi parlate di 216, ma non si capisce bene dove li avete presi) e non dite mai che più di 100 miliardi sono tutti vostri, effetto delle norme scriteriate che avete varato da quando siete al Governo. Non parliamo poi del fatto che anche prima il caro illustre ministro Giorgetti si occupava di superbonus, perché era Ministro dello sviluppo economico durante il Governo Draghi. Che guardi a se stesso, quindi, e si metta uno specchio nello studio e nel suo ufficio, quando parla di disastri creati dal superbonus, perché una buona parte sono colpa sua e del malgoverno che lui ha fatto della misura, non noi. Noi, infatti, la misura l'avevamo ideata in maniera completamente diversa. Essa è stata cambiata da una ventina di norme successive rispetto a come l'aveva varata il Governo Conte II. quindi a Giorgetti per i disastri dell'economia: quelli fatti negli ultimi anni dal superbonus e quelli fatti dalla mancata visione di futuro del Paese che sta causando ancora oggi. Tolto questo, vi dimenticate sempre di dire invece quali sono stati gli incassi. Tutte le imprese lamentano infatti una pressione fiscale in questo Paese al 60 per cento, ma quando si parla dei ricavi del superbonus magicamente la pressione fiscale scende sotto il 20 per cento, perché quello è il ritorno che viene dichiarato

al 20 per cento di ipotetico ritorno. Ci sono inoltre i contributi che vanno a finire nelle casse dell'INPS per circa 700.000 lavoratori che senza il superbonus non ci sarebbero stati. Chissà come mai l'Agenzia delle entrate dichiara 140 140 miliardi di maggiori entrate fiscali nel nostro Paese nel triennio 2021-2023. Chissà da dove saranno piovuti mai! *(Applausi)*. Chissà qual è stato il motore che ha fatto entrare questi 140 miliardi quando il superbonus cubava intorno ai 70 miliardi. Parliamo addirittura di un motore che non ha fruttato il 50 per cento, ma addirittura il 200 per cento sulle maggiori entrate dello Stato. I conti vanno fatti sapendo leggere i numeri e non fantasticando a destra e a manca. Qualcun altro sostiene anche che questa sia stata una misura da Robin Hood al contrario. No: l'avete resa voi una misura da Robin Hood al contrario, che ha favorito solo le fasce ricche della popolazione, perché noi l'abbiamo pensata per tutti, prevalentemente per le fasce povere, perché lo sconto in fattura serve a chi non ha capienza fiscale. Chi non aveva il capitale ha ceduto il credito all'azienda che ha fatto i lavori o alle banche, anche facendoselo decurtare. Coloro che avevano il capitale, i ricchi amici vostri, se lo sono scaricato da soli, tenendosi il profitto del 10 per cento. Quindi chi ha cancellato lo sconto in fattura siete voi! I Robin Hood al contrario, che fanno i favori ai ricchi, siete sempre voi! Lo dimostrano i 28 miliardi di utili delle banche a cui voi non avete voluto tassare gli extraprofitti. *(Applausi)*. Togliete il reddito di cittadinanza e lasciate 28 miliardi di utili aggiuntivi alle banche. Siete voi che favorite i ricchi e aumentate la povertà! Abbiate il coraggio di metterci la faccia e dirlo ai cittadini italiani. Diteglielo!

roboante, vorrei ringraziare con questo intervento tutto il Governo e *in primis* il ministro Giorgetti, soprattutto per aver rinviato la *sugar tax*

La *sugar tax*, in particolare, venendo incontro a quello che è stato un emendamento che come Lega abbiamo depositato, intendeva cercare di tutelare un intero comparto che era in subbuglio, vista la notizia che era comparsa.

Bisogna trovare cioè le rispettive e opportune coperture. Abbiamo anche fatto una sorta di provocazione, che qualcuno ha letto in questo modo; se cioè c'è difficoltà a reperire le risorse, noi abbiamo sostanzialmente messo in evidenza nel nostro emendamento che possiamo anche cercare di ridurre magari le spese per le missioni internazionali. In un momento di difficoltà infatti, forse è meglio prima guardare a casa nostra e poi magari guardare all'estero (tendenzialmente bisognerebbe cercare di ragionare in questa maniera). Poi il Governo ha trovato le risorse con altri capitoli di spesa. La riformulazione l'abbiamo accettata e siamo assolutamente soddisfatti, perché comunque non erano scontati né il rinvio della *plastic tax* né tantomeno quello della *sugar tax*. Quindi complimenti al Governo. Visto che c'è una sorta di giochino

anzi, sono due, perché cerco di essere riconoscente in politica - è proprio il ministro Giorgetti, che fin dall'inizio ci mostrava le tabelle, facendo capire che questa misura avrebbe inevitabilmente portato tempo delle difficoltà di bilancio. Quindi è vero che era Ministro del Governo Draghi, però ricordiamoci che il Governo Draghi cade perché il MoVimento 5 Stelle decide di non dargli più la fiducia. Quindi, vuol dire che la linea politica del Governo la dettavate certamente voi e non eravamo noi a essere incisivi, come probabilmente qualcuno può pensare e immaginare.

arrabbierà. Quindi, avremmo dovuto fare esattamente il contrario se avessimo guardato solo l'interesse elettorale. Però qui c'è in campo un interesse che è ben più alto di quello elettorale ed è l'interesse di un Paese. Guardate che i debiti da non ce li siamo inventati noi: sono certificati nel 2023 da Eurostat, che rivede il *deficit* al rialzo di 40 miliardi, proprio perché verifica i conti dello Stato. Eurostat non è una maggioranza di Governo, ma è un ente che sovrintende

a toppare clamorosamente su una misura come questa. Non so chi era a capo della Ragioneria; la politica c'entra - lo dico sempre - fino a un certo punto, poi ci sono anche i tecnici e i funzionari. Sappiamo bene quante volte volevamo approvare qualcosa, ma non l'abbiamo potuto fare perché ci veniva opposto il *niet* sostanzialmente chiaro e deciso da parte della Ragioneria: non si può, non c'è la copertura, la stima non è corretta, la relazione tecnica non regge e quindi non si può fare.

quasi come la cifra intera messa in campo sul PNRR, vuol dire che qui c'è stata una svista clamorosa. O forse c'è un errore politico in partenza, che è quello di non aver fatto conto di un meccanismo di autorizzazione di questa misura, e quindi, succede che ogni anno lo Stato scopre all'ultimo minuto

di fronte a questo, in campagna elettorale - e lo dico a tutti, anche agli alleati - sarebbe molto più facile dire che proroghiamo, andiamo avanti, aspettiamo le elezioni. di fronte a una spesa fuori controllo, un buon padre di famiglia cosa dovrebbe fare? Cerca di mettere a posto i conti, soprattutto alla luce del fatto che abbiamo, con il Patto di stabilità europeo e con la crescita del debito, tutta una serie di occhi puntati contro di noi che non ci consentono di avere un margine di manovra tale da pensare alle campagne elettorali. Noi abbiamo la necessità di tenere i conti in ordine. Ho sentito molti dire bisogna aiutare le famiglie più bisognose, che bisogna continuare a prevedere le misure per quelli che rischiano di soffrire, le bollette che salgono, i costi energetici... sì, però dopo, per mantenere certe misure che abbiamo messo in campo e per prevederne delle altre, abbiamo necessariamente bisogno di avere i conti in ordine. Questo è stato il meccanismo: alleggerire il debito, soprattutto nel prossimo triennio, che è quello più complicato alla luce di tutto quanto a livello internazionale sta accadendo. Questo è stato il ragionamento del ministro Giorgetti. Capisco che qualcuno Ma avere la responsabilità di un Dicastero così importante significa anche fare qualcosa che può apparentemente risultare impopolare, ma finalizzato al bene dei cittadini. Se poi va in *default* lo Stato italiano; se non abbiamo i soldi per pagare gli stipendi e le pensioni; se poi non ci sono più soldi per mantenere certe misure, chi glielo va a spiegare ai cittadini che bisognava intervenire prima? È la stessa cosa che avremmo dovuto fare prima sul superbonus, che però non si è riusciti a fare e che questo Governo, appena presa in mano questa patata bollente, ha cercato - con difficoltà, perché non è assolutamente semplice risolvere problemi del genere - pian piano di mettere in campo delle contromisure che potessero in qualche modo limitarne gli effetti sotto la finanza pubblica, tutelando sì le imprese, per esempio con lo spalmare i crediti d'imposta da superbonus in dieci anni. Io ho letto su «Il Sole 24 ore» - non sono un tecnico, però mi piace ogni tanto leggere e studiare alla fine, chi viene penalizzato in minima parte sono soprattutto le banche che, anziché compensare in quattro anni, dovranno compensare

Questo è quello su cui noi vogliamo puntare. Quindi, con molta serietà si fanno le manovre, anche impopolari, ma alla luce di un risultato importante. Questo Governo vuole andare avanti con le proprie misure, si vuole impegnare. Il debito, grazie a questa misura, anziché salire dal 137,3 al 137,8 scenderà quest'anno al 137,2 perché ci sono anche i mercati internazionali. Io sento qualcuno dall'altra parte dire di fare attenzione, che c'è l'Europa, ci sono i mercati, dobbiamo stare attenti, il Paese rischia di non avere la fiducia. E allora non si può avere - come dico sempre io - la solita logica italiana per cui io voglio la botte piena e la moglie ubriaca. No, bisogna essere seri e fare le cose come si devono fare. Bisogna prendersi la responsabilità per questo? Lo si fa e sicuramente un Ministro come Giorgetti le cose le sa fare bene, così come il presidente del Consiglio Meloni, che indubbiamente vuole andare nella direzione di far sì che si possano avere le risorse per prorogare altre misure. Le banche hanno avuto - ci tengo a dirlo - lauti guadagni - come leggo sempre da alcuni giornali - dalla circolazione dei crediti e sono state esentate dal rispondere delle truffe ai danni dello Stato. Tra l'altro, E poi abbiamo previsto una serie di controlli, il coinvolgimento degli enti locali nei controlli, con la possibilità di trattenere sul territorio una parte che ci possono dare una mano. Questo può essere importante, per controllare chi ha truffato lo Stato, magari qualche difformità qualche situazione particolare. È giusto farlo, perché si dice sempre che bisogna aumentare i controlli. Con questo provvedimento noi ci avvaliamo della collaborazione degli enti locali proprio per aumentare i controlli sul territorio e, a fronte di controlli di truffe ben effettuati, gli enti locali avranno delle agevolazioni dirette e tratterranno delle risorse sul sul territorio. Questa è, sì, una misura che vuole venire incontro per cercare di risolvere il tema. Non è una misura propagandistica o populistica. Tutti avrebbero voluto portare avanti tutto quello che si voleva. Sento dire che si vogliono aumentare le pensioni, avanti col superbonus, tiriamo via questo, soldi di qui, soldi di là. Questo lo comprendo, ma, a un certo punto, bisogna trovare le coperture - la coperta è corta, e lo sappiamo - e i conti devono rimanere in ordine. Questa è la priorità di questo Governo ed è il motivo per cui mi avvio alla conclusione - oggi il ministro Giorgetti ha tenuto a precisare che le previsioni della Commissione europea sono in linea con le nostre. Naturalmente sul debito gravano questi aspetti del superbonus, però i dati europei sul rapporto debito-PIL, quelli gli effetti di questo provvedimento, che sarà positivo per i prossimi tre anni. Quindi possiamo stare tranquilli? Sì. Per quale motivo? Abbiamo avuto il coraggio di intervenire, anche a rischio di perdere magari qualche voto elettorale. Presidente, senatori, senatrici, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grandissima attenzione l'intervento che mi ha preceduto del capogruppo della Lega, il senatore Romeo. E devo dire che praticamente sarebbe stato molto meglio se questo intervento lo avesse fatto in una riunione della maggioranza di Governo e se lo avessero fatto i suoi Ministri in quello che è il luogo preposto per fare questo dibattito, cioè il Consiglio dei ministri. Noi abbiamo passato le ultime settimane e le ultime ore prigionieri in in Commissione finanze, perché i nodi non risolti della maggioranza si sono tutti scaricati su questo Parlamento e sulla stampa italiana, tra l'altro in un dibattito che ha creato soltanto un elemento sicuro: una grandissima incertezza su quello che sarà il futuro della grande della grande questione della cessione del credito in Italia e, quindi, della stabilità economica e finanziaria delle nostre banche e delle nostre imprese; non per ultimo, quello che accade ai cittadini che hanno cantieri aperti nelle loro abitazioni. Questo è il primo dato politico di questa vicenda: la maggioranza, invece di arrivare in Parlamento con un pacchetto di proposte e misure volte a risolvere i nodi del 110, in realtà ci ha scaricato le sue tensioni qui, fino fino al punto che ieri si aveva l'aggiunto, cioè l'aiutino e il rinforzino in Commissione con la nomina subitanea, poi interrotta dal Presidente del Senato, di un consigliere in più in quota Fratelli d'Italia, per coprire la posizione di Forza Italia. Voglio dire che in questo momento nel dibattito Forza Italia sin dall'inizio non è stata presente. *(Applausi)*. La situazione è tale che comunque verrà messa la fiducia su questo provvedimento. E ciò la dice lunga sulla solidità di questa maggioranza su cose fondamentali e strategiche, come non solo la visione sul debito e sulle entrate e le uscite del nostro Paese, ma anche la visione strategica in campo energetico, sul rischio sismico, sulla sicurezza delle nostre abitazioni, nonché - lo dico sommessamente - sul comparto edile, che dà edile, che dà lavoro, in un modo o nell'altro, a circa il 90 per cento delle piccole e medie imprese del nostro Paese, le quali si trovano da oggi in una situazione di grandissima incertezza e di grandissima preoccupazione. Andiamo al merito. A parte l'intervento del senatore Romeo, che almeno ci ha messo la faccia, questo di oggi è un dibattito da Topolinia. Si è parlato della proroga della *sugar tax* e della *plastic tax* come di una grandissima conquista - una norma che ancora non ha mai visto la luce nel nostro Paese - ma non si è entrati nel merito merito della spiegazione agli italiani di un provvedimento che riguarda milioni di cittadini. Nessuno ci ha messo la faccia. Do atto al senatore Romeo che almeno lui l'ha fatto. In questo contesto, poi, vorrei dire alcune cose: io non sono una che vuole difendere ad oltranza il 110 per cento contro tutto e tutti. Se c'è una cosa che non sopporto è l'ideologizzazione delle norme, quando le norme diventano feticcio. Le norme hanno uno scopo, servono a qualcosa; sono strumenti, possono cambiare e possono essere modificate nel corso del tempo in base alle necessità. Però non posso neanche ascoltare una mistificazione e una demonizzazione di quella che è stata in Italia una realtà. Il superbonus è stato introdotto nel 2020 dal Governo Conte II come una leva economica, cioè come un grande strumento di leva economica e finanziaria per sollevare l'Italia da una fase difficilissima, perché l'Italia - non so se ve lo ricordate - era chiusa in casa, la nostra economia era bloccata e serviva uno *shock test*. È servito lo *stress test*? Signori, siete venuti qui durante la legge di bilancio - la vostra prima legge di bilancio, che era ancora quella di Draghi - a dirci che l'Italia aveva avuto una crescita esponenziale del PIL con *record* mai registrati prima, arrivando a più del 12 per cento, cioè una crescita che noi abbiamo visto solo nel momento del *boom* economico dopo la seconda guerra mondiale. Quindi, probabilmente, poiché gran parte di questo volano è stato introdotto da questo strumento, ciò ha funzionato. Ha funzionato, ma guardate che la cosa più innovativa del 110 per cento non è stata l'aliquota, che sicuramente è stata piuttosto appetibile, ma è stata la cessione del credito; è stato lo sconto in fattura, la cessione del credito. *(Applausi)*. Quello è stato lo strumento che ha permesso ciò di cui parlava prima la la senatrice Pirro, cioè a persone che non avrebbero mai avuto la possibilità di mettere in sicurezza gli edifici in cui abitavano - pensiamo ai condomini popolari, tra l'altro quelli più colpiti da quest'ultima manovra - di farlo, o a persone o famiglie che non avrebbero avuto la possibilità di mettere

che ha scatenato una grande leva democratica. Ricordo che gli italiani sono per la maggior parte proprietari della propria casa, perché la casa è stato l'elemento di risparmio degli italiani. Ci può piacere o no, ma questa è la nostra storia: le persone si sposavano, accendevano il mutuo per tutta la vita

Siffatto strumento ha permesso, grazie alla sua entrata in vigore, di raggiungere questa leva e di far lavorare milioni di persone.

all'ultimo dei lavoratori, tutti tracciati, tutti a contratto e senza nero, perché in questa misura il nero non paga. Guardate bene che un'altra cosa fatta nei *bonus* - secondo me, è un grosso errore - è aver tolto il 50 per cento delle detrazioni dalle ristrutturazioni ordinarie delle case, arrivando al 36-30 per cento. Io ricordo il dibattito di quel provvedimento: quando si mise quella era per sconfiggere il nero e la quota era data non per fare un regalo a qualcuno, ma era una soglia che consentiva di dire che così non si facevano più i lavori in nero, perché alla gente non conveniva e si è fatto emergere PIL. le argomentazioni riguardano il timore di capire esattamente, perché non riusciamo a capire quanto questa misura ha cubato in maniera limpida. Perché non sappiamo esattamente non soltanto quanto esce e quanto si prende di cessione, ma quanto

ho scoperto che il Servizio studi della Camera ha certificato anno per anno il saldo di tutti gli interventi dei *bonus* in Italia, partendo dal passato. Sul 2021 - quindi rimango al 2021 - il saldo dato non solo dalle entrate e dalle uscite di cassa della Ragioneria, e via dicendo, ma anche dall'impatto di quanto noi abbiamo cubato dalla gente che ha pagato le tasse, ha lavorato, dalle cedolari dell'IVA e tutto il

Fermo restando che sicuramente tutti eravamo d'accordo - e lo abbiamo fatto anche durante il Governo Draghi - nell'operare un *décalage* di questi provvedimenti, una cosa non andava fatta: l'accelerazione, cioè la rincorsa. Durante la rincorsa dell'accelerazione a cambiare le regole in corsa, infatti, è accaduto che chi poteva fare tutto in sei mesi ha fatto tutto in sei mesi e quindi a chi doveva monitorare - e noi non c'eravamo più - è saltata la bussola dell'orientamento di quello che stava

in questo Paese e come verrà fatto per garantire l'efficienza energetica dei nostri edifici, per affrontare il costo dell'energia in modo strutturale e per risolvere una questione enorme del rischio sismico e

il coraggio di fare iniziative a leva, parlare dell'economia delle imprese, dare forza, energia e certezza di regole. Un Paese che cambia le regole ogni cinque minuti è un Paese in cui non si può investire, è impossibile fare investimenti e infatti si va via.

partire dall'ultimo intervento della collega Lorenzin, che ho visto sinceramente un po' in imbarazzo rispetto ad alcuni interventi che credo ormai

oggi soprattutto il Partito Democratico debba ringraziare la serietà di questa maggioranza di Governo che su una cosa che non funziona, alla vigilia della campagna elettorale, si assume la responsabilità di dire basta. Rispetto a questo provvedimento una cosa è certa:

poco rispetto. Ebbene, rivendicano due provvedimenti che vanno considerati nella dimensione di quest'Italia che ha diverse stagioni politiche. Ringrazio anche il contributo che è arrivato da Italia Viva in Commissione, che ha rivendicato di non essere in maggioranza e sceglie e vota rispetto ai singoli provvedimenti che sono utili al Paese. Credo che dobbiamo smetterla di fare un racconto di quel si è parlato di un incidente nella maggioranza, e io penso ai colleghi di Forza Italia, anche noi eravamo utilitaristi: potevamo dire che di spese fiscali ne avevamo fatte per circa 760 miliardi negli ultimi anni potevamo decidere di continuare ad aggiungerne 12 o 15, per cui io plaudo al rigore, alla compostezza, alla misura del ministro Giorgetti; al rigore, alla compostezza, alla misura del *premier* Meloni e di tutti i Ministri della maggioranza. Sarebbe stato facile speculare su un provvedimento che - come è

che questo Governo potrà fare e immaginare mettendo in sicurezza i conti del Paese rispetto agli investimenti internazionali; lo *spread* che è andato tanto di moda oggi è in sicurezza, e sono tutte cose per cui la gente ci guarda. Come Come diceva anche il collega Romeo, questa è stata una delle più grandi speculazioni. Se voi andate in giro e chiedete alle imprese serie, vedete che sono poche le imprese che si sono avventurate su questo strumento. Abbiamo visto e ascoltato vicende di un negozio di generi alimentari e si sono messe a fare i superbonus con i consorzi, con tutti i *broker.* Questo, quindi, è un provvedimento che nasce oggettivamente male e a cui, con grande responsabilità, si mette la parola fine e questo serve a tutti, e servirà anche a voi. Io penso - spero

Concordo anche con i colleghi di Italia Viva sul fatto che bisognerà intervenire con ulteriori nuovi provvedimenti per mettere in sicurezza le imprese e rispetto al rapporto con le banche. Il Governo Meloni, rispetto a quella norma che chiedeva di mettere in campo un minimo degli extra profitti, ha fatto una scelta coraggiosa. Insomma, è intervenuta. Poi sappiamo che c'è stata la scelta delle banche di mettere le risorse e quindi rafforzare la struttura bancaria. tutte politiche serie che un Governo, che vuole guardare a una prospettiva di medio e lungo periodo, mette in campo; con la serietà di Giorgetti, che dice basta,

gli amici del popolo, o chi frequenta soltanto i poveri, insomma, è davvero surreale. Questo provvedimento non solo ha interessato circa 2.360.000 italiani; rispetto anche alla difesa d'ufficio, non ha interessato le prime case dei

cosa si poteva fare con 200 miliardi di euro su quelle 124 aree interne, con 1.930 Comuni e 4 milioni e mezzo di italiani, di cui il 50 per cento è popolazione anziana, per intervenire sui trasporti; insomma, tutto quell'effetto leva che

elementi di serietà che noi proviamo a mettere nel dibattito politico. Si confrontano due visioni diverse. La nostra è maggioranza in Italia e oggi, proprio alla vigilia delle elezioni europee, la responsabilità di un Ministro, di un Governo, di fare anche una scelta impopolare, per mettere fine a una misura che non ha mai funzionato all'inizio, penso sia un elemento di serietà. Con questa dimensione, un Paese con una grande storia esisteva prima di noi - qualcuno richiamava

nell'utilizzare le prerogative di Regolamento. Il presidente La Russa le ha messe a posto ipotizzando che la nostra Commissione possa avere, già per le future sedute, un nuovo membro. Grazie al relatore Salvitti, grazie al lavoro della Commissione e proviamo ad andare avanti.

non è mai un provvedimento impopolare: mai, assolutamente mai. *(Applausi)*. Quanto ho ascoltato è quella che probabilmente avrebbe dovuto essere la finalità con la quale era

non facilitando le fasce più deboli e non lasciando alcun tipo di punto di riferimento che potesse comunque facilitare l'intervento sulle fasce più deboli della nostra società, ha generato il fatto che chi aveva la capacità di carattere progettuale potesse mettere

questa maggioranza a mettere un freno rispetto a questo provvedimento. Semmai ci fosse stato un errore da parte di questo Governo, è stato quello di non essere intervenuti lo scorso anno in maniera così decisa in modo tale da bloccare il declino. il declino. *(Applausi)*. Non c'era un controllo da parte di nessuno. Non c'era il controllo primario, che è quello di chi usufruisce poi del bene rivalutato rivalutato dal punto di vista edilizio e energetico. Abbiamo visto prezzi schizzare alle stelle perché non c'è stato più un controllo, nemmeno quello primario, di chi usufruiva del bene stesso.

quello che adesso è nelle loro possibilità, potremmo sicuramente recuperare molto più rispetto a quanto è stato recuperato fino ad ora ed eventualmente mettere quelle somme a disposizione delle fasce della nostra società che non hanno le possibilità di mettere a posto le proprie case ed efficientarle secondo quanto previsto dagli indirizzi europei. Andremo avanti con dei provvedimenti in questo senso, in modo tale da rilanciare da rilanciare un settore che raggiunge l'obiettivo europeo delle case *green*, e lo faremo sicuramente utilizzando anche quanto ci ritorna dall'emersione delle frodi.

a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1092, di conversione del del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020,

nuova finestra"). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39, nel testo proposto dalla Commissione.

stante la circostanza temporale, ricordando un grande italiano che oggi avrebbe compiuto trentacinque anni, Antonio Megalizzi. Credo sia doveroso ricordarlo, indipendentemente dalle contingenze della nostra vicenda di oggi, proprio perché, alla vigilia di un appuntamento elettorale come quello al quale gli italiani e gli europei sono chiamati i prossimi 8 e 9 giugno, gli ideali di Antonio Megalizzi, la sua testimonianza e il suo sogno spezzato possono in qualche misura essere ricondotti dentro la nostra esperienza e l'impegno a far sì che la sua memoria non resti qualcosa di incompiuto. Fatta questa chiosa, che ritenevo in ogni caso indispensabile, vorrei sottolineare alcuni aspetti tutti politici rispetto all'atto che è stato appena annunciato in questa sede dal Governo, di fronte ai banchi totalmente vuoti di Forza Italia, un partito di maggioranza che non ha partecipato, lasciando a tutto il resto della maggioranza e all'opposizione il compito di intervenire in discussione generale, e che non ha ascoltato i rimbrotti, le frecciate e i richiami che gli esponenti autorevoli di Fratelli d'Italia e della Lega gli hanno indirizzato in questa sede. Probabilmente lo leggeranno attraverso le agenzie, ma resta un fatto prima politico di una fiducia che è forse - anzi, toglierei il dubitativo - totalmente imposta dal Governo contro la propria maggioranza. nelle sue diverse accezioni e sfumature... *(Commenti).* Contro la propria maggioranza, senatore Romeo, perché non si fida di un pezzo significativo della propria maggioranza.

È contro la propria maggioranza perché, come dicevo, le minoranze, sia pure in un quadro di diversa interpretazione, diversa impostazione e diverso approccio sul merito dei contenuti di questo provvedimento, certamente non avevano causato nessun atto ostruzionistico e certamente non si sono poste in una dimensione tale da impedire una corretta attività di prosecuzione di quest'Assemblea nella conclusione di un corretto e normale procedimento di traduzione in legge dei lavori che sono usciti dalla Commissione. È di tutta evidenza quello che è accaduto nei giorni precedenti all'inizio dei lavori e cioè lo scontro - perché di questo bisogna parlare - tra il vice premier Tajani, che ha parlato a nome di Forza Italia, il ministro Giorgetti, che ha rimandato al mittente le osservazioni del Vice premier, il quale ha tenuto a precisare che la proposta fatta dal ministro Giorgetti non era quella del Governo, ma era del Ministro *uti singuli*, poi stato smentito in questa sede. Infatti, il vice premier Tajani e Forza Italia sono stati totalmente smentiti dal resto della maggioranza, ma si sono assunti l'onere - e questo lo riconosciamo - di procedere nonostante l'atteggiamento ostruzionistico di Forza Italia, nonostante le iniziative finalizzate a impedire la prosecuzione e nonostante le bugie che Forza Italia ha voluto trasmettere all'esterno del Senato, con la complicità di un servizio pubblico *(Applausi)* che è riuscito a dire agli italiani che quel partito che non ha partecipato al voto in Commissione era stato determinante per il rinvio della *sugar tax*. Ora, è la prima volta che nella Repubblica italiana accade che un partito che non vota un provvedimento diventi il protagonista degli effetti giuridici. *(Applausi)*. Siamo arrivati alla trasformazione della realtà grazie al servizio pubblico e, vorrei dire, anche grazie a qualcuno che si è dimenticato che nel servizio pubblico esiste semplicemente il contraddittorio. Bisognerebbe soltanto mettere chi era ieri sera in Commissione a fianco di chi ha reso alcune dichiarazioni e raccontare le cose come sono, perché gli italiani hanno il diritto di sapere, attraverso il mezzo fondamentale del nostro servizio pubblico, la verità e ce l'hanno sia in quanto è un loro diritto soggettivo, sia in quanto sono soggetti contribuenti che pagano non per avere il bollettino e la velina del partito di governo, ma per conoscere la realtà. Quindi è inevitabile che, di fronte a quello che è accaduto ieri, si siano palesate le situazioni che oggi il ministro Ciriani è stato costretto a mettere in campo, ricondurre alla ragione, attraverso lo strumento coattivo della fiducia, un pezzo di maggioranza che, recalcitrante, nella serata di ieri non ha votato l'emendamento del Governo che conteneva una serie di questioni. Lo vorrei dire anche per sgombrare il campo rispetto ad alcune interpretazioni un po' facilone che ho sentito nel corso di queste ore all'esterno di quest'Aula. Noi

ma non abdichiamo al nostro diritto-dovere di partecipare al processo legislativo con le nostre idee, con le nostre proposte e con i nostri suggerimenti migliorativi, perché è a questo che serve il Parlamento ed è a questo che serve, almeno nel nostro concetto, un'opposizione che non si chiude dentro una logica rigida di contrapposizione, ma mette sul campo una serie di misure e sfida la maggioranza

noi siamo comunque riusciti, facendo una battaglia, a inserire tre questioni che il Governo non aveva previsto. Il Governo non aveva previsto l'estensione del sismabonus a tutte le zone terremotate per le quali era stato emanato il provvedimento di emergenza. C'era il rischio che pagassero i pagassero i più deboli in una filiera nella quale si rischiava di scaricare -anche su quelli che non c'entrano nulla con la vicenda del superbonus - una situazione per la quale lo Stato si era impegnato in un processo di ricostruzione, di sostegno e di ausilio, che rischiava però di venir meno. Noi abbiamo fatto la battaglia per estendere il sismabonus a tutte le zone terremotate. Noi abbiamo chiesto che venisse introdotto il terzo settore all'interno di questo segmento, con specifiche agevolazioni. Sono sufficienti? No. Bisogna fare di più? Sì. È stato fatto qualcosa? Sì. Un riformista non pretende tutto subito. Un riformista fa le battaglie per introdurre progressivamente, in maniera omogenea, il miglioramento della realtà. *(Applausi)*. Infine, e rivendico a pieno titolo la nostra paternità su questa scelta, noi siamo stati determinanti per il rinvio della *sugar tax*. *(Applausi)*. Se non ci fossimo stati noi, oggi gli italiani pagherebbero di più e Forza Italia, che oggi abbandona il dibattito e che ieri ha abbandonato la Commissione, dice una falsità, perché, se fosse andata come volevano loro, oggi gli italiani pagherebbero la *sugar tax,* perché inevitabilmente tutto questo non si sarebbe potuto realizzare. Insomma, abbiamo fatto tre cose concrete, che aiutano le persone e che non alzano le tasse. A quel punto, una volta ottenute, che cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto buttare tutto nel cestino? Ci ha insegnato Alcide De Gasperi che la politica vuol dire realizzare. Poi c'è la politica politicante, quella che insegue il *gossip* o quella che pensa alle tattiche asfittiche delle rincorse nei corridoi, dei *tweet*, degli *spin* e degli *influencer*. noi abbiamo voluto mettere in campo in queste ore una differenza tra chi, anche all'opposizione, ha una cultura di Governo e chi, restando al Governo, ha invece una cultura dell'opposizione. È su questo punto, signor Presidente, che noi, nel momento in cui vogliamo denunciare la situazione che si sta realizzando all'interno di quest'Aula, riteniamo di dover sottolineare e rivendicare. Nel momento in cui annunceremo, come faremo domani, il voto contrario rispetto al provvedimento e alla fiducia, vogliamo anche dire che, di fronte a una maggioranza sfibrata che è andata in atto in queste ore, si può stare in due modi, che sono entrambi legittimi, ma che, come tali, non possono essere demonizzati dagli uni, né dagli altri. Si può pensare di fare il muro contro muro, con il risultato di compattare una maggioranza incrinata, o si può scegliere di entrare negli interstizi delle contraddizioni altrui, in nome del bene comune e per dilatare le sue contraddizioni. Un riformista fa questa cosa.

una scelta oligarchica, un errore drammatico, una vergogna, diceva nel 2017. Peggio ancora nel 2021: addirittura, una mortificazione del Parlamento, una deriva antidemocratica. deriva antidemocratica. Deve aver cambiato idea. Giusto: si può cambiare idea; è possibile, dato che ora il Presidente del Consiglio, per frenare quello che è successo ieri

Qui ognuno ovviamente rivendica i suoi, però molti emendamenti erano uguali per tutti i Gruppi, di opposizione in particolare. Devo dire che c'erano tutte le condizioni per fare una discussione di merito e per trovare soluzioni

mancata per tutto il giorno una forza di maggioranza, che ieri ha rivendicato di aver fatto passare certe norme. Questo è il dato che dovete dire ai cittadini e alle Vi siete sciacquati la bocca molto spesso con orgoglio e io sottolineo questa cosa, l'ho sempre detta e la ridico: voi avete sempre detto tecnici, ci sono Governi politici, noi siamo un Governo politico e dureremo tutta la legislatura". Però, Presidente, Ministro, quante fiducie avete messo fino ad oggi? Questo è l'antipasto del premierato? Cioè decidete sostanzialmente nel Governo e poi, di fatto, mortificate il Parlamento, perché gli impedite di contribuire? Tra maggioranza e opposizione dev'essere chiaro che non ci devono essere pasticci. Io su questo non concordo con chi ha votato a favore, cioè c'è un problema

hanno tale caratteristica. Avete posto la fiducia di fronte a questi dati e quasi sempre c'è di mezzo la questione del famoso superbonus. Allora il problema è politico, non è una questione sul merito,

ragione, non è accettabile un simile modo di utilizzare le fiducie. È una mortificazione nei confronti del Parlamento e dei parlamentari.

questa è imposizione della maggioranza nei confronti dell'opposizione. Non vogliamo sovvertire il risultato, che noi diventiamo maggioranza e voi opposizione. È una dialettica che deve trovare però un confronto di merito, su una questione imposta. Per questa ragione, non vi permetteremo di continuare ad andare avanti così. Lo abbiamo già spiegato, l'ha già detto il mio Presidente

durante la discussione generale su questa fiducia, in due parti nette e distinte. La seconda riguarderà il merito e alcune cose di questo decreto, che non concerne il superbonus al 110 per cento, perché dal 31 dicembre 2023, com'è noto, non vi sono spese che possano essere accompagnate dal 110 per cento, se non per le aree terremotate. Questo provvedimento riguarda altre spese, quelle con i *bonus* quasi ordinari, con il *décalage* oggi al 70 per cento, e quindi continuare a dire che stiamo mettendo un freno al 110 per cento è nelle cose una stupidaggine. La prima parte dell'intervento non può non essere dedicata al metodo e al motivo politico per cui oggi stiamo discutendo questa questione di fiducia, perché la questione di fiducia sui provvedimenti viene posta normalmente in un ramo del Parlamento, la Camera dei deputati, perché gli strumenti ostruzionistici, che sono più incidenti ed invadenti, forse, dei lavori parlamentari, possono possono mettere a rischio l'approvazione di un provvedimento nei termini di scadenza, come un decreto-legge dopo sessanta giorni. Vi sono ventiquattr'ore di fermo delle attività, vi sono gli ordini del giorno e il doppio voto. La questione di fiducia si pone quindi quando quegli elementi ostruzionistici incidono sulla possibilità di conversione del decreto-legge in quest'Aula, perché magari si deve accelerare per via di un monte emendativo molto alto e allora, pur non essendoci strumenti in mano alle opposizioni, si ritiene di voler chiudere prima la discussione, magari per approvarlo in poco tempo oppure per inviarlo alla Camera, che avrà l'onere di convertirlo in sede definitiva. cento dei casi, le motivazioni con cui si pone la questione di fiducia. Questo è il primo caso in questa legislatura e non ne ricordo altri

si è manifestato plasticamente anche durante la discussione generale di oggi, quando nessun esponente di Forza Italia è stato mai presente in Aula,

da quel componente della Commissione, introdotto con lettera del presidente Malan al Presidente del Senato, che va ringraziato, perché per fortuna ha fermato quello che era uno scempio democratico e istituzionale.

un Ministro della Repubblica, quello dell'economia e delle finanze, attraverso la stampa ha detto al Vice Presidente del Consiglio, nonché Ministro degli affari

una persona seria e rigorosa. Sono certo che c'era una condivisione e che quindi tutto è diventato un caso politico in funzione elettorale per le elezioni europee che stanno per arrivare e ciò riguarda esclusivamente la maggioranza.

fosse tempo di discutere cinque emendamenti. Il tempo c'era, non c'era la fiducia nelle forze politiche di maggioranza. Questo è ciò che è accaduto oggi: non c'era la fiducia. Dopodiché è chiaro che ci sono dei Gruppi di finta opposizione che vanno in soccorso alla maggioranza quando serve e mi riferisco ovviamente al Gruppo Italia Viva, che ha votato quando non c'era la certezza dei numeri un altro componente del Gruppo per le Autonomie ha deciso di non partecipare all'ultima fase della discussione, a garanzia del fatto che ci sarebbe stata comunque una maggioranza, nonostante il fatto che Forza Italia con il suo unico componente poteva non votare quel testo.

dell'entrata in vigore della *sugar tax,* che la sua attività è stata quella di astenersi sull'emendamento che dispone tale proroga; pertanto, casomai, è nonostante Forza Italia, come giustamente ha detto il presidente Garavaglia in Commissione, che quell'emendamento è stato approvato. Veniamo al merito, perché penso di avere ancora pochi minuti a disposizione,

non solo non tutte le frodi, ma il 95 per cento di quelle frodi non riguardano il 110 per cento, che è nato con una serie di strumenti di controllo come nessun altro provvedimento in questo Paese, con l'asseverazione del progettista, l'asseverazione del tributarista, le comunicazioni all'Agenzia e le possibilità ispettive dell'Agenzia e di ogni possibilità ispettive dell'Agenzia e di ogni organo ispettivo, compresa la Guardia di finanza. *(Applausi)*. Che non ci fossero regole e che non ci fossero controlli è quindi assolutamente falso, anche perché, se ci sono tentativi di truffa come su ogni misura dello Stato, evidentemente i controlli ci sono. A chi dice basta spese gratuite, ricordo che c'era qualcuno che il 30 marzo 2020 scriveva una lettera all'allora Presidente del Consiglio dicendo che con un *click* molto

per cento, che con la detrazione fiscale e con tutte quegli elementi che, come il Centro studi della Camera e lo studio del Cresme hanno dimostrato in modo plateale, ha portato un beneficio economico. Qui il tema vero è stata la cessione dei crediti, su cui è evidente che c'è stata una forzatura a livello europeo che ha messo il nostro Paese sotto la lente di ingrandimento, ma ricordo che qualcuno diceva che per l'Europa la pacchia era finita, riferimento a temi che non riguardavano per nulla l'economia, ma questa volta sarebbe dovuto andare in Europa a dire che la pacchia è finita e che la cessione del credito è uno strumento che agevola anche i non abbienti su ogni su ogni misura fiscale, su ogni misura del credito d'imposta (Transizione 4.0 e tutti i crediti di imposta sull'edilizia, anche quelli a 70, al 65, al 50 per cento, altrimenti chi non ha capienza fiscale non potrà mai utilizzare quelle misure). Per il suo tramite, Presidente, vorrei ricordare al di quel provvedimento, che è nato per finire il 31 dicembre 2021 ed è stato gestito dalla Presidenza del Consiglio di Giuseppe Conte e dal MoVimento 5 Stelle fino al febbraio del 2021, dopodiché c'erano altri, come il ministro Giorgetti, che da quaranta mesi ha in mano quella misura, ma evidentemente non ha saputo intervenire per evitare quello che oggi definisce un buco di bilancio. *(Applausi)*. Quella misura, quando è nata, in quella fase, aveva una scadenza temporale certa, aveva

di migliorare le condizioni del nostro patrimonio edilizio, cosa che oggi ci vedrà in vantaggio rispetto alla direttiva Case *green*, che in un modo o nell'altro dovrà andare avanti, e aveva soprattutto un effetto dirompente sulla crescita economica che era necessaria in una fase successiva alla pandemia che aveva distrutto l'economia italiana. Quella misura ha rilanciato l'edilizia, settore industriale fondamentale di questo Paese, che era in crisi dal 2008 e l'ha portata ad essere il vero

in campagna elettorale, promettere delle cose e dopo dire che è arrivato il tempo della responsabilità. Quella responsabilità la stanno pagando i cittadini italiani. Signor Presidente, penso di poter condividere con le senatrici e i senatori presenti che tutto avremmo voluto in queste ore, tranne che fare un dibattito più politico sulle responsabilità della maggioranza e non di merito su un decreto-legge che poteva anche avere un senso se avesse avuto una finalità non strumentale. «Il superbonus è fondamentale. L'edilizia è cresciuta del 15 per cento. Se uno truffa, bisogna prendersela con il truffatore, ma il superbonus è fondamentale» (Matteo Salvini, febbraio 2022). «Siamo pronti a tutelare i diritti del superbonus e a migliorare le agevolazioni edilizie. Il superbonus ha avuto un senso» (settembre 2022, Giorgia Meloni). Potrei continuare all'infinito, solo per ricordarvi il sostegno ad un provvedimento che è diventato la bandiera del ministro dell'economia Giorgetti, il

quindi una di quelle personalità della maggioranza che ha più cognizione di quello che è successo negli ultimi quattro anni, che sono i quattro anni che sono quelli in cui mettete in discussione gli effetti del superbonus. Dico questo perché, signor Presidente, l'ipocrisia è quella strana malattia che fa criticare i comportamenti altrui, salvo poi imitarli e anche nel modo più sbagliato. Nel 2020, ministro Ciriani, quando il ministro Gualtieri diede vita al superbonus, nel quadro con cui noi costruimmo quella misura, scolpito l'impegno che ha appena ricordato il presidente Patuanelli. Quella misura fu fatta in emergenza assoluta, tutte le imprese edili italiane che chiedevano e supplicavano un intervento, come anche tutte le organizzazioni sindacali. Quella misura doveva iniziare nel 2020, in piena pandemia, e doveva concludersi nel 2021. È stata portata avanti, per il dibattito che tutti conoscete, nel 2022 dal Governo Draghi ed è stata prorogata per diciannove mesi da voi. Assumetevene la responsabilità. Le villette unifamiliari con il superbonus sono una straordinaria intuizione di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. Porta la loro firma quel provvedimento del 10 agosto 2023. la responsabilità almeno di guardarvi allo specchio e dire: allora abbiamo fatto male i calcoli; allora, forse, non ci siamo ritrovati. Allora, siccome siete gli stessi che vietano ai loro parlamentari di presentare emendamenti durante la legge di bilancio e siete gli stessi che, non potendo nascondere i numeri, decidono di non scriverli nemmeno, perché è quello che avete fatto nell'ultimo Documento di economia e finanza, abbiate il coraggio di dire che non avete uno straccio di idea di politica economica, che non avete uno straccio di idea di politica industriale e che non avete il coraggio di allargare la base fiscale per ridurre la pressione fiscale. Signor Presidente, ministro Ciriani, lo abbiamo detto più volte al ministro Giorgetti: non si può governare un Paese come l'Italia pensando di non reperire le risorse attraverso la leva fiscale. Se non allargate la base fiscale, non diminuiremo mai la pressione fiscale. Lo avete scritto voi nel DEF che aumenterà dello 0,3 per cento l'anno prossimo, non l'abbiamo scritto noi. Se ora non tornano i conti e se, all'improvviso, l'alibi degli alibi è diventato il superbonus, guardate che, alla fine, finirà come finisce per tutti coloro che non hanno un'idea di Paese. Finirete fuori strada. Questo provvedimento, nel merito del quale voglio entrare e sicuramente ci entreremo domani nel dibattito sul sul voto di fiducia, prevede la ripartizione obbligatoria in dieci anni delle detrazioni. Le detrazioni per spese sostenute nel 2024 relative al superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus sono ripartite in dieci quote annuali anziché quattro e cinque Ma cosa vi hanno fatto i disabili? Cosa vi hanno fatto le persone che hanno bisogno di aiuto? Cosa vi hanno fatto le persone che hanno bisogno del sostegno dello Stato? Cosa vi hanno fatto coloro che ancora non sono usciti dalla crisi legata al sisma? Sapete Sapete perché chiedo cosa vi hanno fatto? Perché, se uno guarda gli interventi in questo provvedimento ed entra nel merito, scopre che ad un certo punto le imprese edili che hanno acquistato crediti anche per effetto dello sconto in fattura continueranno ad utilizzarli in base all'odierna ripartizione in quattro rate. Poi uno guarda le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, per i quali invece viene previsto l'obbligo di ripartizione in sei anni delle quote utilizzabili del 2025 relative ai crediti d'imposta da superbonus e *bonus* sempre per barriere architettoniche e sismabonus, compreso sisma bonus acquisti. Poi ci si rende conto rispetto alle risorse che avevamo chiesto di mettere per le aree che vengono dalla ricostruzione pro terremoto che lì in realtà hanno deciso di ridurre le risorse a 35 milioni. In sintesi, il Governo ha posto gran parte dell'onere del blocco del superbonus sulle famiglie e ha penalizzato in misura rilevante una parte delle banche, mentre per le imprese edili la situazione non è cambiata dal punto di vista formale. Nella sostanza, gli effetti delle misure introdotte complicano ulteriormente la gestione del superbonus e avranno ricadute pesanti sull'andamento dei lavori. Un'altra questione ci preoccupa oltre al divieto di compensazione dei crediti, altro tema per il quale avevamo proposto di trovare una soluzione che consentisse a tutte le imprese che si trovano in gravissima crisi di liquidità almeno di recuperare i crediti che hanno con lo Stato, almeno di compensarli. Proviamo ad andare loro incontro. Anche lì, il no secco del Ministero dell'economia, come se fosse colpa delle imprese avere quei crediti che in realtà avevano un'altra dimensione temporale. Per non parlare dell'insufficienza delle risorse per gli interventi che ho già sottolineato per i territori colpiti dal sisma. Mi riferisco soprattutto a Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, territori che si aspettavano una risposta da questo provvedimento che non arriverà ed è bene che gli eletti e le elette in quei territori ci mettano la faccia e spieghino che, nonostante il voto di fiducia non messo sull'opposizione, ma messo contro Forza Italia, oggi questa era come si vede dai suoi banchi. Ministro Ciriani, mi auguro che vengano domani per il voto di fiducia, altrimenti si apre un problema molto serio. *(Applausi)*. Noi siamo convinti che quel problema lo avrete il 10 giugno, però segnaliamo l'assenza di Forza Italia dai suoi banchi. I senatori di tale Gruppo non hanno partecipato alla discussione, non hanno preso la parola e hanno deciso per il momento di lanciare un segnale questa sera. Vedremo domani. Abbiamo contestato con la collega Tajani e con gli altri colleghi in Commissione finanze l'insufficienza delle risorse per gli interventi per la riqualificazione degli immobili degli enti la vostra incapacità di raccogliere i contributi che sono arrivati, legati al coinvolgimento dei Comuni nei controlli sul superbonus. Anche qui, ai Comuni che effettuano le segnalazioni non viene garantito il riconoscimento della quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative ai tributi statali e alle

il primo anno con le Camere nel pieno della loro vita parlamentare e noi, avendo solo il tendenziale, conosceremo il perimetro dei saldi solo con la nota di aggiornamento al DEF. La scusa utilizzata è stata quella che cambia il ciclo di bilancio in Europa e cambiamo le regole. Come abbiamo già denunciato qui, ministro Ciriani, durante il confronto e il dibattito sul DEF, DEF, non vi venga in mente di modificare la legge sulla contabilità sull'altare della modifica del ciclo di bilancio in Europa, perché quelle modifiche o le facciamo insieme o sarà durissima la nostra reazione. Non vi consentiremo di dare al Ministro dell'economia, a questo Ministro dell'economia, in queste condizioni, la delega in bianco per spostare durante l'anno le risorse da un Ministero all'altro, perché questo non è mai avvenuto e mai consentiremo Lo dico sapendo quello che stiamo percependo. Il ciclo di bilancio è cambiato: le modifiche le faremo, ma le faremo in maniera mirata, chirurgica condivisa, esattamente come le facemmo nel 2016, quando modificammo la legge di contabilità di bilancio e passammo dalla vecchia stabilità alla nuova legge di bilancio con l'80 per cento del voto parlamentare. So che quella del coinvolgimento delle opposizioni che non coltivate, che non avete sulla pelle e nella quale non credete. Ma mi auguro, anche a partire da questo dibattito, che in alcune parti della maggioranza si inizi a percepire la necessità di unire il Parlamento e di non scavare sempre di più dentro questo fossato che non solo allontana noi, perché abbiamo una visione del Paese completamente diversa, ma aumenta anche i contrasti e le contrapposizioni nel nostro territorio. Signora Presidente, termino auspicando per domani un cambio di rotta, che non avverrà. Vedremo se domani Forza Italia sarà presente, come immaginiamo. Ovviamente è stata piegata sull'altare della ragion ragion di superbonus del ministro Giorgetti. Il vice presidente del Consiglio Tajani ha tenuto duro: la lotta di Forza Italia è durata quarantott'ore all'ennesimo voto di fiducia. Avete superato tutti i *record* nei primi diciannove mesi di Governo, sia nel numero di decreti-legge che nel numero di fiducie. Se non fosse una cosa molto seria, potrei farvi un in bocca al lupo; non ve lo farò perché speriamo di mandarvi a casa nel più breve tempo possibile. Lo speriamo per il Paese, lo speriamo per le italiane e gli italiani.

Signor Presidente, so che un collega è già intervenuto su questo argomento, ma tengo a testimoniare la solidarietà del Gruppo Fratelli d'Italia con il primo ministro della Repubblica slovacca, Robert Fico,

Signor Presidente, il 12 maggio scorso si è celebrata la Giornata mondiale della fibromialgia, una patologia a lungo invisibile oppure minimizzata, nonostante da più di trent'anni sia stata inserita dall'Organizzazione mondiale della sanità nella classificazione internazionale della malattia e dei problemi collegati. Questa Giornata nasce quindi per sensibilizzare e invitare a non sottovalutare una malattia fortemente invalidante e che solo in Italia riguarda milioni di persone. La fibromialgia, infatti, è una condizione clinica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico cronico e diffuso, spesso associata a stanchezza, disturbi del sonno, problemi di attenzione e memoria, ansia e depressione. La fibromialgia è più frequente nelle donne rispetto agli uomini e può svilupparsi a qualsiasi età. A livello nazionale si calcola che ne sia affetto fino al 3,5 per cento della popolazione. Lo scorso 29 febbraio alla Camera sono state approvate sei mozioni di tutti i Gruppi politici per riconoscere la fibromialgia come malattia cronica invalidante, nonché per la definizione dei protocolli terapeutici, dello sviluppo dei centri specializzati per la cura e la ricerca, dell'istituzione del registro nazionale presso il Ministero della salute. Accanto alle mozioni vi sono poi addirittura diciotto proposte di legge presentate tra Camera e Senato. Nonostante la forte e trasversale attenzione del Parlamento attorno a questa tematica, il lavoro della competente Commissione del Senato è ancora in una fase di stallo. Serve una robusta accelerazione per dare ai medici, ai ricercatori e soprattutto ai malati il sostegno che non è stato dato per via della costante sottovalutazione di questa malattia. Ed è per questo, Presidente, che proprio in ragione della Giornata mondiale mondiale della fibromialgia, mi rivolgo a lei affinché possa farsi portatore di questo messaggio per una rapida calendarizzazione delle proposte presentate e già esaminate dalla 10a Commissione del Senato, proposte - ricordo - sottoscritte da quasi tutti i Gruppi politici.

nell'Emilia Romagna, in particolare nella Romagna, che ha reagito come sempre, con coraggio e determinazione, senza mai piangersi addosso, e ha ripulito dal fango le case e le aziende del proprio territorio. soprattutto lo straordinario impegno delle nuove generazioni che sono venute con la loro forza e il loro coraggio a supportarci in un momento molto difficile e con gioia hanno dato luce alle giornate buie dei romagnoli. L'azione del Governo, al netto delle passerelle a favore di telecamera, è stata tardiva e inadeguata e ancora oggi molte famiglie attendono sostegni e ristori. Lasciamo stare il primo passaggio di due mesi di attesa per un commissario, cosa che non era mai successa. Lasciamo stare tutto quello che è successo strumentalmente e politicamente, la discussione nata in quella fase. Non era mai successo che una tragedia del nostro territorio portasse a discussioni politiche. Lasciamo stare le azioni che mancano sul territorio, però alcuni dati sono oggettivi ed è importante che questa Assemblea li conosca. Ad oggi, i danni ammontano a 8,8 miliardi, per la ricostruzione pubblica e privata, ed erogati dalla struttura commissariale del Governo, fino ad oggi, siamo a 743 milioni. È passato un anno. Per i privati in particolare, dei 3,5 miliardi cui si faceva riferimento, per il momento sono arrivati, sia dalla struttura commissariale che dal Governo, 304 milioni. Questi sono i dati oggettivi. La mancanza di dirigenti a livello nazionale sul nostro territorio è gravissima. Durante il periodo del terremoto c'erano state quasi 1.200 persone in aggiunta, e adesso siamo a poche centinaia. È soprattutto un appello che lancio all'Assemblea e ai colleghi: facciamo attenzione e continuiamo a presentare emendamenti per inserire i beni mobili all'interno dei ristori. Per il momento non ci sono, e sono presenti solamente i beni immobili, ma l'alluvione non è un terremoto. Quello che è successo nella nostra terra ha portato via alla maggior parte delle persone i beni mobili. Quindi, per l'ennesima volta, facciamo un appello, ad un anno di distanza, per inserire i beni mobili all'interno dei ristori.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

stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria"